Prima di dare la parola per la replica ai senatori Questori, ai quali chiedo che contestualmente esprimano il parere sugli ordini del giorno presentati, vorrei informare l'Assemblea così come meglio spiegherà il senatore Questore Franco Paolo nel suo intervento di replica - nuove ed ulteriori misure di contenimento dei costi del Senato della Repubblica sono state adottate dal Consiglio di Presidenza che si è riunito nella seduta di ieri, al termine dei lavori dell'Aula. Le spese relative all'esercizio del 2011 saranno ulteriormente ridotte per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro, pari all'1 per cento rispetto al 2010. Nuove misure consolideranno il *trend* di riduzione della spesa in misura del meno 1,5 per cento nel 2012, del meno 3,5 per cento nel 2013 e del meno 6 per cento nel 2014, calcolati sul valore storico della spesa del 2010.

Grazie, Presidente.

dove sono indicati i valori dei risparmi che saranno versati al bilancio dello Stato come ulteriormente determinati ieri dal Consiglio di Presidenza.

fornire questo importante contributo al nostro impegno come senatori Questori, che continuerà nell'adempimento delle indicazioni che ci sono state date ai fini della riduzione dei

Grazie, Presidente.

Se dovessi dare un titolo sintetico di taglio giornalistico all'indicazione principale che emerge dai contributi dei colleghi intervenuti (che ringrazio a nome del Collegio dei senatori Questori, sia per le parole di apprezzamento e sostegno espresse riguardo al nostro operato, sia - soprattutto - per i suggerimenti, le sollecitazioni e anche, ovviamente, le inevitabili sottolineature critiche), parlerei di un invito a progettare il cambiamento. Stiamo vivendo un passaggio molto delicato per la vita del Paese e non possiamo sottrarci a una riflessione radicale sul nostro *modus operandi*, che però non si limiti più a generiche promesse o a prospettare in modo vago futuri interventi. Noi tutti siamo chiamati - nell'esercizio della nostra piena autonomia, che è poi responsabilità - a dare risposte credibili e concrete come abbiamo appena sentito dal Presidente e dal collega Franco. Nell'ambito delle proprie competenze, i senatori Questori e il Consiglio di Presidenza si sono mossi nella ferma consapevolezza che, in un difficile momento dell'economia del Paese e nel contesto delle manovre di risanamento tracciate dai decreti-legge n. 78 del 2010 e n. 98 del 2011, i documenti di bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e per il triennio 2011-2013 dovessero essere una doverosa risposta di adesione e d'impegno concreto da parte del Senato. la manovra prospettata, ponendosi in diretta continuità con l'indirizzo già fissato nei bilanci degli anni precedenti, doveva tracciare un percorso di grande rigore per gli anni a venire, dovendo al contempo essere sostenibile, concretamente praticabile, e contemperare tale finalità con l'efficiente funzionamento dell'istituzione parlamentare, dal quale - non dimentichiamolo - dipende il funzionamento della stessa democrazia. È bene ricordare che in effetti questo percorso di attenta gestione delle risorse finanziarie non nasce oggi, ma trae inizio già a partire dal 2006, quando l'incremento annuale della spesa ha cominciato drasticamente a scendere dalle percentuali prossime al 10,2 per cento del 2002 a quelle più modeste del 2,88 per cento, del 2,77 per cento

caratterizzata da un'incisiva - sia pur progressiva - riduzione della spesa stessa. Una fase che non può che essere frutto di un'opera di razionalizzazione strutturale, da portare avanti con l'obiettivo di coniugare rigore finanziario e piena funzionalità dell'organo parlamentare. Si tratta di una sfida impegnativa, che può essere superata con successo attraverso il costante incremento dell'efficienza amministrativa, il ripensamento di tutte le spese, in particolare di quelle che non trovano una *ratio* giustificativa nel diretto rapporto con l'attività parlamentare, nonché attraverso la migliore allocazione Ciò che mi preme sottolineare a tale riguardo è che già nei documenti inizialmente sottoposti all'esame dell'Aula era contenuto questo cambio di marcia, ma in effetti ci siamo resi conto - e a tal fine è risultato senz'altro prezioso il contributo, in termini di stimolo e suggerimenti, di tutti voi, di tutti voi, anche attraverso la presentazione dell'ordine del giorno G100, ampiamente condiviso - che l'assoluta eccezionalità del momento richiedeva uno sforzo aggiuntivo, un segnale più chiaro e deciso che si stava facendo ancora di più sul serio e che si stava ponendo in atto un approccio ancor più rigoroso e incisivo alla gestione delle risorse a nostra disposizione. Tutto ciò è evidenziato anche dalla eccezionalità della procedura che stiamo seguendo, innovando nella prassi del Senato con l'introduzione di una sorta di Nota di variazioni. Questa procedura, infatti, ha consentito correttamente al Consiglio di Presidenza, in considerazione del dibattito svolto in Aula, di adottare fin da subito e all'unanimità le decisioni ritenute opportune, al fine di dare risalto contabile a quello sforzo Per effetto di queste ultime modifiche, si prevede quindi un'ulteriore riduzione, così come abbiamo sentito, rispetto a quella già conseguita dello 0,34 per cento delle spese relative all'esercizio 2011, fino a concorrenza dell'1 per cento, espresso in termini nominali, per un valore complessivo di di riduzione pari a euro 5.952.816 euro rispetto al 2011. Per effetto poi dell'altro impegno contenuto nell'ordine del giorno richiamato, in sede di presentazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 dovremo prevedere interventi chiaramente di natura strutturale, volti a rafforzare nell'entità il *trend* di riduzione della spesa complessiva, per portarlo a valori pari a meno 1,5 per cento, meno 3,5 per cento e meno 6 per cento, rispettivamente, nel 2012, 2013 e 2014, sempre

ai quali, per valutarne l'intera portata, andrebbero sommati gli effetti derivanti dal tasso di inflazione che interverrà nel periodo considerato. Si tratta quindi di obiettivi particolarmente ambiziosi, per mantenere fede ai quali sarà necessario uno sforzo di analisi della spesa e dei meccanismi che la regolano davvero considerevole. Essi dovranno poi necessariamente tradursi in tempi rapidi (non dimentichiamo infatti che i primi effetti andranno contabilizzati già dal prossimo bilancio annuale e triennale) in vere e proprie riforme strutturali, a partire dai principali ambiti di intervento, che mi sembrano tutti richiamati e riassunti nell'ordine del giorno di cui dicevo prima. È questa la sfida alla quale nessuno può sottrarsi. Ma questo, come dicevo pocanzi, è il punto di approdo di un quadro organico di interventi delineati nel corso dell'ultimo anno. Ritengo perciò doveroso provare il percorso compiuto, che si compone di vari momenti. Il primo *step* è caratterizzato dalle misure proposte dal Collegio dei senatori Questori, d'intesa con il Presidente, in varie riprese, approvate dal Consiglio di Presidenza (dapprima il 7 giugno e poi il 26 luglio), quindi calate nel bilancio presentato Voglio ricordarle in breve, partendo dalla decisione di bloccare, per il triennio, la crescita della dotazione ordinaria, mantenendola al livello del 2010, conseguendo per tale via già un primo consistente risparmio per il bilancio dello Stato pari a circa 50 milioni di euro. Ciò significa che le risorse finanziarie a Ciò significa che le risorse finanziarie a disposizione del Senato nei prossimi anni, alla luce delle previsioni relative al tasso di inflazione medio atteso per gli anni 2010-2013, si ridurranno del 10 per cento. Si tratta per il Senato di un vincolo così stringente sul versante delle entrate (rispetto alle quali la dotazione costituisce l'88 per cento), che, inevitabilmente, le spese, le quali, com'è noto, rispondono in larghissima parte a dinamiche di crescita obbligatoria, dovranno essere contenute almeno nella stessa misura. È all'interno di questa cornice che è stato calibrato il quadro programmatico degli interventi di risparmio da effettuare. I settori di intervento sono noti. Sul versante del trattamento economico dei parlamentari

blocco degli adeguamenti contrattuali e la non applicazione dell'aumento del 3,2 per cento riconosciuto ai dipendenti della noi non ci siamo iscritti al *club* della gara a chi è più bravo fra Camera e Senato (ovvero: ognuno faccia quel che può quando non c'è materia comune), ma se citiamo il dato è per un rispetto doveroso nei confronti dei nostri dipendenti, la quasi totalità dei cui sindacati, con grande senso di responsabilità, ha sottoscritto con la Rappresentanza guidata dalla senatrice Mauro il congelamento di tali adeguamenti, che erano previsti in base ad una norma di salvaguardia. Sullo stesso contributo responsabile contiamo anche nella fase che si apre ora

agli stanziamenti di bilancio a carattere non vincolato, rispetto ai quali sono previsti risparmi derivanti dalla dematerializzazione degli atti parlamentari e dalla dismissione di locazioni e da contratti di utenze. Non sono interventi di poco conto, se si pensa che il loro importo complessivo porta, tra riduzione delle spese ed entrate, ad un totale di 120 milioni di euro fino al 2014. Corre l'obbligo di precisare che, per quanto riguarda i risparmi da versare al bilancio dello Stato ai sensi dei due decreti citati, la struttura del documento di bilancio si è dovuta in qualche modo adattare alle disposizioni di legge, computando e rappresentando come "spesa effettiva" somme che si configurano sostanzialmente come "tagli" e "risparmi". Appare corretto quindi a mio avviso computarli nella sostanza come tali. Tuttavia, va precisato che tale pacchetto di misure non si esauriva qui. I senatori Questori - lo ha già detto il senatore Questore Franco nella sua relazione iniziale - avevano già assunto l'impegno di proporre al Consiglio di Presidenza, in tempi assai rapidi, processo di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa. Quanto ai primi, è evidente che occorre intervenire, d'intesa con la Camera dei deputati, a rivedere istituti attinenti alle competenze dei parlamentari in genere. È noto peraltro che l'intervento riguardante le indennità, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2011, richiede una modifica legislativa; tuttavia, appare opportuno che i due rami del Parlamento rivendichino su questa materia una piena autonomia, non solo formale, nelle decisioni da assumere in modo responsabile e non eterodiretto. Allo stesso modo occorre poi rivedere l'istituto del vitalizio attraverso una riforma, da realizzarsi avendo al riguardo un doveroso sistema di valorizzazione della contribuzione e fermi restando i diritti acquisiti. Non dobbiamo dimenticare peraltro Il processo di riduzione del trattamento complessivo dei senatori al fine di partecipare al generale sforzo di riduzione della spesa pubblica è partito con la legge finanziaria 2006 (con cui l'importo dell'indennità parlamentare è stato ridotto è poi successivamente proseguito con la legge finanziaria 2008 (che ha bloccato per cinque anni gli incrementi dell'indennità spettanti a diritto vigente, dal 2008 al 2012, con effetto anche sui vitalizi). Non si dimentichi inoltre che nel 2007 è stata approvata una riforma degli assegni vitalizi, che ha sensibilmente ridotto la misura di tali prestazioni e ha raddoppiato il periodo minimo di mandato richiesto per maturare il diritto all'assegno vitalizio. in tempi ravvicinati le nostre competenze economiche non deve farci perdere di vista un dato: il trattamento economico dei parlamentari, nel complesso, è concepito come condizione dell'esercizio indipendente di una fondamentale funzione costituzionale e, al tempo stesso, come garanzia che tutti i cittadini, senza riguardo al patrimonio o al reddito, possano realmente concorrere alle elezioni delle Camere. Ho fatto poi accenno alla riorganizzazione amministrativa. In effetti, sul versante della spesa obbligatoria l'obiettivo del controllo sugli andamenti della spesa é affidato anche ad un piano di riduzione dell'organico in un quadro di riorganizzazione dell'Amministrazione. A tale riguardo, A tale riguardo, non posso mancare di sottolineare che, se negli anni 2001-2005 si è registrato un deciso aumento del personale (passato da 869 a 1.100 unità), l'inversione di tendenza si è potuta realizzare solo a partire dal 2006, per arrivare, oggi, ad una consistenza numerica di 952 unità. Ed è previsto che questo *trend* continui, stante il blocco del *turnover*. Ecco perché ritengo utile soffermarmi un attimo sul tema della riorganizzazione, che è stato toccato anche in alcuni ordini del giorno e interventi. Dopo un decennio dall'approvazione della riforma organizzativa del 2001, appare venuto il tempo di operare una ricognizione sulla rispondenza del progetto fatto allora. Sono passati molti anni, ci sono state forti innovazioni anche nel modo di lavorare (ad esempio esternalizzazione e devoluzione di molte attività), vi è stato un forte impulso alla informatizzazione delle attività, sia amministrativa che parlamentare (anche con effetti di sinergie ed economie in termini di fabbisogno di risorse di personale). Più in generale, si è registrata un'evoluzione delle funzioni del Parlamento, sia nei mutati rapporti di fatto con il Governo, sia nell'ambito di un contesto di produzione normativa multilivello (Regioni, Stato, Unione europea). Occorre interrogarsi sulle ricadute organizzative di questa evoluzione. Ma oltre a ciò, si tratta di interrogarsi sulla validità e l'efficacia di scelte organizzative fatte in passato, nonché dei principali processi amministrativi di supporto all'attività istituzionale, analizzandone i costi/benefici e, conseguentemente, fissando precise strategie di intervento, in grado di produrre effettivamente la riduzione degli organici prevista in decisioni del Consiglio di Presidenza, ma garantendo al tempo stesso gli usuali standard dei servizi di supporto all'attività parlamentare. Ecco quindi la sfida che siamo certi l'Amministrazione del Senato saprà del Senato saprà affrontare: approntare un rigoroso piano di riduzione della pianta organica in un quadro di riorganizzazione da definire in modo da costruire un modello organizzativo che, a fronte dei risparmi ottenuti, sappia garantire un elevato livello dei servizi. In tale contesto si inseriscono diversi interventi dei colleghi, che come noi avvertono anche la necessità di operare per dare vita a forme di cooperazione strutturata tra le Amministrazioni delle due Camere, anche alla luce dei passi concreti che sono stati stati già compiuti in qualche settore, ad iniziare dalla realizzazione del polo bibliotecario e dagli interventi in ordine alle segreterie delle delegazioni parlamentari presso gli organismi internazionali. L'idea fondante deve essere quella per cui - fatta salva l'esigenza di assicurare l'assoluta indipendenza e parità di poteri di ciascuna Camera nella fase della deliberazione - è ragionevole ricercare sinergie sempre più forti nella fase anteriore, quella conoscitiva, nonché in tutte le attività nelle quali il Parlamento si presenta La questione è sollevata anche in diversi ordini del giorno e, più dettagliatamente, nel G2 a firma del senatore Grillo, al quale risponderà compiutamente il collega Cicolani. Tengo solo a sottolineare, in merito, che oggi è necessario compiere un balzo in avanti su questa strada al fine di garantire una maggiore funzionalità

di ciascuna Camera, si deve pertanto procedere per ricercare intese volte a definire nuove ed ulteriori forme di collaborazione, integrazione e unificazione tra le attività delle due Amministrazioni. Queste innovazioni di natura organizzativa dovrebbero poi accompagnarsi ad un processo di omogeneizzazione delle norme che regolano il personale

il ricorso a consulenze copre funzione di supporto diretto all'attività politica non di competenza del personale del Senato. Quanto poi all'aspetto, sottolineato negli ordini del giorni dei senatori Giaretta, Astore, Lannutti e nell'intervento della collega Leddi, concernente il sensibile incremento della spesa per le segreterie esso è da ascrivere alle modifiche normative introdotte da deliberazioni del Consiglio di Presidenza del dicembre 2009 e del 2010 che hanno disposto, in primo luogo, l'introduzione della possibilità che i collaboratori delle segreterie particolari - così come avviene da lungo tempo presso l'altro ramo del Parlamento

Tale sostanziale innovazione, sollecitata da autorevoli componenti del Consiglio di Presidenza allo scopo di offrire una maggior tutela al lavoratore, ha determinato l'innalzamento considerevole degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione (l'aliquota contributiva INPS a carico del datore di lavoro è più elevata, e a ciò deve aggiungersi il costo relativo In secondo luogo, le modifiche hanno comportato l'istituzione di dotazioni di segreteria per Presidenti di organi che ne erano sprovvisti: Commissione contenziosa, Consiglio di garanzia, Consiglio di disciplina. Ciò ha determinato un conseguente maggiore onere. Mi sia consentito infine di fornire

di ogni settimana, viene riproposta attraverso un progetto grafico dedicato il resoconto dell'attività parlamentare svolta dall'Aula e dalle Commissioni e la presentazione delle attività culturali ed istituzionali promosse dal Senato. Durante la pausa estiva è prevista la messa in onda di contenuti che riprodurranno in particolare le iniziative realizzate dal Senato per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Verranno anche utilizzati materiali messi a disposizione dall'Istituto Luce e dalla RAI. Verranno riproposte le principali iniziative istituzionali svoltesi nell'Aula di Palazzo con la riproposizione delle iniziative promosse dal Senato nell'anno 2011 rivolte ai giovani, nonché il resoconto dell'attività legislativa. Si tratta ovviamente di un primo passo, senatore Mascitelli, realizzato a costo zero - ci tengo a dirlo - dall'Ufficio stampa, che merita di essere ringraziato per l'iniziativa volta a rendere il canale satellitare un sempre più valido strumento di comunicazione istituzionale e di trasparenza dell'Istituzione. Dicevo, progettare il cambiamento: tutto questo si può fare se, cercandone la strada, non prendiamo scorciatoie, soprattutto in momenti come questi dove la risposta al solo percorso mediatico confonde inevitabilmente gli sforzi fatti sul concreto. Ecco perché le regole da esercitare sono ancora di più quelle della trasparenza. Insieme alla riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa, di cui ho detto, occorre la riforma delle disposizioni sul bilancio, con la possibilità di prevedere un bilancio pluriennale che traguardi, così come evidenziato dal dibattito, un orizzonte più vasto e una programmazione funzionale delle spese e degli interventi, la possibilità di dividere ed evidenziare dettagliatamente le singole poste che riguardano spese direttamente connesse al funzionamento delle Istituzioni e quelle di natura previdenziale. Mai più un preventivo nel preventivo, ha ragione il senatore Mercatali, e l'obiettivo, a partire dal prossimo anno, di presentare, discutere ed approvare nel mese di marzo il consuntivo 2011 e il preventivo 2012 rappresenterà un altro passo in avanti sulla credibilità degli impegni presi in quest'Aula.

Molti colleghi intervenendo si sono preoccupati dell'onorabilità del senatore, altri della sua dignità; a noi, Questori del Senato della Repubblica, spetta di preoccuparci di seguire scrupolosamente i nostri compiti, compiti, dettati soprattutto dalle linee guida assegnateci, senza cadere nella trappola di chi, parlando di responsabilità, pensa sempre a quella degli altri e mai a cominciare ad esercitare la propria. A noi interessa, certamente, l'onorabilità dei nostri senatori, ma soprattutto che rimanga sempre alta l'onorabilità del Senato della Repubblica italiana.

In relazione agli ordini del giorno presentati, dichiaro inammissibile l'ordine del giorno G30, a firma del senatore Belisario e altri senatori, il quale, nel prevedere la soppressione di misure a favore di ex parlamentari che costituiscono ormai un diritto quesito, si pone in contrasto con i principi generali dell'ordinamento e con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Signor Presidente, inizio con l'ordine del giorno G100, a firma dei senatori Gasparri, Finocchiaro, Bricolo, Sbarbati, Viespoli e Baio,

occupato l'Aula in questi giorni, e su cui esprimo parere favorevole. Tale parere favorevole ovviamente influenza

coerente e compatibile. Ricordo brevemente che questo ordine del giorno tiene conto della riduzione di circa 6 milioni di euro, operata a valle del dibattito dal Consiglio di Presidenza nella serata di ieri, e della auspicata riduzione

della coerenza con l'ordine del giorno G100. In particolare, chiederei - e questa è una richiesta di carattere generale

dire credibilmente se si riesca a ridurre di una certa percentuale una determinata spesa senza un'analisi approfondita.

Il nostro Paese, ad oggi, ha scelto un'altra strada: quella del *forfait* per l'attività di supporto dei parlamentari, ritenendo - e forse, stando ai dati che sono stati riferiti dal senatore Malan nel suo intervento, ha avuto ragione il legislatore - che questa scelta forfetaria fosse congruente congruente e coerente con un'idea di minore spesa dell'attività parlamentare. Quindi, finché non verrà modificato questo aspetto, il parere su questi ordini del giorno non può che essere contrario.

Senato sono 14: si tratta di un numero abbastanza modesto, e sufficiente soltanto per l'utilizzo istituzionale del parco mezzi.

una reiterazione di un testo diverso. nonché un opportuno adeguamento e definizione delle norme che regolano l'attività e il trattamento del personale. Anche tale principio della rivisitazione dell'organizzazione del personale è espresso nelle sulla ridefinizione delle norme che regolano l'attività e il trattamento del personale si danno delle indicazioni molto più complesse.

legge. Credo che la legge sull'anagrafe patrimoniale non escluda l'utilizzo di Internet: non lo prevede, ma nemmeno lo esclude. In ogni caso, per non addentrarmi in una vicenda che è già stata discussa a lungo, con l'espressione «con riferimento ai singoli componenti del Senato», si possa aggiungere «su base volontaria», ovvero che gli uffici predispongano tale possibilità di trasparenza per tutti i senatori che lo

prendo atto di questa riformulazione. A questo punto però, siccome il suo ordine del giorno non tocca solo l'aspetto dei parlamentari ma è articolatissimo e riguarda anche altri aspetti,

Presidente, l'ordine del giorno G30, che lei ha dichiarato inammissibile,

dell'ordine del giorno G17 dichiarato ammissibile lo scorso anno nella seduta del 21 settembre 2010, che è stato poi votato e respinto. Allora, mi chiedo se questa prassi viene interpretata *ad libitum*, oppure, a seconda delle circostanze di tempo e di spazio,

Presidente, sono molto preoccupato da questa decisione, e il Gruppo dell'Italia dei Valori, che ha

G100, non sono stati chiamati tutti, per poterlo condividere o meno. La pregherei pertanto di far sì che questo dibattito abbia delle regole un po' diverse, non quelle classiche che prevedono solo dichiarazioni di voto, al unire alla dichiarazione di voto anche un nuovo intervento - per chi lo vuol fare - relativamente al merito del bilancio. Questo credo sia corretto, senza voler intralciare minimamente

Contrariamente alle mie abitudini, questa volta dovrete accettare la mia lentezza, che vuole essere commisurata alla doverosa attenzione, virgola per virgola,

pensavamo che non ci fosse bisogno di un ordine del giorno per ribadire che gli articoli 3 e successivi di tale regolamento interno del Senato dovessero essere rispettati.

convertito, nell'articolo 1 e negli articoli successivi, in particolare il 4, sulla sospensione dei *benefit* per gli ex Presidenti del Senato, deve essere tenuto in consiferazione.

sul riordino della disciplina delle indennità parlamentari, la tempistica era stata posta, ed era a partire dall'inizio della prossima legislatura, mentre nell'ordine del giorno G100 si lascia tutto sul vago, nel senso che si fa riferimento ad un'intesa con l'altro ramo del Parlamento.

delle valutazioni critiche e delle proposte avanzate nel corso del dibattito, molto intenso, che abbiamo sviluppato sul progetto originariamente presentato dal Consiglio di Presidenza stesso. fino al punto di presentare, per il momento della decisione che sta per giungere, proposte modificative, variazioni del progetto originario che recepiscano le indicazioni di fondo contenute nell'ordine del giorno unitario che è stato elaborato attraverso un lunghissimo lavoro, per il quale credo debbano essere ringraziati tutti e in particolare il Presidente della Commissione bilancio, che lo ha coordinato. che in particolare, anche per la comunicazione esterna, valorizzerei molto un dato che emerge con chiarezza, se esaminiamo il quadro comparativo tra la previsione della spesa dello Stato e la previsione della spesa del Senato della Repubblica, così come emerge dalla tabella della penultima pagina del nostro progetto di bilancio. Signor Presidente, nell'anno nell'anno finanziario 2011, laddove si documenta che la spesa complessiva dello Stato si riduce in cifra assoluta rispetto all'anno finanziario 2010, 2010, prima della variazione introdotta sulla base dell'ordine del giorno, emergeva uno scarto tra il livello di riduzione della cifra assoluta della spesa dello Stato nel suo complesso e il livello di risparmio realizzato dal Senato, rispetto al 2010. PRESIDENTE. Non eravamo in sintonia. MORANDO *(PD)*. Esatto. Era una disparità particolarmente grave, a mio giudizio, sotto il profilo politico e per il rapporto tra il Senato della Repubblica e il Paese. Quelle decisioni di riduzione della spesa nel campo della sanità, della scuola, dell'organizzazione della sicurezza e così via, che il Senato della Repubblica aveva deliberato per la spesa totale dello Stato,

l'uno contro l'altro («È colpa di voi che avete governato prima», «No, è colpa di voi che governate adesso») ma attraverso un confronto di merito, si sia arrivati a determinare per il 2011, addirittura in corso d'opera, una scelta più coerente con l'obiettivo di impegnare il Senato in una riduzione in cifra assoluta analoga a quella imposta alla spesa dello Stato nel suo complesso e a definire - ciò che più rileva

se non riusciremo a prevedere davvero - ed è un impegno molto serio per il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei senatori Questori - un bilancio pluriennale impegnativo, non potremo realizzare gli obiettivi quantitativi che sono fissati nell'ordine del giorno; il contrario avverrà se invece procederemo immediatamente

gli obiettivi che abbiamo fissato per la spesa totale dello Stato per i prossimi anni. Li riassumo molto rapidamente. Per realizzare l'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio al 2014, come sanno i colleghi, la spesa nominale delle pubbliche amministrazioni non potrà più crescere, cioè dovrà mantenersi uguale a quella del 2011. Con questo ordine del giorno fissiamo invece per la spesa totale del Senato obiettivi di riduzione particolarmente significativi, che addirittura, al netto dell'inflazione, raggiungono il 6-7 per cento complessivo rispetto al bilancio del 2010. Ne consegue che la «cura dimagrante» che imponiamo al Senato, rispetto alla «cura dimagrante» assolutamente indispensabile che imponiamo alla spesa totale delle pubbliche amministrazioni, è assai più rigorosa e più severa.

Sostanzialmente il dibattito di ieri sera, che poi è sfociato in un Consiglio di Presidenza, nasce dalla presentazione di un ordine del giorno dell'opposizione che fissava obiettivi abbastanza rigorosi, a volte anche pseudo-draconiani, ma che dava un indirizzo e un segnale di svolta. Su questa presentazione si è attivata una serrata, ma responsabile, trattativa con la maggioranza, che è sfociata nell'ordine del giorno G100, che io apprezzo.

spesa pubblica e si è dato per gli anni a seguire addirittura obiettivi ancora più rigorosi, in maniera tale da essere sempre più da esempio nei confronti dei cittadini. Se, come diceva bene lei, il Senato ha approvato delle leggi di riduzione della spesa pubblica, intervenendo anche su settori strategici del nostro Paese, privandoli in tutto o in parte dei finanziamenti pregressi, era un paradosso che non facesse altrettanto per il contenimento delle proprie spese. Quindi, piena condivisione del suo intervento e un ringraziamento personale per averlo spiegato anche a

vorrei ricordare ai colleghi intervenuti prima che più di una volta ci lamentiamo del fatto che al Senato non viene data la possibilità di incidere sulle leggi che ci passano sotto il naso, se non per dire semplicemente «sì» o «no».

in questo senso noi aderiamo convintamente all'ordine del giorno G100, al quale peraltro anche l'Italia dei Valori ha partecipato con un contributo che è stato comunque apprezzato e definito positivamente nell'accoglimento di diversi ordini del giorno da essa presentati.

Il primo motivo, come ho già detto durante la discussione generale, è l'assurda, ipocrita, mistificatoria operazione mediatica che tende a definire costi della politica il bilancio del Senato, piuttosto che quello della Camera. Questo serve semplicemente a creare un polverone mediatico che va a coprire i veri costi della politica, che sono i 40, 50, 60 miliardi di euro all'anno di cui la Corte dei conti ci parla da anni nella sua relazione ufficiale. La responsabilità di ciascun senatore è indicare e tagliare quei costi della politica, e la responsabilità per il bilancio del Senato è comunicare che il bilancio vero del Senato è attorno a 400 milioni di euro all'anno, pari al 5 per mille del totale della spesa pubblica. La nostra responsabilità non è tanto nel tagliare, anche doverosamente, quei 400 milioni: la nostra responsabilità politica è nel tagliare i 40, 50, 60 miliardi di euro di malversazioni. con lo *spread* con i *bund* tedeschi che è andato oltre i 400 punti base, francamente prima votiamo questo bilancio meglio è, per poterci occupare delle cose vere e serie che interessano 60 milioni di cittadini. La seconda motivazione, signor Presidente, è che, detto delle quantità irrilevanti, la qualità contiene tre argomenti seri che

perché a sedici anni dalla riforma pensionistica Dini, che applica con grande lentezza nel tempo il *pro rata* ed il passaggio al sistema contributivo e che si applica a tutti i cristiani e non cristiani di questa Repubblica, ancora Senato e Camera applicano il metodo retributivo? E su questo abbiamo presentato un preciso ordine del giorno tendente a far sì che, fatti salvi i diritti acquisiti, almeno dall'anno prossimo si applichi agli ex senatori e agli ex dipendenti del Senato la riforma Dini, come per tutti gli altri normali cittadini. secondo argomento, altrettanto poco incisivo nell'ordine del giorno, è ciò che riguarda, sempre nella irrilevanza macroeconomica delle quantità, le spese di manutenzione, terza ed ultima questione la voce più rilevante del bilancio del Senato sono le risorse che vanno ai Gruppi, risorse che come sappiamo creano, tra l'altro, delle distorsioni, perché ci sono condizioni pregresse che garantiscono alte retribuzioni e addirittura portano ai Gruppi un fardello di risorse superiori al costo delle stesse retribuzioni e altro personale che invece essi sono costretti a far lavorare in condizioni di retribuzione piuttosto inique. Per queste due ragioni, la mistificazione sui costi della politica e i tre specifici argomenti che, nonostante la quasi unanimità, nell'ordine del giorno sono indicati vagamente, mentre negli ordini del giorno che abbiamo presentato noi sono puntuali e specifici, dichiaro ancora la mia astensione su questo ordine del giorno. Il che non mi preclude ovviamente di votare a favore del bilancio del Senato così come i senatori Questori lo hanno presentato, per le motivazioni che ho già detto.

ma credo che nel compromesso ci dovessero entrare un po' tutti, soprattutto coloro che erano intervenuti nel dibattito e che credo avessero portato alcune idee.

innanzitutto quella fretta improvvisa che avete avuto ieri sera - non so perché - quando si poteva fare da tanto tempo un discorso con molta serenità; e ci vedo una mancanza di impegni temporali.

Credo che quando si fa un accordo, quando si decide di fare una determinata cosa, debbano essere scanditi anche i tempi, perché di queste promesse credo che questo Parlamento ne abbia sentito parlare tante e tante volte. Secondo punto: ci mancano, signor Presidente, tante cose richieste anche da semplici senatori. La tutela del senatore la si fa con la buona comunicazione, signor Presidente.

Non dobbiamo risparmiare perché ci attaccano: dobbiamo risparmiare perché le spese del Senato e della Camera si sono ingigantite - l'ho affermato e lo affermo oggi - negli anni per colpa di tutti i partiti.

noi facciamo degli sforzi. Ma avremmo dovuto farlo indipendentemente, signor Presidente, dalla crisi. Saremmo dovuti intervenire perché ormai la spesa è arrivata a livelli insopportabili. Quando si dice che ridurremo il personale, signor Presidente,

E allora, a proposito del personale, perché non date delle risposte? Soprattutto sugli organi istituzionali, signor Presidente. È giusto che non si ponga oggi il problema di modifica del Regolamento su alcuni argomenti? È giusto che i Gruppi siano 8, oggi?

senatore Adragna, è vero che l'aumento del personale corrisponde alla sistemazione legale del personale? È vero, però una riflessione la dobbiamo fare. Il Senato un milione in più nel proprio bilancio per una sistemazione in base ai contratti di ordine nazionale, ma è giusto che si abbiano che si abbiano tante spese nel Consiglio di Presidenza per le proprie segreterie? Credo di no e che vada rivisto, senza punizioni, senza voler metterci il cilicio, perché è giusto che il Senato abbia una propria pianta organica e un proprio metodo di lavoro. Se però si fanno assunzioni e poi magari qualcuno sta da altre parti, credo che una riflessione la dobbiamo assolutamente fare. Chi ha parlato di finanziamento surrettizio, alcune volte da parte di alcuni partiti, credo abbia detto la verità e, per carità di Patria, non voglio andare oltre. Lo stesso dicasi per i cosiddetti deliberati

Senza voler penalizzare nessuno, chiedo: è giusto che i Gruppi guadagnino sul personale deliberato? Credo di no.

mi hanno rivolto. In questo ordine del giorno sono contenute, viste in coordinamento tra loro, due importantissime modifiche rispetto anche al calcolo dei cosiddetti tendenziali del bilancio pubblico. Sono espressi due principi fondamentali che si rilevano in due espressioni. La prima è quella relativa alle riduzioni rispetto al valore nominale, quindi al valore assoluto: riferimento alla spesa tendenziale, ma consideriamo il valore assoluto, quindi le riduzioni sono non solo effettive, ma anzi superiori a quelle indicate dalla percentuale, perché scontano l'inflazione. Questo principio è ulteriormente rafforzato dal secondo, quello cioè della introduzione del metodo cosiddetto *zero-base.* Che cosa significa? Che nessuna spesa, di per sé, viene assunta l'anno successivo come trascinamento dell'anno precedente. Questi sono sue due principi assolutamente necessari. Perché è importante il metodo *zero-base*? Perché, signor Presidente, aderendo anche ad una sua indicazione,

dell'unico modo che abbiamo visto in questi tempi di tagliare le spese, quello dei tagli lineari. Abbiamo cioè introdotto un principio di riferimento alla spesa nominale senza trascinamenti, e questo è stato corroborato dal metodo *zero-base,* che significa la possibilità di di verificare ogni anno, direi posta per posta, il bilancio che ci viene illustrato. Ciò significa che le riduzioni di spesa potranno essere orientate

del giorno. Come sapete, la Presidenza non ha contingentato i tempi. È evidente che lascerò libertà di intervento a chiunque; sta alla vostra capacità di articolazione e di gestione

trasformare quest'ordine del giorno - che noi consideriamo qualificante - in raccomandazione ne snatura completamente la funzione, per le due seguenti

tutto ciò che è aggiuntivo o integrativo va bene. La richiesta più specifica, per quest'ordine del giorno G26 e per il successivo G36, è invece di procedere alla votazione per parti separate, disgiungendo la premessa

dice che il Senato si impegna, ad esempio, «a riorganizzare i servizi di ristorazione e barbieria, prendendo in considerazione modalità di ripartizione dei costi diversi da quelli attuali». Poi, arriviamo a votare l'ordine del giorno G26 che invece dice che i costi vanno ridotti comunque del 50 per cento. Come è possibile? Abbiamo già votato in merito ai servizi. Mi chiedo come sia possibile votare tre cose diverse.

Presidente, *ad adiuvandum* rispetto a quello che diceva la senatrice Bonino, a me pare di avere ascoltato (e ho ascoltato con molta attenzione) che nel momento in cui i senatori Questori hanno espresso il parere,

Presidente, francamente sono un po' meravigliato da questa discussione, da ultimo dall'intervento del senatore Bruno. La votazione per parti separate della premessa e del dispositivo si è sempre fatta: costituisce una prassi correntissima e normalissima. Nel caso di specie, vorrei poter dire che noi abbiamo qualche difficoltà di condivisione

Mascitelli. Ritengo che le istituzioni e la politica si difendano anche con la sobrietà, l'austerità e la trasparenza. Non ho difficoltà ad affermare che vi sono voci di bilancio

che almeno noi - e non parlo del Paese - avremmo il diritto di conoscere e che invece non riusciamo a conoscere neanche noi. Allora, si potrebbe fare di più, si potrebbe risparmiare e anche in questo modo si potrebbe riuscire a riaffermare il primato della politica. Io non mi vergogno di fare parte di quella che è definita l'odiata casta, rispetto alle ultra-caste che dettano ordini alla politica!

"Il link apre una nuova finestra"). Tra l'altro, senatore Franco, lei ricorderà che in occasione della riunione che si è tenuta nel Consiglio di Presidenza, la senatrice Baio aveva già chiarito questa posizione, cioè che avrebbe mantenuto in vita alcuni ordini del giorno

accettando le considerazioni del collega Baldassarri, resta la posizione contraria del Collegio dei senatori Questori, in quanto, nella discussione fatta insieme agli altri Gruppi politici, anche il tema dei vitalizi è stato compreso nella rivisitazione della complessiva indennità parlamentare. Attività di supporto e vitalizi sono stati messi insieme nell'articolo 1 della manovra, e quindi quindi seguono un loro binario a partire dall'inizio della prossima legislatura. 2012 le conclusioni di questo lavoro ci sembra inappropriato, per cui resta il parere contrario.

Presidente, non entro nel merito del problema della preclusione, perché comunque abbiamo votato precedentemente un ordine del giorno sul vitalizio. Certamente Certamente accetto questa riformulazione, prendendo atto che in effetti una parte dei contenuti, sia pure in forma più generica, erano ripresi dall'ordine del Abbiamo effettivamente raggiunto dei risultati importanti. Dal punto di vista del bilancio, si sono definiti un quadro economico e un sistema di procedure che sono un passo in avanti notevole rispetto alla

l'esercizio 2011 è stato realizzato - e non si poteva fare diversamente, visto il tempo limitato - attraverso un prosciugamento dei fondi di riserva, sia in parte corrente che in parte capitale. Nell'immediato non si poteva che fare così, ma mi auguro che il Collegio dei senatori Questori trasferirà questo risparmio in voci effettive di bilancio.

sono riflessi immediati anche sui costi di funzionamento del Senato. Prendo atto altresì del suo impegno a sostenere l'idea che il lavoro delle Commissioni ha pari dignità di quello

perché chi le parla, come voi, ha tanto lavorato in Commissione e ha sempre avuto a cuore la significatività e l'importanza del lavoro in quella sede e della presenza in Commissione dei componenti.

Presidente, nel cogliere con favore sia i principi esposti nell'ordine del giorno G6 del collega Giaretta che il suo impegno ad addivenire a una svolta rispetto all'organizzazione del lavoro parlamentare in Aula e nelle Commissioni, vorrei farle presente che di fatto non ci possiamo limitare a esprimere un parere o un voto soltanto sull'ultimo capoverso, là dove si afferma: « a prevedere una modalità di erogazione in modo proporzionale alla presenza in Aula e nelle Commissioni di appartenenza, operando la totale ritenuta nel caso di assenze superiori al 50 per cento». Spesse volte, infatti, proprio perché non c'è un'organizzazione efficiente del lavoro delle Commissioni, le stesse Commissioni alle quali noi apparteniamo si sovrappongano, talché siamo obbligati a decidere se partecipare a una o ad un'altra.

con l'approvazione dell'ordine del giorno G100 e confermo il ritiro dell'ordine del giorno G5 per dare modo alla Presidenza e al Collegio dei senatori Questori di affrontare e risolvere le delicate questioni tecniche che si pongono per la ristrutturazione del contributo del Senato ai Gruppi, di cui al capitolo 1.08, e in particolare la voce di

01.08.02, almeno un milione e mezzo potrebbe e dovrebbe essere tagliato immediatamente. che, per 12 ex dipendenti dei Gruppi estinti, il Gruppo Misto ha ricevuto fino ad oggi mediamente 10.000 euro al mese di rimborso forfetario,

sono persone che da anni non mettono piede in Senato o in uffici collegati al Senato e ciò nonostante continuano a ricevere dai Gruppi stipendi di livello medio-alto, come è testimoniato dall'entità di questo rimborso. Ora, immagino che il Gruppo Misto avrà proceduto o procederà al più presto al recesso dal rapporto di lavoro con queste persone, ma è comunque certo che tra di esse e il Senato non intercorre alcun rapporto, né di lavoro né di altro genere. Quindi il milione e mezzo erogato dal Senato come rimborso al Gruppo Misto per almeno dodici di questi rapporti di lavoro non può avere più alcuna ragion d'essere. Colleghi, se non siamo capaci di tagliare neppure una spesa come questa, della quale è evidentissima l'inutilità e addirittura la grave ingiustizia sociale, non possiamo essere credibili quando annunciamo misure di riduzione della spesa pubblica, riferite ad altre amministrazioni, enormemente maggiori per entità e di attuazione ben più difficile. Collega Azzollini, se non siamo capaci di eliminare questo milione e mezzo, come la mettiamo con il metodo *zero-base*? Al mio intervento su questo punto del 22 giugno ha dato una risposta, e molto incisiva, solo il Presidente del Gruppo Misto; non la Presidenza del Senato, non il Collegio dei senatori Temo che non mi risponderanno neanche in questa sede, ma avverto che al silenzio della Presidenza e del Collegio dei senatori Questori non corrisponderà da parte mia una rinuncia a tenere sotto osservazione questa voce di spesa e a chiedere in proposito una piena trasparenza.

che tanto effetto negativo hanno prodotto in termini di politiche economiche: niente rigore, freno alla crescita, iniquità sociale - nel piccolo del bilancio del Senato, nella microeconomia del bilancio, abbiamo indicato tre precise aree di contenimento. Tra queste, c'è proprio quella dei trasferimenti ai Gruppi parlamentari,

affermata nel G100 e confermata adesso. Questa è l'unica motivazione per cui invece rifiutiamo di dare una risposta nel senso

confermo la richiesta di votazione. Ho detto prima che sul bilancio è stato fatto parecchio. Penso si dovesse fare di più. Sono certo che saremo costretti a fare di più, di fronte al quadro generale. Qui il tema non è una una richiesta di riduzione di spesa. Il contributo ai Gruppi è circa il 6 per cento del bilancio, è stato comunque contenuto di un punto e mezzo quest'anno, ed è una delle condizioni della parità tra Governo e Parlamento e tra maggioranza ed opposizione. Tuttavia, si tratta di una cifra rilevante - appunto il 6 per cento circa del totale delle spese di bilancio - e sono denari pubblici attualmente, quando escono dalle casse del Senato ed entrano nelle casse dei Gruppi, per un incomprensibile miracolo diventano denari privati, senza alcun dovere di rispondere all'opinione pubblica di come vengono impegnati. Faccio presente che questa è una grave anomalia, perché, sul contributo elettorale che ricevono, i partiti hanno obblighi di rendicontazione all'opinione pubblica, di trasparenza e di pubblicità. Non è possibile immaginare che fondi pubblici così rilevanti vengano

di trasparenza e di informazione dell'opinione pubblica. Non capisco perché non lo si debba fare, visto che ognuno di noi appartiene ad un partito politico che è soggetto a queste regole, quando tratta i dati di bilancio.

Si sottraggono i 4.000 euro che vengono dati normalmente ai senatori e si danno al Senato; il Senato paga direttamente i collaboratori di cui esiste un contratto, e naturalmente non paga quelli per cui non esiste un contratto. Si elimina alla radice il rischio virtuale - però purtroppo anche molto realistico

che potrebbe garantire un barlume di serietà del Senato di fronte all'opinione pubblica. Non è la risoluzione dei problemi del bilancio, però è una scelta che permette al Senato di apparire cristallino di fronte alle critiche dell'opinione pubblica. Non capisco il motivo per cui il Collegio dei senatori Questori esprima parere contrario, ma mi rimetto al suo giudizio. Comunque, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha già depositato un disegno di legge che propone esattamente lo stesso concetto.

non si capisce il perché. Forse ci sarà un'occasione futura in cui avremo questo chiarimento. Chiedo la votazione

Signor Presidente, la questione è molto simile sia a quella illustrata poco fa dal senatore Pardi, sia a quella contenuta nell'ordine del giorno G24 dei senatori Ferrara e Fleres,

Anche noi chiedevamo un impegno al Collegio dei senatori Questori a prevedere che ai collaboratori interni dei singoli senatori sia estesa la disciplina del rapporto diretto - a tempo determinato e non incluso nei ruoli - già esistente tra l'Amministrazione del Senato ed i consulenti o segretari dei senatori componenti

Presidente, abbiamo letto con attenzione l'ordine del giorno G8 della senatrice Bonino, sia in ordine a quelle parti che poi

vogliamo procedere in questa direzione, perché è indispensabile, pur nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle persone

formulare un parere, diciamo, convinto, nel senso di saper ben discernere le competenze che assolutamente spettano a noi nel trattamento di questi dati e le competenze che dovrebbero essere valutate a livello legislativo.

per non dare un parere superficiale o senza l'approfondita cognizione di causa che noi vorremmo avere nell'affrontare un tema così rilevante come quello proposto dalla senatrice Bonino.

in realtà, chiede semplicemente di fare proprie mille richieste che abbiamo sentito in questo dibattito, in cui tutta una serie di incomprensioni sono nate anche dalla mancanza di conoscenza di molti nostri colleghi,

e non è successo nessun pandemonio, perché la trasparenza e la conoscenza aiutano ad una lotta che dobbiamo fare per razionalizzare le spese, ma anche per non finire in un turbinio di demagogia che non ci fa bene. Cosa vi chiede ancora? Di fare l'elenco delle proprietà immobiliari del Senato. Lo abbiamo già fatto; me lo avete già dato. Vi si chiede di farlo strutturalmente, perché è un dato importante. Non capisco.

pensano giusto: cari senatori *peones* diversi dalla casta nella casta, questo ordine del giorno chiede - su base volontaria, per carità

senza violare nessuna *privacy* e nessuna legge. Onorevoli colleghi, è vero che viviamo in un momento, come dire, in in cui non sembra che neanche noi riusciamo a fare la differenza tra i costi della politica e i costi della partitocrazia, che fino a prova contraria sono aspetti diversi e che attengono a molti altri settori, dalla legge elettorale ai rimborsi elettorali, però poi

Tant'è che per iscritto già lo dovete fare. Vi prego allora: se c'è una riforma sostenibile che culturalmente ci può far fare un cambio di passo e di rapporto è esattamente quella dell'informazione e della

la lettera di liberatoria; 17 hanno terminato le procedure. Io, che non rincorro i tagli, che non mi faccio veramente l'idea che bisogna mandare tutti in taxi o anche a piedi non credo che solamente la strada dei tagli ci faccia fare un cambiamento davvero di ruolo delle istituzioni, vi chiedo di approvare questo ordine del giorno, che si riferisce a informazione e conoscenza interna a questa Camera e rispetto all'opinione pubblica.

senatori Questori e un gruppo di lavoro, per arrivare a una soluzione meglio studiata e più condivisa tecnicamente e per impedire possibilmente che l'Aula si trovi a votare un ordine del giorno che non sia frutto di uno studio attento tra senatori Questori e proponente, o proponenti.

Presidente, anche adesso, seppur molto brevemente, voglio dare il mio contributo, perché sono molto lieto di aver appreso che alcune consulenze sono state pubblicate sul sito dei radicali.

2,58 milioni di euro per i fabbricati, 3,54 milioni per gli impianti di sicurezza e 625.000 euro per la manutenzione straordinaria degli ascensori

circa 19 milioni di euro - ossia quasi 40 miliardi del vecchio conio -

1,325 milioni per le spese di rappresentanza. Insomma, signor Presidente, non la faccio lunga. Con tutto il rispetto per la meritoria opera dei senatori Questori, è necessaria più trasparenza, maggiore sobrietà e - lo ripeto ancora una volta - anzitutto trasparenza. Tagliando le spese gonfiate e senza cedere alle prediche a gettone ed ai moralismi di facciata, anche da parte dei tanti cattivi maestri che ogni giorno ci vorrebbero dare lezioni,

in cui si chiede che vi sia trasparenza nella gestione delle gare d'appalto per per i lavori e per l'acquisto di beni e servizi del Senato, non fa altro che chiedere l'applicazione dell'articolo 37 del Regolamento interno per il bilancio del Senato. Quindi, non stiamo chiedendo qualcosa di particolarmente trascendentale.

nel mese di giugno abbiamo avanzato la richiesta di ricevere l'elenco delle gare d'appalto che sono state eseguite con importo superiore a 100.000 euro con indicate le procedure ed i soggetti

Lo stesso identico ordine del giorno - poi vi dirò in cosa è leggermente cambiato - è stato approvato

Signor Presidente, sul piano della trasparenza e poi ovviamente della serena comunicazione all'interno dell'attività istituzionale, credo che se questo ordine del giorno viene accettato accettato come raccomandazione si fa un passo indietro rispetto all'anno scorso. Ora, capisco che lei con la sua saggezza mi dirà che è meglio un passo indietro che cadere in avanti...

tratta dell'obbligo per coloro che fanno parte delle commissioni di gara, per la gestione di appalti, di dichiarare se hanno rapporti di parentela con chi vince la gara.

Ho già parlato del problema relativo alla tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti delle società esterne presenti in Senato quando sono intervenuta l'altro ieri in sede di discussione generale

rispettino la legislazione sul lavoro e le norme dei contratti collettivi di categoria. Aggiungo un'ultima novità, cioè la denuncia dell'ultimo ricatto avvenuto ai danni dei dipendenti della ditta Gemeaz Cusin,

a sottoscrivere la seguente rinuncia: «Il sottoscritto (...) dichiara che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro la Gemeaz Cusin sarà autorizzata a trattenere le ferie godute e non maturate alla data di chiusura del rapporto di lavoro». Preciso che questi lavoratori percepiscono miseri compensi e quindi, alla risoluzione del rapporto, si vedranno togliere un ulteriore importo in caso di ferie godute e non maturate. Al danno di non poter usufruire delle ferie nel periodo voluto, a causa della chiusura dei lavori del Senato solo nel mese di agosto, periodo in cui sono costretti a stare in ferie, si unirà la beffa di dover restituire importi per motivi non a loro imputabili.

ai dipendenti che lavorano presso il ristorante del Senato, perché hanno anche loro una dignità. Ritengo che quanto avvenuto non possa che essere condannato da tutti noi. *(Applausi dai

il mio quarto bilancio: sono stati accolti degli ordini del giorno che poi sono rimasti lettera morta, figuriamoci le raccomandazioni!

ma verso un sistema bancario che ogni giorno vessa i risparmiatori, i consumatori e gli utenti. Colgo l'occasione per ringraziare 137 senatori

raccomandazione è essenzialmente legato a un fatto lessicale e semantico del dispositivo. ad esempio, è previsto dalla legge che negli appalti si debba fare un monitoraggio del rispetto della legislazione del lavoro. Non deve farlo il Consiglio di Presidenza o il Collegio dei senatori Questori, ma il soggetto responsabile e titolato dell'appalto. La raccomandazione in quel caso coglieva lo spirito di ciò che l'ordine del giorno prevedeva, ma che non rispondeva però alla lettera.

È bene che lei e tutta l'Aula sappiate che abbiamo intenzione di procedere non a un rinnovo della convenzione, bensì a una procedura di gara che genera una discontinuità.

Lo stavamo accogliendo nella logica dei chiarimenti espressi dai senatori Questori, i quali hanno smentito sostanzialmente l'ipotesi del rinnovo e hanno chiarito che non si andrà al rinnovo, ma si procederà ad una gara.

alla luce del chiarimento ufficiale del Collegio dei senatori Questori, confermato dalla Presidenza, che non è un orientamento ma è una decisione di procedere, alla scadenza della convenzione, a una procedura di assegnazione pubblica, ad una gara, e non ad un rinnovo della convenzione, alla luce di queste di queste affermazioni, lei è pronto a ritirare l'ordine del giorno? Viene meno il presupposto, dal quale lei partiva, del rinnovo della convenzione. Questo, al fine di seguire anche l'osservazione del senatore Lusi ed evitare di commettere involontariamente degli errori. Presidente, sono disponibile a ritirare l'ordine del giorno, alla luce di questi chiarimenti, però non capisco dove sia lo scandalo quando un senatore della Repubblica

Partendo dal presupposto che tutti possiamo sbagliare (*errare humanum est, perseverare diabolicum*), ritengo, alla luce di una rivisitazione più attenta del tema, che sia più coerente la decisione che ho assunto oggi rispetto a quella pregressa, perché nessuno è infallibile. Quindi, sono convinto nel merito di questa inammissibilità, perché per i miei modesti studi giuridici ritengo che, in una fase di diritti quesiti, in relazione alle regole che disciplinano un determinato istituto, non si possa intervenire *ex abrupto* dall'oggi al domani se non con una questione cosa che si sta facendo, tant'è vero che sia la Camera che il Senato sono d'accordo nel disciplinare per la prossima legislatura un regime diverso dei vitalizi rispetto a quello compiuto sinora. Pertanto, si deve applicare la disciplina per moduli temporali e non in pendenza di legislatura. Ma su questo vi è condivisione da parte di tutti. Tra l'altro, nel confermare le inammissibilità nel merito, mi fa piacere anche essere in coerenza con l'altro ramo del Parlamento. Non esiste un'esigenza di duplicazione, ma su questo tema ritengo che il Parlamento abbia quasi il dovere etico, politico, politico, istituzionale di essere coerente nelle scelte, perché lungi da noi l'idea di dare al Paese una rappresentazione delle Camere che la pensano diversamente su temi sensibili. Il tema è importante, è stato dibattuto, e ritengo si siano trovate importantissime convergenze sulla disciplina dei nuovi

Fini, entrare nel merito di queste valutazioni, che naturalmente attengono all'Aula. Dovevo questa risposta, e spero di essere stato esauriente. La presidente Finocchiaro ha presentato un ordine del giorno che

«delibera che: la Conferenza dei Capigruppo delinei rapidamente, d'intesa con la Camera dei deputati, un apposito *iter* per la ridefinizione delle indennità parlamentari secondo quanto previsto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2011». Su questo, non ho nessuna contrarietà, perché è una materia strettamente attinente al bilancio. Le mie perplessità vengono dopo, dove si legge: «nonché che i disegni di legge, già calendarizzati nella 1a Commissione affari costituzionali, riguardanti la riduzione del numero dei parlamentari, le norme sulle incompatibilità del ruolo di parlamentare con l'appartenenza ad altre assemblee elettive e con i corrispondenti incarichi di Governo;

nessuna affinità con il tema che stiamo trattando, così come le norme sulle incompatibilità e la riduzione del numero dei parlamentari. Sono temi che fanno parte dell'agenda politica parlamentare, e potrebbero trovare ingresso nella sede propria di mozioni

Signor Presidente, la ringrazio per questa interlocuzione così motivata. ordine del giorno (chiamiamolo così, anche se probabilmente l'archetipo al quale si ispira non è quello di un tradizionale riprende letteralmente e pedissequamente la prima parte dell'ordine del giorno comune approvato alla Camera dei deputati, con il concorso dei voti dell'opposizione e della maggioranza,

intendo dire che ci muoviamo su una materia che non è controversa nel merito, né potrebbe esserlo, visto che il Senato e la Camera, per la sua parte, sono già impegnati nelle Commissioni sui temi a cui qui si fa riferimento;

sotto il versante delle riforme istituzionali, sia stata considerata come una parte importante della discussione svolta alla Camera, che ora si sta facendo al Senato, in occasione della votazione sul bilancio interno.

unito, da una parte, ad una riaffermazione orgogliosa del parlamentarismo e, dall'altra parte, ad una valutazione del nesso inscindibile tra costo delle istituzioni ed efficacia delle decisioni politiche, parlamentari, legislative;

si sta promuovendo nel nostro sistema rispondono insieme ad un'esigenza di contenimento dei costi che non sono giustificati dalla qualità e tempestività della risposta istituzionale.

hanno una rilevanza costituzionale e vengono considerati dalla Costituzione uno strumento assolutamente importante. Ma di questo ciascuno di noi è convinto, quindi è inutile che insista

Presidente, comprendiamo perfettamente le sue decisioni che, in termini formali e sostanziali, riteniamo dovute, essendo questa una discussione sul bilancio interno del Senato. La parte ammessa

delle indennità parlamentari secondo le medie europee e le valutazioni che più volte abbiamo fatto. Quindi riteniamo che questa parte dell'ordine del giorno sia confacente alle norme esistenti. Personalmente, confrontandomi con la presidente Finocchiaro

tant'è vero che ciò che non può essere contenuto nell'ordine del giorno è già nel calendario della Commissione affari costituzionali. Mi riferisco, per esempio, al tema, delicatissimo, della riduzione dei parlamentari. Non voglio, proprio per il clima costruttivo che si è realizzato in questi giorni, anche nella difficile discussione del bilancio, richiamare precedenti riforme costituzionali e il *referendum* che non ha consentito l'operatività di decisioni già assunte in passato. Quindi, le tralascio, anche perché le abbiamo già richiamate in altre occasioni. Questo, per dire la sincerità di intenti di ciascuno. Poi gli atti parlamentari, le votazioni e le assunzioni di responsabilità

politica. All'inizio della discussione sui costi della politica, abbiamo richiamato tutti i costi degli apparati pubblici e accantonato tutti i discorsi che riguardano i sindacati e altre forme di rappresentanza, per i quali pure dovrebbero attuarsi norme costituzionali che sono rimaste lungamente disattese, riguardanti

Ho chiesto la parola soltanto per ribadire alcune considerazioni, la prima delle quali è che credo che il Presidente del Senato abbia formalmente ragione nell'assumere la decisione che ha assunto rispetto all'ordine del giorno e che la senatrice Finocchiaro abbia politicamente ragione nel porre

e credo possa essere colto uno spunto di percorso nell'ordine del giorno della senatrice Finocchiaro - che in sede di Conferenza dei Capigruppo

il miglior segnale per dire che siamo consapevoli di aver fatto un pezzo di strada, ma abbiamo tutti la comune certezza che il vero costo da superare sono, a volte, l'inefficienza e l'improduttività parlamentari e che il miglior modo per risparmiare è quello di fare finalmente le riforme

faccio mio il suo invito e mi impegno affinché alla ripresa dei lavori si fissi un programma dei lavori della Commissione affari costituzionali che tocchi il tema delle grandi riforme. Alla ripresa ci riuniremo in Conferenza dei Capigruppo e chiederemo alla Commissione affari costituzionali di porre all'ordine del giorno i progetti di riforma che le saranno stati stati trasmessi, anche quello governativo che è stato deliberato due settimane fa in Consiglio dei ministri, per avviare a settembre una fase che chiamiamo costituente del Senato, che è impegnato da tempo a dibattere su disegni di legge di riforma.

delle quali il Senato è stato investito. Dobbiamo fugare ogni eventuale motivo di critica da parte dei cittadini e di chiunque sia, anche di forze politiche, sull'ipotesi che il Senato non intenda lavorare sulle riforme. Abbiamo il dovere di farlo, dobbiamo farlo, lo faremo da settembre in poi.

si è sviluppata attorno all'eterno dibattito tra ciò che si vuole, ciò che deve e ciò che si può fare. Credo che l'esito finale sia un finale sia un risultato che va oltre ogni più ottimistica previsione (specie se si paragona a quanto è stato fatto negli anni passati) dato che i risultati raggiunti sono stati a dir poco eccezionali, visto che da una spesa del 17,34 per cento, come percentuale dell'indennità

Se volessimo fare un paragone con quello che succede nelle società per azioni, avrebbe avuto il significato di una Assemblea i cui pacchetti di maggioranza sfiduciavano al momento dell'approvazione del bilancio il proprio consiglio di amministrazione. Probabilmente così non è e così non è stato, tanto che poi siamo arrivati ad un ordine del giorno, firmato pure dal presidente Viespoli e da me condiviso, che ha voluto indirizzare, non già correggere ed emendare, l'opera del Consiglio di Presidenza e dei senatori Questori verso cose migliori che debbano essere fatte

il Presidente del Senato, che rappresenta la seconda carica dello Stato, e tutte le persone che si sono impegnate affinché il voto su questo bilancio fosse il più ampio e condiviso possibile. Credo che discutendo del bilancio servano due premesse fondamentali. Una è di carattere economico, ed era già stata richiamata

di consumi intermedi, tra cui ci sono 30 o 40 miliardi che corrispondono ai costi della politica. Allora, credo che oggi, approvando il bilancio del Senato, noi dobbiamo assumerci un impegno molto preciso anche molto urgente nell'intervenire sui costi della politica. Serve anche un'altra premessa: noi siamo eletti dal popolo italiano e rappresentiamo il Senato della Repubblica. Credo che lo dobbiamo fare con autorevolezza, perché dobbiamo difendere questa istituzione: non può essere denigrata e calpestata ogni giorno dalla stampa. I cittadini non si riconoscono più in noi e credo che anche, ma non solo, le scelte che vengono fatte con il bilancio noi dobbiamo dare dei segnali affinché si cerchi di recuperare questo iato. Un'altra considerazione, che in buona parte è accolta nell'ordine del giorno condiviso quasi da tutti i Gruppi, è che questo bilancio, così com'era arrivato in Aula inizialmente, non era sufficientemente chiaro chiaro e comprensibile ai più. In alcuni interventi in discussione generale questo elemento era stato posto, e prontamente e correttamente si è cercato di intervenire proprio sugli aspetti della trasparenza, ma anche della della ridefinizione di alcune voci di bilancio. Credo che anche questo sia un segnale positivo che noi diamo. Entrando nel merito specifico del bilancio, voglio riferirmi a tre aspetti che hanno caratterizzato il nostro Gruppo politico Per il Terzo Polo: ApI-FLI. Noi abbiamo cercato di incidere su tre

i nostri vitalizi e il costo del personale, che è l'altra grande voce. Parlando dei dipendenti, mi sento - ci sentiamo - di esprimere innanzitutto un atteggiamento di gratitudine di gratitudine per il lavoro che svolgono sempre al servizio del popolo italiano: lavorano infatti in un'istituzione che è al servizio del popolo.

e ai funzionari del Senato cercheremo di costruire una risposta adeguata, proprio a partire dai nostri compensi e dai nostri vitalizi. Conosco benissimo la distinzione tra vitalizio e pensione; credo però occorra un atto di responsabilità La seconda voce che abbiamo individuato è quella relativa ai contributi che vengono elargiti ai Gruppi per il loro funzionamento e ai partiti attraverso i rimborsi elettorali.

la vita politica e anche l'attività dei Gruppi costa; sappiamo benissimo che costa, ma in un momento in cui il Paese si trova in una situazione di estrema gravità economica e finanziaria (non è casuale che questo pomeriggio il Presidente del Consiglio venga qui per questo)

il contratto; non compete a me e quindi invito poi la dirigenza e i senatori Questori ad assumersi tale responsabilità.

con le nostre parole e azioni affermare l'autorevolezza del luogo in cui ci troviamo. A tal fine auspichiamo che tutti gli obiettivi contenuti in modo preciso e completo nell'ordine del giorno che noi stessi abbiamo approvato siano resi effettivi a partire dal prossimo anno. In fondo, l'intervento e la presa di posizione del collega, senatore Baldassarri, che ringrazio, andava proprio in questa direzione, non era di contrarietà in sé ai

eletti, rappresentativo della crisi profonda di tutte le democrazie occidentali. Sappiamo che non è solo e non è tanto riscrivendo il bilancio del Senato che si riuscirà a colmare questa dicotomia: siamo certi che occorrano scelte che possano contribuire a riscrivere un patto di fiducia e di fraternità tra cittadini ed eletti. In conclusione, riteniamo che dobbiamo continuare il percorso che abbiamo intrapreso speriamo di poterlo fare insieme. Il Gruppo per il Terzo Polo (ApI-FLI) voterà a favore sia del rendiconto che del bilancio di previsione

unanime. Termino con le parole di Aldo Moro, che ha detto che si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con le sue difficoltà. In questo momento stiamo vivendo un momento di terribile difficoltà A noi è chiesto di vivere questo tempo e di fare scelte di responsabilità, a partire anche dal bilancio che oggi approviamo. Dobbiamo assumerci probabilmente una responsabilità maggiore.

esprimerà voto contrario sulla tardiva e anche - lasciatemelo dire - un po' rattoppata e rappezzata proposta di bilancio interno che ci è stata presentata.

Tutti hanno detto, e stanno dicendo, di essere d'accordo che tagliare i rami secchi, gli sprechi e le inefficienze rappresenta non solo una necessità evidente a tutti, ma un dovere, cui nessuno in questo momento può sottrarsi. E questo, non solo per le esigenze di riduzione della spesa pubblica, ma soprattutto per far recuperare un minimo senso di credibilità alla nostra politica, al nostro ruolo e alle nostre funzioni. Il punto è che nessuno vuole tagliare per primo il ramo su cui è seduto. Avremmo anche noi potuto stupirvi con l'esposizione di tabelle di comparazione con i costi ed i trattamenti degli altri Parlamenti europei, ma in queste tabelline - che forse, per qualche istante, sono riuscite a tranquillizzare la coscienza di qualcuno - è sfuggito di inserire un particolare non affatto marginale: manca la cifra etica. È questa la cifra che dà credibilità alle istituzioni, perché in nessun Parlamento europeo (francese, tedesco o inglese) è consentito al proprio interno o all'interno dei Governi che essi sostengono che vi siano rappresentanti del popolo indagati, imputati o - peggio - condannati. Durante la discussione è stato fatto il paragone con il Parlamento tedesco, con quello Karl-Theodor zu Guttenberg ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da Ministro della difesa tedesco, perché era stato accusato di aver copiato parti della sua tesi di dottorato; il deputato democratico di New York Anthony Weiner ha deciso di lasciare l'incarico dopo essere stato coinvolto in uno scandalo a luci rosse; Georges Tron, segretario di Stato francese alla funzione pubblica, si è dimesso perché accusato di aggressione. Immaginate soltanto per un attimo cosa sarebbe del nostro Parlamento, se applicassimo questa cifra etica. È forse allora - e soltanto allora capirete perché il popolo italiano non si è mai sognato di porsi il problema di chiedere l'entità degli emolumenti di uomini come Enrico Berlinguer, Giorgio Almirante o Aldo Moro. La cifra etica, però, si misura anche dall'utilità che le istituzioni producono per il proprio Paese, perché purtroppo i comportamenti (meno recenti, ma anche recentissimi) di questa maggioranza del Parlamento hanno diciamo la verità fino in fondo - prima il sospetto, ora l'indignazione per il fatto che l'attività delle Aule parlamenti abbia la principale preoccupazione, anzi, l'unico scopo, di salvare il Capo del Governo dai suoi guai giudiziari e la stessa maggioranza

Riteniamo semplicemente che questa sia un'altra occasione persa da parte di una politica irresponsabile, che sta facendo di tutto per far perdere credibilità alle istituzioni per mancanza di un buon esempio. senatori Questori, so che non dipende tutto dal vostro lavoro e dal vostro impegno, ma ben altri erano i segnali di cui l'Italia aveva e ha bisogno, a partire dalle istituzioni centrali, per scendere poi agli uffici periferici degli enti locali, del parastato e del sottogoverno. Non marginali riduzioni di sprechi e inefficienze, ma decisioni forti e ispirate al rigore: sarebbe stato necessario il segnale che la politica si riappropriasse dello spessore morale di una classe dirigente degna di questo nome, che, di fronte alle gravi difficoltà del suo Paese, reagisce con misure vere, concrete e immediate, tali da esercitare una guida morale per il Paese. Avremmo potuto dire anche noi

di fronte agli ordini di grandezza di una spesa pubblica e di un debito pubblico che continuano ad autoalimentarsi, perché sappiamo tutti molto bene che il vero risparmio arriverebbe soltanto dalla drastica riduzione dell'apparato amministrativo dello Stato e da molti altri tagli, più volte promessi e mai applicati: abolizione delle Province, snellimento delle Regioni, eliminazione del sottobosco di società parassite ed enti inutili. Ma resta il fatto che mentre il Paese sta con il fiato sospeso perché i picchi del differenziale del tasso di interesse dei nostri titoli di Stato stanno vanificando e bruciando i sacrifici fatti e quelli nuovi richiesti, mentre la manovra economica varata poche settimane fa da questo Governo comincia a pesare in modo concreto nelle tasche degli italiani, le persone normali, le persone normali, i lavoratori, i pensionati, i precari, quelli che non appartengono a nessuna categoria protetta, cominciano a pretendere che i sacrifici vengano ripartiti in modo equo. Chiedono che la stagione di austerità richiesta agli altri tocchi ancor prima i privilegi di chi siede in Parlamento, di chi siede nei Consigli regionali e nelle Giunte delle 110 Province italiane. Qualcuno dirà che è una presunzione inaudita. Noi diciamo che è una reazione giusta e scontata. Avremmo potuto benissimo dire che in un Paese come il nostro, dove esistono 8 milioni di poveri, di cui 3 davvero nell'indigenza assoluta, che annovera con sempre più frequenza nuovi poveri le famiglie numerose (come a dire che la nascita di un figlio in Italia è diventata un fattore di povertà), non fa un buon servizio la doppiezza e l'ipocrisia di una certa politica. Non serve dire «tagliamo», Non serve dire «tagliamo», se poi si sposta il momento alle calende greche o se si usano artifici contabili per cancellare voci insignificanti e farne entrare altre per compensazione. Alla vigilia della presentazione della manovra economica di luglio il ministro Tremonti annunciò: «Sui costi della politica l'intervento del Governo ha disegnato un radicale e rivoluzionario cambiamento». Si riferiva ai 6 articoli del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, di cui il primo è un vero capolavoro di ipocrisia: l'istituzione di una mega commissione presieduta dal Presidente dell'ISTAT con quattro esperti di chiara fama per capire come riformare i trattamenti economici dei parlamentari, purché avvenga a partire dalla prossima legislatura. il primo a non credere a questi risparmi è stato proprio Tremonti, tant'è che all'articolo 5 dello stesso decreto-legge convoglia tutti i futuribili risparmi non al Fondo di ammortamento dei

è difficile che qualcuno si accorga veramente dei risparmi che sono stati prodotti. A queste parole poi si sono aggiunte quelle del ministro Calderoli che, anche lui, ha annunciato una sua risposta vera, concreta e immediata alla questione del costo della macchina pubblica. E cosa ha proposto? Una riforma costituzionale che ancora una volta, per i tempi che richiede, rinvia tutto alla prossima legislatura. Il peggiore errore in cui state cadendo e il grave problema in cui ci state trascinando e di cui fate finta di non rendervi conto è che questo Parlamento sta delegittimando se stesso. Non riuscite a capire che la nostra democrazia da tempo non si regge più soltanto sulla gamba delle istituzioni rappresentative la società chiede che per la gestione della cosa pubblica vi sia sobrietà, rigore morale e l'abolizione, ora e non domani, di sprechi e privilegi. e non quelli del Paese rischia di isolarci ancora di più dall'opinione pubblica, innescando meccanismi - questi sì pericolosi, non le scontate campagne di di stampa - di delegittimazione delle nostre istituzioni che questo Paese, ora più che mai, non può permettersi.

io rivolgo ai colleghi senatori): «Egregio direttore, come si può vivere in un Paese dove gli scandali investono tutti gli schieramenti politici? Dove furbi, affaristi, intrallazzatori, truffatori, ruffiani, faccendieri sono "agganciati" a partiti e politici? Dove si mettono i *ticket* sulla sanità senza ridurre l'enorme spesa della politica e degli enti inutili? Dove stipendi e pensioni non sono rapportati al caro costo della vita? Dove i giovani rischiano di rimanere senza un lavoro o precari a vita?». Questa è la domanda che un cittadino normale ha rivolto all'opinione pubblica. Onorevoli colleghi, noi dell'Italia dei Valori riteniamo che questa sia stata un'altra occasione persa per tentare di iniziare a dare una risposta a tale domanda

Signor Presidente, colleghi senatori Questori, colleghi, il bilancio è di per sé l'atto politico fondamentale di ogni Amministrazione, nel quale, tramite le cifre, sono delineati obiettivi e finalità, così come emergono anche nelle relazioni di accompagnamento. D'altra parte, esso va D'altra parte esso va approvato o meno proprio sulla verifica della congruità e dell'efficacia, rispetto agli obiettivi e alle finalità da raggiungere, per cui, proprio nella fase in cui viene discusso e prima di essere deliberato, è possibile apportare modifiche più o meno sostanziali senza stravolgerlo, pena le dimissioni di chi lo ha redatto per sfiducia conclamata.

da quella approvazione sono poi intervenute, a seguito e conseguentemente alle già approvate disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria previste dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011. Il mio Gruppo intende dare atto ai senatori Questori di aver tentato di coniugare l'efficacia del funzionamento della macchina amministrativa con la necessità di moralizzare e tagliare la spesa, tenendo nella dovuta considerazione l'eccezionalità della situazione economica del Paese, che ha chiesto gravi sacrifici ai cittadini, nonché l'esigenza del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dall'Europa. Compito peraltro assai difficile, tenendo conto che siamo già al consumo dei sette dodicesimi della spesa e che si tratta di un bilancio in cui le spese fisse per stipendi del personale sono la voce preponderante. D'altra parte, se è vero che non si può e non si deve legiferare sotto la pressione di una opinione pubblica scatenata dall'antipolitica, non solo contro i parlamentari, signor Presidente, ma contro le stesse istituzioni, è pur vero che bisogna dare subito delle risposte chiare e responsabili alla sete di giustizia che la protesta sociale esprime ancorché fomentata in modo sconsiderato contro tutto e senza distinzioni, con grave pericolo, così come più volte sottolineato dal Capo dello Stato, per la tenuta democratica del Paese e per le istituzioni che lo governano.

Credo che non si debbano ascoltare soltanto gli esponenti dei Gruppi maggiori, perché spesso il vino buono sta nelle botti piccole, come si dice dalle nostre parti, e i partiti piccoli spesso sono stati il sale della democrazia; e anche in questo sessione di bilancio hanno contribuito ad

Credo di poter dire che l'intervento dei senatori Questori, e il successivo confronto di questi con i rappresentanti di tutti i Gruppi politici presenti in Senato, abbia saggiamente evitato la suggestione di interventi interni ed esterni che potevano condizionare le decisioni assunte, codificate invece in un ordine del giorno largamente condiviso, per il quale voglio esprimere un ringraziamento, oltre che ai Questori, ai membri del Consiglio di Presidenza e al senatore Azzollini, che si è prodigato con equilibrio a raccogliere le indicazioni più valide espresse dai vari Gruppi. L'ordine del giorno traccia la strada per una riforma complessiva del bilancio, aspetto non sufficientemente sottolineato, ed obbliga a predisporre un documento finanziario di accompagnamento nelle more della riforma del regolamento volta a prevedere un bilancio pluriennale che, entro l'orizzonte temporale di una legislatura, contenga anche una programmazione funzionale delle spese e degli interventi da effettuare, corredata da modifiche espositive e comunicative che consentano una maggiore leggibilità e trasparenza.

la decisione di proseguire nel processo di razionalizzazione e progressiva riduzione effettiva della spesa, mediante la sua costante revisione e avendo come punto di riferimento non il criterio della spesa storica, ma quello della base zero, anche d'intesa con la Camera dei deputati. La decisione di mantenere invariata nel triennio la dotazione ordinaria (che peraltro rappresenta l'entrata principale del Senato) assicura un consistente risparmio al bilancio dello Stato, mentre la previsione di una riduzione della spesa relativa all'esercizio 2011 fino a concorrenza dell'1 per cento (introdotta grazie alla citata riunione) impegna ad apportare ai documenti di bilancio per lo stesso esercizio le conseguenti modifiche.

Ed ha avuto un'ampia assicurazione, anche da lei, Presidente, che è intervenuto nella fase finale della nostra discussione, che tagli lineari non saranno fatti. Di questo siamo soddisfatti. I nostri suggerimenti sono stati quasi tutti accolti, a dimostrazione che è necessario tenere il dibattito sempre aperto tra tutti i Gruppi politici e non soltanto tra i due Gruppi maggioritari. Saremmo stati ancor più soddisfatti, però, se si fosse accolta la nostra proposta di aprire un confronto anche sulla previdenza dei dipendenti, sul finanziamento dei Gruppi politici e non solo sui vitalizi. Tale tema va affrontato con riguardo al ruolo e alle funzioni che i parlamentari svolgono, non in chiave demagogica, e con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale.

che il vitalizio non sia una delle prerogative che spettano a deputati e senatori che cessano dal loro mandato, non avete da fare altro che ri-nun-ciar-vi.

ha messo a fuoco più l'esigenza politica dell'efficacia mediatica delle proposte avanzate (che ho considerato per lo più, salvo alcune, molto estemporanee), che non l'esigenza di contribuire nel merito a migliorare l'efficacia funzionale del bilancio del Senato. Quando si parla di bilancio, ci si riferisce ad un atto che è tecnico e politico, sul quale bisogna intervenire perché ci sia effettivamente un'efficacia funzionale delle poste che mettiamo a bilancio, che sono indirizzate a finalità e ad obiettivi che devono essere perseguiti nell'arco temporale in cui il bilancio è vigente. Di questo stiamo parlando, non di tutte le altre questioni che possono anche entrare a corredo, ma non sono la sostanza del bilancio; questa è la verità. l'esigenza di migliorare l'efficacia funzionale non è stata sufficientemente sottolineata. La spesa del Senato, infatti, negli ultimi anni è divenuta incompatibile con lo stato della finanza pubblica e con le esigenze di trasparenza e vi abbiamo posto rimedio con l'ordine del giorno che abbiamo sottoscritto tutti quanti o quasi tutti. Poiché noi utilizziamo risorse pubbliche, è necessario anche che rendiamo conto del loro utilizzo ai cittadini ed è una cosa giusta. Credo pure che saranno necessarie le nuove direttive che abbiamo abbozzato, concernenti una diversa metodologia contabile di gestione della spesa e anche, signor Presidente, del controllo, a mio parere non sufficientemente sottolineato, nonché nuove norme tecniche regolamentate per l'amministrazione e la contabilità a tutela dell'istituzione del Senato, della sua e della nostra onorabilità, che è ora, Presidente, di difendere, senza timore e con coraggio, accettando la sfida,

a meno che non ci sono fatti da denunciare, «nessuno più di me e nessuno meno di me». Siccome io ritengo di essere una persona corretta, che qua dentro fa il suo lavoro come l'ha sempre fatto, penso che anche i miei colleghi siano persone altrettanto corrette, che fanno il loro lavoro e lo hanno sempre fatto, a meno che qualcuno voglia dimostrare il contrario, senatore Questore Cicolani)*, senza dire sempre che qui dentro succede questo e quello e senza mai imputare a chi di dovere le cose che si dicono. È troppo facile, Presidente, è qualunquismo da strapazzo che non fa altro che negare il decoro della nostra istituzione, dando fiato alle trombe esterne per dire ciò che dicono, su cui, Presidente, le chiedo effettivamente, anche a nome del mio Gruppo, di spendere la sua autorevole parola perché questo linciaggio sistematico e generalizzato deve finire! deve finire! Quando si parla di privilegi, dobbiamo precisare che alcuni lo sono e noi abbiamo l'intenzione doverosa e corretta di porvi fine, ma altri sono prerogative e la prerogativa è legata alla funzione istituzionale che noi esercitiamo. Allora, o la funzione ha un alto valore istituzionale, perché è al servizio

con una rinnovata responsabilità, senza voler poi dire che in passato le cose erano fatte senza riflessione e senza correttezza. Lavoriamo nel senso di una giusta razionalizzazione, che tiene conto ovviamente delle richieste che ci vengono dai cittadini e siamo in sintonia con i cittadini che qui rappresentiamo. Non ci dimentichiamo mai che il popolo è sovrano, come recita la nostra Costituzione. Bene ha spiegato il collega Morando in precedenza che le riduzioni, le economie che prevediamo con questo bilancio questo un giusto esempio - sono assolutamente maggiori di quelle riduzioni ed economie che abbiamo chiesto al Paese nell'ultima manovra finanziaria che abbiamo approvato. Abbiamo sentito parlare di un taglio su questo bilancio di 120 milioni, al quale proprio in seduta odierna abbiamo applicato un'ulteriore riduzione di 6 milioni. Più che di tagli, vorrei parlare di economie,

Non capiamo le contestazioni che ha fatto l'Italia dei Valori su quest'ultima riduzione di 6 milioni:

è un partito molto anomalo, per certi versi. Ricordo ancora un vostro parlamentare che, intervenendo in sede di bilancio, ha detto che con l'indennità

con il costo che ha la nostra attività e quindi valutando se l'investimento raffrontato ai risultati è accettabile o meno: questo dobbiamo chiedercelo, ovviamente, ogni giorno e non soltanto quando esaminiamo il nostro bilancio.

inoltre tagliare tutti i vincoli alla libertà d'impresa, perché a questo sono attualmente legati tutti i costi che ci sono nel non fare. Il Paese è bloccato e non fa, e il non fare ha

ce ne facciamo comunque carico nel senso che, qui eletti, ci assumiamo la responsabilità di riformare anche questo aspetto del nostro Paese. Anche questo è legato a una riforma federale

oggi approveremo il bilancio consuntivo e preventivo del Senato. Oggi pomeriggio il Presidente del Consiglio sarà in Aula nel tentativo estremo di dare risposte adeguate ad una crisi che ci sta travolgendo: una crisi inedita, senza precedenti, che mescola le economie dei Paesi, la finanza, le speculazioni finanziarie, in un gioco delle tre carte difficile da comprendere. C'è un legame fra questi due atti? C'è, eccome. Fra le cause della crisi del nostro Paese, c'è un debito fra i più alti del mondo, che va ridotto, tagliato, e per ridurlo bisogna che il Paese torni a crescere. Quante volte lo abbiamo detto nei dibattiti in quest'Aula e invece voi non siete stati capaci di farlo. Bisogna fare tagli alla spesa e sacrifici senza precedenti per le imprese, le famiglie, i cittadini: tutti devono e dovranno fare sacrifici. Il Paese oggi è più povero e lo sarà ancora di più. Ma per chiedere sacrifici inediti, serve una classe politica credibile, seria e responsabile. Non si possono chiedere sacrifici al Paese se non si è disposti a farli. Ecco il legame fra i due avvenimenti di questa giornata, fra le decisioni che dobbiamo prendere. Il bilancio che stiamo per approvare risponde a questa esigenza? Si poteva fare anche di più, ma quella che approviamo con l'ordine del giorno della maggioranza e del Partito Democratico è una risposta adeguata, seria e responsabile.

ma in questo momento serviva qualcosa di più ed era compito del Parlamento dare un *input*, un indirizzo, degli obiettivi precisi. Noi non ci siamo sottratti all'impegno. Una volta tanto ci avete ascoltato, ci siamo parlati e abbiamo trovato una convergenza significativa e importante. è la buona politica, un po' di buona politica, un esempio per il Paese, quello che ci chiedono i nostri cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ecco che cosa non avete fatto sulla crisi: ascoltarci, parlare. E avete fatto male, molto male, purtroppo per il Paese.

alla ristorazione, dalla presenza in Parlamento ai viaggi, al personale, agli appalti e alle auto blu, fino ad arrivare ai Presidenti e ai benefici che avevano gli ex Presidenti. Tagliare in questa misura e con questa importanza significa ridiscutere seriamente molte cose, ma assieme - come abbiamo dimostrato con l'approvazione di questo ordine del giorno e come dimostreremo con l'approvazione del bilancio - possiamo farlo. farlo. È un messaggio forte, quello che viene dalla decisione che stiamo prendendo. Oggi, dopo questa decisione, noi e voi saremo più credibili di fronte al Paese, perché ci mettiamo la nostra faccia, invece voi non avete fatto sulla crisi, dicendo prima che non c'era e poi rinviando ogni decisione al 2014. E avete fatto male anche in questo caso. Guardate che se il capofamiglia se il capofamiglia non ci mette mai la faccia, la famiglia prima o poi lo sfiducia, e fa bene. Adesso nel nostro Paese siamo in questa situazione. Ma torniamo a noi, al nostro bilancio.

perché è giusto nel merito e perché ci rende un po' più credibili agli occhi dei nostri cittadini. In quattro anni, fare tagli per 160‑170 milioni, in un bilancio che non è neanche di 600 milioni, è una prova di grande coraggio e responsabilità civile, e vigileremo perché ciò venga fatto, punto per punto. Oggi c'è un pesante attacco alla politica, ai partiti, alle istituzioni democratiche. Noi siamo i rappresentanti della sovranità popolare: sta a noi fare di tutto per respingere un attacco che, attraverso noi, attenta al principio della rappresentanza, della sovranità popolare e della democrazia. Se viene snaturata e irrisa la rappresentanza politica, cioè noi, il Parlamento, viene snaturata e irrisa la democrazia. E una democrazia irrisa dai suoi cittadini non è più una democrazia. Ricordiamolo a noi stessi, ma ricordiamolo sempre ai nostri cittadini. Oggi noi prendiamo una decisione che ci fa sentire più vicini ai nostri cittadini e ci fa girare un po' di più a testa alta tra di loro. Ogni tanto la buona politica vince. Speriamo che la nostra decisione, l'ascoltarci, il dialogare, questo esempio di oggi - questo piccolo esempio di oggi, se vogliamo, perché il nostro bilancio rappresenta una piccola percentuale del bilancio dello Stato - sia un utile esempio per come affrontare un problema più serio è più complesso come la crisi che attraversa il Paese, che ha bisogno di scelte coraggiose e di una classe politica coraggiosa e credibile, cosa che voi, purtroppo, non avete dimostrato di essere.

Non è un fatto episodico, perché in tutti i bilanci approvati in questa legislatura non abbiamo mai aumentato la spesa in termini nominali. Questo vuol dire che già prima di questo bilancio avevamo ridotto le spese in termini reali tra il 4 e il 5 per cento. In passato non era accaduto neppure una volta. Oggi accade per il terzo anno consecutivo, e con l'ordine del giorno approvato prendiamo il medesimo impegno per i prossimi anni. Quindi, vorrei evitare che su questo punto ci fosse l'atteggiamento che tutti sono pronti a

reali. Non si può imputare al Senato di aver ridotto meno di quanto magari si sia ridotto altrove, quando noi già dall'inizio di questa legislatura, indipendentemente dal fatto di aver diagnosticato o meno la crisi economica, abbiamo attuato una politica che

legislatura nel modo in cui bisognava farlo, cioè riducendo il deficit e, di conseguenza, ponendo un freno alla crescita del debito pubblico, mentre altri, che poi dicono di aver fatto le diagnosi giuste, ci dicevano di aumentare la spesa,

appunto, da una politica che qui ci veniva suggerita da coloro che oggi ci dicono che loro l'avevano detto prima. Ma torniamo, come credo sia più normale, al bilancio del Senato.

Del resto è la continuazione di una politica che va avanti da tempo. Ricordiamo - vale la pena di dirlo ancora - che le indennità dei parlamentari sono state ridotte del 10 per cento

termini nominali, dal 2001 e che sono state ulteriormente ridotte di 1.000 euro al mese in termini netti all'inizio di quest'anno. Ricordiamo, per quanto sia possibile, all'esterno, all'esterno, che il Parlamento ha agito in particolare sui compensi ai parlamentari. Spiace qui non avere nessuno presente della stampa, alla quale pure riserviamo un'ottima tribuna: potremmo fare magari un comunicato sull'assenteismo dei signori giornalisti. La loro assenza potrebbe persino non essere così sgradita se si accompagnasse a un'informazione, che indubbiamente si può avere anche al di fuori di quest'Aula; in altre parole, io credo che da oggi dobbiamo impegnarci tutti quanti a contrastare le menzogne che continuano ad essere diffuse tutti i giorni sui giornali, di tutte le parti politiche, ivi inclusi quelli cosiddetti indipendenti,

Credo che questo sia opportuno ribadirlo. Oggi noi votiamo un documento importante. I 56 centesimi al mese che costa ad ogni cittadino il Senato devono essere amministrati come se fossero 56.000 euro. Sono cifre comunque importanti e dobbiamo amministrarle nel modo migliore, e quello che approviamo oggi è un esempio di amministrare bene, un esempio che non si deve fermare qui. Io credo che la stessa energia, la stessa produttività, lo stesso impegno che abbiamo messo nel ridurre fino ad oggi, e nel prossimo nel prossimo futuro, le spese del Senato dobbiamo anche metterli per colpire determinati eccessi, determinati reali privilegi di persone il cui *status* sta molto al di sopra, dal punto di vista del trattamento economico, dei parlamentari, di istituzioni la cui produttività è anche

pesino di meno sulla vita quotidiana dei cittadini e sulle loro tasse. Colleghi, prima di procedere alla votazione al termine dell'esame di questo bilancio desidero ringraziare i senatori Questori e il presidente Azzollini per l'attenzione e la competenza con le quali hanno affrontato questioni delicate e rilevanti per il contenimento dei costi e delle spese. Lo sforzo del Senato è un segno importante di come anche le istituzioni rappresentative rispondano alle esigenze dell'intero sistema Paese.

In altri termini, tutti i tagli sono effettivi e non sugli andamenti tendenziali. Si è fatta quindi una scelta coraggiosa, trasparente e di assoluto rigore. Questi risultati non hanno precedenti e rappresentano un punto di arrivo che nasce dal contributo e dal confronto di tutti i Gruppi. Sono decisioni serie e straordinarie, come ha chiarito con precisione poc'anzi il senatore Morando. Questo dimostra che è possibile lavorare insieme per il bene del Paese e si possono, si devono affrontare insieme le scelte necessarie, anche se dure ed impegnative. Ringrazio infine, consentitemelo, l'Amministrazione, che ha saputo rispondere alle esigenze del contenimento della spesa pubblica con vero senso di responsabilità: è meritevole del nostro convinto apprezzamento. La maggioranza assoluta dei sindacati ha infatti accettato di bloccare gli adeguamenti stipendiali del 3,2 per cento, non recependo misure di favore che sono state invece concesse ai dipendenti di altre Amministrazioni, come ha ricordato stamattina il senatore Questore Adragna. Al segretario generale, dottoressa Serafin, e per suo tramite a tutti i dipendenti del Senato, assunti con concorsi particolarmente difficili, rigorosi e la cui alta professionalità è da tutti noi riconosciuta, va dunque il nostro pieno e totale apprezzamento. Credo che il lavoro che abbiamo realizzato dimostri che è possibile, e a volte è doveroso, coniugare eccellenza, merito e responsabilità. Le istituzioni - ricordiamolo - sono un patrimonio di tutti, che va difeso. Ed oggi credo che lo abbiamo fatto con serietà e coerenza, e io posso sentirmi e mi sento orgoglioso di presiedere questa assise, in particolar modo in una giornata come questa. Vi comunico che sto per trasmettere al ministro Tremonti la lettera con cui formalizzo la rinunzia a 24 milioni di euro, grazie al bilancio che sta per essere approvato tra qualche attimo. Mi sembrava doveroso informare Prima della votazione finale, vorrei informarvi che, per quanto riguarda il prosieguo dei lavori, la seduta riprenderà alle ore 15,30 con l'informativa del Sottosegretario per gli affari esteri. Seguirà la discussione del disegno di legge sul Fondo monetario internazionale e delle ratifiche di Accordi internazionali. Come già comunicato ai Gruppi, l'informativa del Presidente del Consiglio, in relazione al differimento alle ore 17,30 del previo intervento presso la Camera dei deputati, avrà luogo al Senato alle ore 19,30, sempre con trasmissione diretta televisiva. Avverto infine, previa intesa intercorsa tra i Capigruppo, che la riapertura dell'Assemblea dopo la pausa estiva sarà anticipata alla giornata di mercoledì 7 settembre per lo svolgimento di argomenti di sindacato ispettivo.

su cui si sta concentrando l'attenzione della comunità internazionale per la brutalità delle inaccettabili violenze condotte contro la popolazione civile. Come sapete, il Governo ha preso ieri una decisione importante: il ministro Frattini ha richiamato a Roma, per consultazioni, il nostro ambasciatore a Damasco Achille Amerio, per dare un forte segnale politico di riprovazione nei confronti dell'orribile repressione posta in essere dal regime siriano, auspicando che anche gli altri Paesi dell'Unione europea adottino la stessa misura. Abbiamo scelto per primi di richiamare il nostro ambasciatore, perché per l'Italia, che è in prima linea a livello internazionale per promuovere i diritti umani, questi vili attacchi contro i civili sono assolutamente intollerabili. Il Governo ha ritenuto inoltre fondamentale promuovere un'azione da parte delle Nazioni Unite. Il nostro Ministro degli affari esteri ha chiesto e ottenuto che venisse convocata una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza per esaminare la crisi siriana. Il Consiglio di Sicurezza si è quindi riunito in tre sessioni, l'ultima nel corso di questa notte. Al momento, non sono ancora state adottate decisioni. Come sapete, vi sono infatti due linee di pensiero in seno al Consiglio sul formato della presa di posizione da adottare. Come sottolineato dal ministro Frattini, il Governo ritiene che si debba arrivare ad una risoluzione delle Nazioni Unite che imponga ad Assad di terminare la repressione. La comunità internazionale deve infatti dimostrarsi compatta nel deplorare questa inaccettabile situazione, che è suscettibile di avere impatti negativi sull'intera regione. La violenta e massiccia repressione attuata quest'ultimo fine settimana - e anche in queste ore - ha in effetti fatto segnare un peggioramento della crisi siriana, che si protrae ormai da fine marzo, quando sono iniziate le manifestazioni popolari volte a condannare la corruzione e a richiedere riforme democratiche nel Paese. Dal mese di marzo sono stati uccisi oltre 1.600 civili, con 12.000 arresti e 3.000 persone scomparse; sono inoltre presenti 10.000 profughi in campi di accoglienza turchi e circa 3.000 in Libano. Alla strategia muscolare applicata dal regime di Assad per spegnere le rivolte, in particolare nella cittadina di Daraa, nel sud del Paese, hanno fatto seguito proteste sempre più diffuse e una repressione sempre più dura, con una spirale di violenza che si è allargata via via a Lattakia, Douma, Homs e diverse altre località del Paese. Con il proseguire delle rivolte, le autorità siriane hanno deciso di seguire la strada della repressione militare, che ha assunto una dimensione sempre più ampia fino ad arrivare al massiccio intervento contro la città di Jisr al-Shagour fra il 4 ed il 6 giugno scorsi, che ha provocato un rilevante esodo di rifugiati siriani verso il confine turco, stimato in circa 10.000 individui, oltre ad un considerevole numero di profughi provenienti da tutte le zone rurali del Paese. Assad si è dimostrato incapace di gestire efficacemente l'ondata di protesta, promettendo riforme senza darvi seguiti concreti, ma limitandosi ad enunciazioni declaratorie e propagandistiche. Egli ha pronunciato tre discorsi, tutti e tre ben al di sotto delle aspettative. Ha adottato misure di parziale liberalizzazione dei partiti politici, ma senza intaccare sostanzialmente il monopolio del Partito ha abolito la legge sullo stato di emergenza, senza incidere sull'atteggiamento dell'apparato di sicurezza siriano; ha messo in cantiere una legge sui *media* da cui, per il momento, non è scaturita nessuna apertura. Anche il dialogo con l'opposizione da lui avviato è rimasto in buona parte sterile, in assenza di un coinvolgimento dei segmenti portanti del movimento di protesta e di un meccanismo credibile per convogliare i risultati dell'esercizio nel processo decisionale. La Conferenza degli intellettuali, autorizzata da Assad e svoltasi il 27 giugno sotto l'occhio attento del Governo, è stata boicottata dalla maggior parte degli oppositori, mentre l'esercizio di «Dialogo Nazionale» organizzato dal regime il 10 e il 12 luglio scorso è stato largamente fallimentare, perché privo delle opposizioni. I movimenti di opposizione, tuttavia, continuano ad essere estremamente parcellizzati e poco organizzati, mentre i due principali centri urbani del Paese, Damasco e soprattutto Aleppo, restano estranei alle proteste.

Preoccupa, inoltre, il rischio di un riemergere delle tensioni settarie fra comunità etniche e religiose, che potrebbero indebolire il fronte della rivolta, ampliando le divisioni, e fomentare ulteriori violenze ed instabilità. La crisi, resa sempre più complessa dai recentissimi eventi, porta con sé un forte rischio di propagarsi ai Paesi vicini e di incidere negativamente sulla stabilità regionale. Il vile attacco contro il convoglio italiano di UNIFIL del 27 maggio l'attentato a Sidone contro il contingente francese e gli incidenti ai confini fra Libano e Israele e sul Golan sono un pericoloso indice di come la tensione possa diffondersi nella regione. Parimenti preoccupa il rilevante numero di rifugiati siriani che hanno attraversato la frontiera con la Turchia e il Libano, con potenziali effetti destabilizzanti sugli equilibri interni dei Paesi confinanti. Dall'inizio della crisi, la comunità internazionale ha seguito da vicino l'evolversi della situazione nel Paese. Da parte europea, abbiamo cercato (sin dal 27 marzo con un passo congiunto a livello europeo nei confronti del ministro degli esteri Moallem) Moallem) d'incoraggiare il regime di Assad ad intraprendere le riforme necessarie, lanciando appelli alla cessazione delle violenze e all'avvio, senza indugio, delle riforme. Ho io stessa trasmesso questo messaggio all'ambasciatore siriano qui a Roma lo scorso 6 aprile, mentre venivano contemporaneamente convocati gli ambasciatori siriani nelle principali capitali europee, esprimendo la nostra forte preoccupazione ed auspicando, da parte siriana, un processo di riforme che potesse portare la Siria sulla strada della democrazia e della tutela della legalità. Alla luce del perdurare delle violenze, sono state fino ad oggi adottate quattro tornate di sanzioni a livello europeo, in coordinamento con gli Stati Uniti, dapprima escludendo Assad, per un motivo di gradualità e per incoraggiarlo ad attuare le riforme, ma, con il protrarsi della repressione e la chiusura del Paese ai *media* e agli organismi umanitari, non abbiamo esitato ad indirizzare sanzioni individuali anche nei suoi confronti, cercando comunque di mantenere aperto un canale di dialogo. Anche a livello regionale, la Siria ha subito un raffreddamento dei rapporti con i suoi abituali interlocutori, primi fa tutti il Qatar e la Turchia, con i quali godeva di ottimi rapporti. L'inaccettabile assalto alle ambasciate francese e americana dell'11 luglio, a seguito della visita ad Hama dei rispettivi ambasciatori, ha allargato il divario esistente fra il regime siriano e la comunità internazionale. Il Consiglio affari esteri del 18 luglio ha adottato il documento "Conclusioni sulla Siria", in cui veniva rivolto alle autorità siriane un appello alla cessazione delle violenze, all'avvio delle riforme e all'accesso nel Paese di *media* ed organismi umanitari.

e ha fatto riferimento alla necessità di una condanna della repressione in atto nel Paese da parte del Consiglio di Sicurezza. Gli ambasciatori siriani nei principali Paesi dell'Unione europea, anche a Roma, sono stati convocati per rinnovare la condanna. Anche da parte statunitense è stata ulteriormente aumentata la pressione sul regime, con le dichiarazioni del segretario di Stato Clinton, che ha definito Assad «non indispensabile». In un tale contesto, in cui la comunità internazionale si interroga sulle numerose sparizioni di oppositori del regime che vengono riportate da diverse fonti, l'ultimo fine settimana ha fatto registrare un orrendo peggioramento della repressione attuata dal regime. campagna di arresti lanciata dalle forze di sicurezza per prevenire i disordini attesi nel periodo del Ramadan (iniziato il 1° agosto), l'ondata di violenze, perquisizioni e fermi indiscriminati che si è abbattuta sulle principali località della Siria teatro delle dimostrazioni antiregime, sembrano aver esacerbato la rabbia della popolazione. La situazione più grave e preoccupante è quella di Hama, dove da ieri all'alba è scattata l'operazione di "riconquista" della città da parte delle Forze armate e di sicurezza, con il supporto di mezzi blindati e carri armati. Già da settimane, da quando le dimostrazioni di massa in città (si è parlato di mezzo milione di persone) avevano costretto i presidi delle forze di sicurezza a ritirarsi dal centro abitato, Hama era stata circondata da un dispositivo militare che faceva presagire il peggio. Se finora le autorità siriane avevano esitato ad intervenire, consapevoli dell'attenzione internazionale attirata sulla città dalla visita degli ambasciatori francese ed americano e del valore simbolico che Hama riveste nella coscienza della comunità sunnita nazionale per le vicende dell'insurrezione della Fratellanza musulmana negli anni Ottanta e la repressione durissima di cui la città fu vittima nel 1982, nell'atmosfera prevalente in questa vigilia di Ramadan era inevitabile che essa venisse considerata come la questione più urgente da regolare. Le notizie che giungono dalla città mettono in luce un inaccettabile livello di violenza contro i civili. Carri armati e blindati starebbero attraversando le vie di Hama con il compito di riconquistare il territorio ai cittadini che in massa si sono ribellati e che avevano disseminato le strade di barricate e ostacoli improvvisati. Vi sono indicazioni che le truppe abbiano fatto ricorso massiccio ad armi pesanti, mentre i cittadini di Hama hanno lasciato intendere di essere determinati ad opporre resistenza. Nonostante sia stato per il momento impossibile condurre accertamenti, è verosimile che il numero delle vittime sia elevato e destinato a crescere ulteriormente con la prosecuzione dell'intervento militare. Oltre che a Hama, disordini si sono registrati nel fine settimana in diverse località. Nell'Est del Paese, Al Bukamal e Deir Ezzor sono state entrambe teatro di proteste ed episodi violenti, alcuni dei quali indicherebbero che tra gli animatori delle proteste ci sono ci sono frange capaci di mettere a segno anche azioni armate complesse. I pesanti arresti condotti nei giorni scorsi, che hanno coinvolto centinaia di persone, non sono riusciti a intaccare le dimostrazioni nei quartieri periferici e nei sobborghi intorno a Damasco, dove nel fine settimana si è registrata una nuova ondata di proteste. A Harasta, Barzeh, Douma, Madamya si sono svolte nuove dimostrazioni, con disordini tra manifestanti e forze di sicurezza. A Kanaker, cittadina a una ventina di chilometri a Sud di Damasco, nonostante la pesante spedizione punitiva messa a segno dalle forze dell'ordine la scorsa settimana, la popolazione è tornata a protestare con rinnovato vigore, dimostrando una volta di più che i metodi adottati per reprimere la contestazione si stanno rivelando controproducenti. Altre violenze si sarebbero verificate lungo l'arteria autostradale principale, che collega Homs a Hama, con scontri a fuoco tra Esercito regolare e gruppi di soldati che avrebbero defezionato. Anche nella provincia di Idleb, nel territorio intorno a Jisr al-Shagour, sarebbero presenti gruppi di disertori con i quali l'Esercito, che da giugno presidia l'area, si sarebbe trovato a ingaggiare scontri a fuoco. La stessa Daraa è tornata a sollevarsi contro il regime e a sostegno della popolazione di Hama. Anziché sortire l'effetto auspicato dal regime di intimidire e dissuadere la popolazione dallo scendere in piazza, gli ultimi avvenimenti mostrano un precipitare della situazione, che lascia presagire un ulteriore innalzamento della violenza e della repressione. Il Governo è profondamente sconvolto da questi orribili atti di violenza perpetrati dalle autorità siriane nel corso degli ultimi giorni, a Hama e in altre città del Paese, che hanno causato un numero intollerabile di vittime. La repressione nei confronti dei manifestanti pacifici deve essere abbandonata immediatamente. Nel puntare le armi verso il suo popolo la dirigenza siriana ha compromesso la propria legittimità. Il ministro Frattini ha, come sapete, rivolto un forte appello alle autorità siriane affinché interrompano, immediatamente e senza indugio, le operazioni delle forze di sicurezza e si astengano da ogni forma di violenza contro i civili. Coloro che sono detenuti illegittimamente devono essere subito liberati. I vertici siriani saranno ritenuti responsabili per le sconcertanti violazioni dei diritti umani effettuate nei confronti dei propri cittadini e, anche su forte impulso dell'Italia, abbiamo adottato ieri nuove sanzioni in ambito Unione europea contro il regime, che ha allargato la lista delle persone sottoposte a misure restrittive. Abbiamo inoltre sospeso i nostri programmi di cooperazione bilaterale con la Siria, ad eccezione del sostegno umanitario ai rifugiati iracheni. Apprezziamo il coraggio e la determinazione del crescente numero di siriani che continuano ad esprimere le proprie legittime aspirazioni attraverso pacifiche proteste, e con questo e con questo obiettivo abbiamo iniziato ad intraprendere alcuni contatti a livello tecnico con elementi dell'opposizione siriana in Europa. La comunità internazionale questa volta non può rimanere indifferente di fronte ai loro sacrifici. Quanto ai prossimi giorni, il mese del Ramadan, con l'apertura delle case a parenti ed amici, le preghiere collettive e la frequentazione assidua delle moschee polarizzerà certamente gli animi e potrà far capire, nei prossimi giorni, l'ampiezza effettiva e la forza della rivolta. Il segnale dato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che si è riunito d'urgenza, darà fiducia agli oppositori. hanno preso le distanze dal regime, quest'ultimo può tuttavia ancora contare sul sostegno iraniano e su un insieme di elementi che militano in favore dello *status quo*: l'incertezza del dopo Assad in un'area di grande rilevanza strategica; le preoccupazioni delle minoranze religiose per i nuovi assetti di potere, magari meno laici; la sfiducia che promana dalla transizione in corso in Egitto;

Ma il processo di riconciliazione nazionale, sia pure accompagnato e incoraggiato in tutte le maniere possibili, non potrà che essere endogeno. La Siria dovrà trovare in se stessa e nella sua storia millenaria la forza, la coesione e la visione per aprirsi ad un nuovo assetto di potere. È da auspicare che i tempi stiano maturando e che il Paese non voglia rassegnarsi alla reiterazione di un conflitto civile a bassa intensità. Per ora appare possibile ritenere che la crisi siriana non debba seguire il corso di quella libica. Il segretario generale della NATO Rasmussen ha escluso al momento l'ipotesi di un intervento militare. Ciò non preclude che si possa accrescere la pressione con misure di carattere diplomatico e sanzionatorio. Non è pensabile che la protesta venga schiacciata schiacciata nel sangue come avvenne nel 1982 nel silenzio della comunità internazionale. Dobbiamo convincere Damasco a fermare la repressione armata, prima che oltrepassi la soglia dell'irreparabile. L'unico tentativo realistico è l'iniziativa in corso a livello Nazioni Unite e Unione europea, per far capire all'ala dura del regime che deve cambiare rotta. La priorità, pertanto, è che alle Nazioni Unite si possa continuare a lavorare attivamente affinché venga raggiunto un consenso all'interno del Consiglio di Sicurezza per una ferma presa di posizione, al fine di continuare e rafforzare la necessaria pressione diplomatica sul regime siriano per interrompere le violenze e favorire al più presto l'avvio di una nuova fase. In questo quadro complesso, anche alla luce del sostegno unanime del Parlamento, il Governo intende continuare a mettere in opera tutte le iniziative diplomatiche più opportune per fare in modo che al popolo siriano, cui l'Italia non farà mancare né il sostegno, né la vicinanza, sia consentito di decidere del proprio futuro.

Sicurezza lavorasse giorno e notte (e lo fa solo in occasioni particolari e quando sono tutti d'accordo: questo non è il caso, perché ovviamente è una situazione diversa da quella della Libia, e ne conosciamo le motivazioni).

non sono successi solamente ieri o l'altro ieri, che era il giorno prima dell'inizio del Ramadan. Forse non tutti sanno (ma sicuramente i nostri colleghi in Aula ne sono informati, perché, se sono pochi, sono quelli che si interessano di estero)

e come sapete il Presidente della commissione siriana dei diritti umani ha parlato di più di cento civili uccisi ad Hama

condivido il ritiro dell'ambasciatore, ma a parte le letterine di prassi inviate a marzo ed aprile e gli inviti a smettere questo genocidio, non ho sentito altro da parte del del Governo. Interrompere i rapporti è una prassi, ma poi servono le iniziative. Ho ascoltato con attenzione quello che ha detto il Governo il Governo e ho riflettuto anche su quello che ho letto sui giornali, che è come aver ascoltato quello che ha detto il Governo, perché si tratta quasi di un copia-incolla di quello che stiamo leggendo in questi giorni. Serve quello scatto in più, che invece manca: mi sarei aspettato molto di più Da un Governo che con il regime degli Assad non ha stretto trattati bilaterali di amicizia folli, come quelli con la Libia, non solo ci saremmo aspettati qualche dichiarazione più pesante sull'accaduto, ma ci saremmo aspettati degli atti concreti contro il regime siriano.

Ciò detto, non significa che non si possa criticare il Governo per il suo modo di usare due pesi e due misure. Se in Libia, del quale regime eravate i più convinti sostenitori, state usando bombe umanitarie, perché in Siria - in cui non ci risultano grossi *business* in corso per il Governo - non proponete qualcosa di simile? Vedete colleghi, lo ripeto: per l'Italia dei Valori la politica estera dovrebbe essere qualcosa di diverso dagli interessi di uno Stato e basta. La diplomazia delle amicizie bilaterali, ed impresentabili, del Presidente Berlusconi ha fatto il suo tempo. E questo è un dato di fatto! Vedete colleghi, noi vorremmo che a dibattere di politica estera fosse l'Unione europea, con al suo interno un Paese fondatore quale l'Italia, saldamente ancorato alle prese di posizione dell'Unione stessa.

Ma non oggi e non la settimana scorsa, proprio come affermato dalla senatrice Contini, ma da mesi sono disponibili prove delle violazioni dei diritti umani accadute in Siria. Perché non si è fatto nulla da allora? Perché la diplomazia che siete chiamati a governare alla Farnesina non prova a proporre soluzioni, non belliche, ma preventive in questi casi?

Perché il nostro Paese non si adopera, anche tramite la sua *intelligence*, per porre le basi di una diplomazia preventiva in aree come quella di cui stiamo Quanto sta accadendo in questi mesi in Siria non è altro che la difesa di un regime dittatoriale che sente traballare la sedia su cui è seduto. Era normale, era scontato che sarebbe successo, così come è successo in Libia pochi mesi fa. Noi dell'Italia dei Valori avremmo voluto sapere che cosa ha fatto il Governo nei mesi scorsi al fine di informarsi correttamente, di stabilire contatti diretti con l'opposizione siriana, al fine di poter pensare di costruire una rete di tutela agli oppositori, così da poter organizzare eventuali azioni di supporto ai civili, da decidersi in un Consiglio di Sicurezza dell'ONU come al solito bloccato dal possibile veto di due regimi inqualificabili come quelli russo e cinese.

non ci sono il gas ed il petrolio che sono presenti in Libia, ma la comunità internazionale, noi cosiddetti occidentali abbiamo il dovere di tutelare la popolazione siriana, così come proviamo a tutelare altre popolazioni, in Libano, in Kosovo, in Africa ed in altri teatri in cui il supporto dei Paesi democratici è efficace rispetto al non proliferare della violenza. Ma al riguardo, voi siete totalmente sordi.

vedere tanti banchi vuoti sicuramente non può non creare in tutti noi una certa amarezza. Mi chiedo come pensiamo di poter riconquistare la fiducia della gente nei confronti della politica se per primi diamo questi questi segnali di disinteresse nei confronti di problemi così grandi che sconvolgono il mondo. Detto questo, signora Presidente,

D'altra parte, non possiamo immaginare un intervento militare oggi in Siria. Non lo possiamo immaginare per motivi geografici ed organizzativi, perché la Cina e la Russia hanno già dichiarato che potrebbero porre il veto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Credo che in Siria si stia verificando qualcosa di simile a quanto sta avvenendo in Libia. Credo che la considerazione che dobbiamo fare sia un coinvolgimento immediato e totale di tutta la comunità internazionale. Credo che linea giusta da seguire possa essere quella espressa dal presidente Obama, ossia cercare di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per isolare Assad. C'è da chiedersi se stiamo facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità. Abbiamo molto Abbiamo molto apprezzato l'intervento di ieri del ministro Frattini, che ha richiamato per consultazioni l'ambasciatore italiano in Siria. Sicuramente è un segnale e una formula diplomatica per mandare per mandare un messaggio a quel Paese, ma per mandarlo anche a tutta la comunità europea e internazionale. L'Italia, però, deve fare qualcosa in più per cercare di isolare Assad politicamente, ma anche nell'opinione pubblica internazionale. Potremmo anche arrivare alla sospensione delle relazioni diplomatiche, e sarebbe un segnale forte. Sarebbe però un segnale meno forte di quei cannoni di cui lei parlava, che uccidono e continueranno a uccidere centinaia di persone.

l'obiettivo di far cadere il regime di Gheddafi. Noi sappiamo che Assad è un macellaio, e non possiamo non dirlo con maggiore forza e maggiore convinzione dopo la strage di Hama di qualche giorno fa.

Gheddafi, hanno commesso dei crimini contro l'umanità, entrambi. Non ho bisogno di rimarcare che anche la globalizzazione può essere una grande occasione per l'umanità. Ma può essere anche un fatto negativo, se consentiamo che i commerci, le relazioni tra i popoli, la democrazia, il benessere, invece di di espandersi, si blocchino davanti alle porte della dittatura. Se viviamo un'era di globalizzazione, dobbiamo sapere che anche la libertà deve essere globale, e che la democrazia deve essere globale, ma non la si può esportare, sempre e comunque, con le armi. Allora la politica, e questo è uno di quei Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite deve fare

grandi problemi, che sta affrontando una grande crisi interna e internazionale. di essere coinvolti, di partecipare e di dare il nostro contributo anche a questi drammi. Da questo dibattito deve venire un messaggio forte e chiaro: il messaggio che il nostro Paese ha i suoi problemi, deve affrontarli e cercare di risolverli, ma non può e non deve dimenticare quanto accade nel mondo. E non può e non deve dimenticare quelle tradizioni di libertà e democrazia che fino ad oggi ci hanno contraddistinto.

Noi occidentali non potremmo mai concepire che l'Esercito spari contro la sua stessa folla. Ma le ultime dichiarazioni del presidente Assad, che addirittura si complimenta con l'Esercito per l'efficace opera di repressione, lasciano tutti noi stupiti. Siamo rassicurati anche per quanto ci ha detto il Sottosegretario, nel senso che l'Italia non potrà essere un protagonista di questa crisi siriana. crisi siriana. Infatti, le risorse del nostro Paese, ciò che noi dovremmo mobilitare, non sarebbero comunque sufficienti, e sono in ogni caso inadeguate, per un'azione militare, che noi indubbiamente non auspichiamo in questo momento. Il quadro che abbiamo è dei meno rassicuranti. Il Presidente siriano, lo sappiamo, è sostenuto dall'Iran, dalla parte radicale libanese, da Hezbollah. Dall'altra parte, chi si oppone a questo regime trova un appoggio velato dell'Arabia Saudita e, in parte, anche della Turchia. Sembra che gli Stati Uniti facciano leva proprio sulla Turchia per indurre il regime siriano ad un comportamento un tantino più responsabile e meno violento. Lei ci ha informati del Consiglio di Sicurezza che è tuttora in corso, ma a noi sembra che nessuna sanzione sia ancora arrivata in merito alla situazione siriana. Conosciamo le posizioni di alcuni membri del Consiglio di Sicurezza che in ogni caso porrebbero un veto: troviamo opposti ad un intervento in Siria la Russia, la Cina, il Brasile, il Libano ed anche il Sudafrica. La Turchia potrà fare poco, secondo noi, anche se sta tentando la via di una riappacificazione. C'è una gravissima crisi in Turchia

quattro sono i campi profughi già allestiti (però Erdogan, dichiarando: «Ospiteremo tutti coloro che fuggono da quel regime», si è già attirato le ire, in quanto, oltre a quella francese e a quella americana, sembra che anche l'ambasciata turca sia stata presa d'assalto I Paesi europei dovranno fare tutto ciò che possono: sensibilizzare e eventualmente sostenere sanzioni contro la Siria. La NATO, per mezzo del suo Segretario generale, ha detto che non vi sarebbero in ogni caso condizioni per un intervento militare. Siamo preoccupati per i nostri militari: abbiamo visto moltiplicarsi gli attentati contro i caschi blu dell'UNIFIL, e siamo presenti su quel territorio. Il quadro è ancora più complesso se lo esaminiamo sotto il profilo religioso: la nostra Chiesa sta chiedendo e raccomandando la via del dialogo, e sappiamo che tutti i cristiani del posto sono molto legati, ahimè, al regime di Assad,

forse solo in Siria un minimo di tutela. Indubbiamente, deploriamo il ricorso alla forza e, come Lega Nord, vorremmo che l'intero Governo si unisse a coloro che raccomandano in questo momento moderazione e prudenza. Vorremmo che il Governo italiano non assecondasse chi ipotizza l'uso della forza e, approfittando della presenza del Governo, vorremmo anche che questo episodio

sull'indirizzo tracciato dalla comunicazione tutt'altro che burocratica della sottosegretario Craxi, penso che il Governo italiano possa contare su un ampio sostegno parlamentare e certo su quello del nostro Gruppo e del nostro Partito. Si tratta naturalmente, in primo luogo, di sviluppare tutte le iniziative possibili per fermare la violenza e la repressione, che ha quel bilancio così aspro di cui l'onorevole Craxi ci ha parlato: 1.600 morti, 3.000 persone scomparse, decine di migliaia di persone arrestate. E tutto questo in una prospettiva che purtroppo, per le notizie e informazioni che abbiamo e che la sua comunicazione ha confermato, non è destinata ad alleggerirsi nelle prossime fasi. L'Italia ha fatto, a nostro parere, in queste settimane quel che doveva fare penso che oggi abbiamo il problema, come sempre in questi casi, del massimo coinvolgimento dell'Unione europea in primo luogo e, secondariamente, di avere dalla Comunità internazionale e dalle Nazioni Unite Unite posizioni che permettano queste iniziative. Non scopriamo oggi le difficoltà che esistono nelle Nazioni Unite, nella comunità internazionale. Sappiamo che l'espressione di una *governance* internazionale su questi problemi avviene in modo contraddittorio e faticoso. può pensare che questo problema sia superato d'improvviso. Tuttavia, questa è una cosa sulla quale bisogna continuare a muoversi con determinazione. Voglio sottolineare solo due aspetti che mi paiono particolarmente importanti: prima di tutto, penso che sia molto importante che l'impegno che oggi viene preso, anche, come la sottosegretario Craxi ha sottolineato, in una situazione di incertezza. Noi non stiamo sostenendo una causa della quale conosciamo con certezza l'esito. Noi sappiamo che, affidandoci ad un processo come quello in corso, tutti corrono dei rischi, perché è un processo

Questo è il quadro che ci si presenta, non solo in Siria, ma nell'insieme della regione. Forse qualcuno s'illudeva che le cosiddette rivoluzioni dei gelsomini arrivassero rapidamente ad uno sbocco chiaro. Oggi vediamo la complicazione di quei processi. Ma questo accresce la nostra responsabilità. L'Europa può giocare un ruolo molto importante per contribuire ad orientare verso uno sbocco di quelle situazioni,

perché noi non possiamo essere costretti ad un'alternativa tra passività di fronte alla violazione dei diritti umani o azione militare. Non può essere che solo attraverso questi due poli si svolga la dialettica politica nella comunità internazionale dove si effettuano le nostre scelte. Ma questo chiama in causa un problema che non mi stanco di ricordare: o i diritti umani e la della democrazia diventano una questione strutturale che fa parte organicamente della politica estera italiana ed europea, o noi ci troveremo in una situazione sempre più difficile. Naturalmente, è difficile pensare che siano alfieri di diritti umani i Paesi che non li praticano a casa loro. Nel Consiglio di Sicurezza noi verifichiamo tale situazione. Allora, bisogna che in tutte le direzioni questa politica venga tenuta aperta e che su questo ci sia una politica coerente: c'è infatti una relazione tra le politiche estere che conduciamo in generale su tutto lo scenario e quello che riusciamo a fare quando ci troviamo di fronte al precipitare di casi come questo. questo è il nostro orientamento e l'indirizzo. Di nuovo ringrazio la sottosegretaria Craxi per il suo intervento, che mi è sembrato chiaro e convincente.

del coordinatore, senatore Bettamio, e di tutto il Gruppo, anche per gli accenti di attenzione e per un risvolto che sta particolarmente a cuore anche a noi, non soltanto all'altra parte politica, ed è il risvolto di carattere umanitario. In tal senso, vorrei indirizzare il mio intervento, molto simile ad una testimonianza, in quanto proprio una settimana fa, come oggi, mi trovavo nei campi di raccolta di profughi siriani nella parte meridionale della Turchia, come membro di una delegazione del Consiglio d'Europa. Eravamo quattro parlamentari di differenti Paesi a testimoniare l'attenzione del Consiglio d'Europa per quel risvolto non secondario che anche il collega Marcenaro ha ricordato poco fa, vale a dire le conseguenze umanitarie per queste persone, oggi profughi, ma anche per coloro che sono rimasti in patria. Va detto subito che nei sette campi di raccolta che la Turchia ha egregiamente organizzato le condizioni sono più che soddisfacenti, salvo naturalmente i problemi ambientali, visto che ci sono dai 45 ai 50 gradi all'ombra di temperatura, con tutte le conseguenze per chi vive sotto autentiche tende, non sotto strutture in cemento. Va detto che altre condizioni, tre pasti al giorno e l'assistenza sanitaria, sono affidate alla generosità dei turchi, che egregiamente, con la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, stanno interpretando un ruolo esemplare. In uno dei campi visitati c'erano esattamente 1.800 profughi, 3.400 nell'altro, su un totale di 8.000 valutati oggi presenti, ma con una punta che ha toccato soltanto un mese fa i 16.000 sfollati. non si tratta, signora Sottosegretario, di un popolo in fuga, ma di persone in attesa di un rientro che danno per scontato e imminente. Non si tratta di un popolo arreso, ma di un popolo orgoglioso, anche in quella parte che ha deciso di fuggire e che è comunque in costante collegamento con chi è rimasto sul territorio. Va detto che l'esplosione di violenza registrata con l'inizio del Ramadan era stata ampiamente annunciata

autentici messaggi da portare verso l'Occidente. Sono messaggi, oltre che accorati, molto critici, come lei ha detto nel suo rapporto, nei confronti dell'Unione europea, dell'ONU, della NATO e di tutte quelle organizzazioni. Ci hanno detto esplicitamente: «Ma cosa state aspettando, forse che ci uccidano tutti? Perché siamo 23 milioni, tutti potenzialmente a rischio». «Non vogliamo aiuti umanitari» - hanno gridato - «abbiamo bisogno che ci aiutate a riconquistare la democrazia nel nostro Paese. Che cosa aspettate, che Assad faccia come fece suo padre nel 1982, quando, dopo aver promesso riforme democratiche, iniziò un repressione spietata che costò la vita» - queste cifre le hanno offerte loro - «a più di 400.000 persone?». Ora, anche il figlio ha promesso queste riforme, come lei ha ricordato, pochi giorni fa ha fatto votare in Parlamento una legge che allarga il contributo democratico ad altri partiti. Un giovane avvocato, che indossava quel che rimaneva di un doppiopetto gessato, scarpe senza lacci e senza calze, ha però ricordato che, finché c'è l'articolo 8 della Costituzione siriana, che dice che il solo partito abilitato a governare è il Partito Baath, quello di Assad, quale riforma è possibile? È una presa in giro, ha sottolineato lui stesso. Abbiamo il dovere di occuparci di queste persone, perché non chiedono aiuto con la mano tesa, ma

hanno sparato addirittura su un corteo funebre che andava a seppellire vittime precedenti. Al di là di questi episodi, che ormai fanno parte della cronaca quotidiana, credo sia arrivato il momento di dare una mano al nostro Governo a capire, e a far capire agli altri, che bisogna intervenire in maniera concreta,

è contenuta interamente nel documento stampato che all'esame del Senato. Sì tratta di un provvedimento che permette il raddoppio delle quote dei Paesi membri nel Fondo monetario: a seguito di un indirizzo dato dal G20 di Londra e della crisi finanziaria, era infatti importante che le risorse monetarie fossero aumentate.

non comporta degli esborsi diretti, ma soltanto di prestare garanzie. Il versamento della quota viene fatto dalla Banca d'Italia, e il Tesoro, quindi, garantisce. Non ci sono esborsi, né oneri per la Tesoreria: alla liquidazione del Fondo, ci potrebbero essere le garanzie date dalla Banca d'Italia, che dovrebbero essere confermate dal Tesoro. la Commissione ha approvato alcuni emendamenti, che recepiscono condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione

due categorie di disposizioni relative ai rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale. Le disposizioni del primo gruppo riguardano l'approvazione di emendamenti allo Statuto del Fondo monetario per consentire la riforma del consiglio di amministrazione, con l'obiettivo di rafforzare la presenza dei Paesi emergenti e in via di sviluppo attraverso la riduzione dei seggi europei. Tali proposte di emendamento allo Statuto del Fondo costituiscono una modifica di un accordo internazionale e, pertanto, devono essere approvate dagli Stati membri con le procedure specificamente previste. La seconda categoria di disposizioni riguarda l'autorizzazione al Governo a provvedere al quattordicesimo aumento della quota di partecipazione al Fondo dell'Italia, che passa da 7.882 milioni a circa 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo, proprio in attuazione di quanto stabilito a Seul, cioè al fine di assicurare una revisione generale che comporti il raddoppio delle quote del Fondo e una redistribuzione per riflettere i cambiamenti intervenuti nell'economia mondiale. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il disegno di legge non comporta aggravi di bilancio relativi al versamento della quota italiana, poiché esso è operato dalla Banca d'Italia con proprio fondi, costituendo una linea di credito a favore del Fondo in un conto corrente appositamente istituito presso la stessa Banca e regolato, relativamente ai rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, dalla Convenzione del 10 dicembre 2007. Gli unici esborsi eventuali potrebbero essere imputabili al versamento di interessi e di differenze di cambio sulle operazioni del Fondo monetario internazionale. Da un punto di vista tecnico, con riferimento alla concessione della garanzia dello Stato alla Banca d'Italia sui versamenti effettuati e da effettuare in favore del Fondo, sia la Ragioneria generale dello Stato che il Dipartimento del tesoro si sono più volte espressi in passato ed è sempre stato

che attribuisce alla Banca d'Italia i proventi derivanti dalla partecipazione italiana al Fondo, in quanto è la Banca d'Italia che versa sulle proprie disponibilità le quote dovute dallo Stato italiano al Fondo monetario internazionale. Da un punto di vista procedurale, si rappresenta che l'impegno assunto nelle sedi internazionali dai Paesi membri è quello di recepire l'incremento delle quote e gli emendamenti allo Statuto non più tardi delle riunioni annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale del 2012.

Tale modifica si fonda sulle seguenti motivazioni: i prestiti in favore del Fondo monetario internazionale sono stati sempre effettuati dalla Banca d'Italia sul presupposto dalla Banca d'Italia sul presupposto (politico e normativo) di una garanzia statale in favore della Banca per la copertura dei rischi connessi (di cambio, d'interesse, eccetera), e ciò in considerazione del fatto che la Banca opera come *agent* dello Stato italiano, che è il soggetto che si impegna con il Fondo monetario internazionale (scelta che, peraltro, è seguita anche da altri Paesi europei); il testo così riformulato è più aderente sia alla prassi da sempre vigente sia all'assetto normativo dei rapporti con il Fondo. Da ultimo, si evidenzia che, mentre in passato i rapporti con il Fondo erano gestiti da tutti i soggetti coinvolti in maniera più pragmatica e informale, da qualche anno si presta maggiore attenzione anche alla cornice normativa di riferimento e, quindi, alla precisione del dettato normativo, in modo che lo stesso sia il più chiaro possibile e senza margini di ambiguità. È stato inoltre necessario all'articolo 6, in conformità al disposto di cui all'articolo 25 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, eliminare l'improprio riferimento all'unità previsionale di base inserendovi il corretto riferimento ai pertinenti programmi e missioni programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello

e, poiché la maggior parte delle decisioni importanti del Fondo richiedono una maggioranza dell'85 per cento dei voti, l'Europa avrebbe, in effetti, un diritto di veto su ogni decisione importante del Fondo monetario, diritto di veto che oggi appartiene appartiene soltanto agli Stati Uniti, che hanno il 17 per cento dei voti. Pertanto, l'ordine del giorno G1, indicate queste considerazioni, invita il Governo ad intraprendere ogni iniziativa per giungere ad una rappresentanza unificata dell'Unione europea, per le ragioni che ho indicato. Mi auguro che possa essere sostenuto e approvato dal Senato.

proprio in questi giorni il sistema finanziario mondiale è sottoposto ad enormi pressioni, che ne hanno messo più volte in dubbio la tenuta. La Grecia è sull'orlo del baratro, gli Usa stanno combattendo un'importante battaglia contro il loro debito, in Italia abbiamo assistito alla farsa dell'approvazione di un decreto-manovra che di rigoroso - al contrario di quanto sbandierato dalla maggioranza - non ha un bel niente, se non la forza con la quale mette le mani nelle tasche e nelle case degli italiani (puntualmente dei meno abbienti).

in una crisi come quella attuale, se un po' di tranquillità può pervadere i nostri animi, questa è sicuramente data dalla presenza della moneta unica europea. Allo stesso modo, è fondamentale che l'Istituto nato nel 1944 e di cui l'Italia è membro dal 1947 (le cui competenze sono a noi ben note) sia messo in condizione di operare nel miglior modo. Fondo monetario internazionale siano molto importanti per consentire - appunto - la riforma del relativo consiglio di amministrazione, con l'obiettivo di rafforzare la presenza dei Paesi emergenti e in via di sviluppo, attraverso la riduzione dei seggi europei.

con cui si è ottenuta nel giro di pochissimo tempo la sostituzione del dimissionario Strauss-Kahn con una delle ministre del Governo francese, ritengo ancora più importante che le modalità di funzionamento del *board* di questo Fondo siano riviste tendendo il più possibile alla giustizia sociale ed all'inclusione di Paesi che, al di là delle loro economie e delle loro monete, rappresentano milioni, se non miliardi di persone. Un ultimo accenno è alla possibilità che con questa modifica dovrebbe diventare più probabile - del direttore esecutivo per l'Europa. Noi del Gruppo Italia dei Valori siamo fortemente favorevoli, perché convinti del fatto che solo un altrettanto convinto europeismo, nei fatti e non a parole (d'altronde questo Governo

che, in altro modo, comunque non arriverebbero mai, e che non sono arrivati con la diplomazia personale e collusa del Presidente del Consiglio. L'Italia dei Valori, anche alla luce della manovra appena licenziata dal Parlamento, voterà a favore di questo provvedimento, con l'auspicio che, allontanando quanto più possibile le decisioni dal livello del Governo italiano, possano discendere maggiori e più corretti frutti per la politica monetaria del nostro Paese lo ripeto, non ascoltando sicuramente le parole che un Presidente del Consiglio pronuncerà oggi e che avranno sicuramente un naso più lungo di quello di Pinocchio.

colleghi, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo su un provvedimento che, come ha bene illustrato il presidente Dini, si pone a conclusione di un processo abbastanza significativo e profondo di revisione da parte del Fondo monetario internazionale del proprio ruolo e del proprio potere di intervento sui mercati mondiali. Sappiamo che il Fondo monetario internazionale esercita dal 1945 un ruolo di promozione della cooperazione monetaria e del commercio mondiale, una funzione di sorveglianza che per la verità negli ultimi anni, a giudicare dai risultati, è stata alquanto deludente, una funzione di correzione degli squilibri e di assistenza ai Paesi membri che si trovano in difficoltà con la bilancia dei pagamenti. Per fare questo ha a disposizione una dotazione che gli viene dai Paesi aderenti, i quali contribuiscono con dei crediti dati per il 25 per cento in valuta nel tempo, il Fondo monetario ha più volte incrementato la propria dotazione attraverso aumenti generali (quello di cui si tratta oggi è il quattordicesimo), talvolta equiproporzionali, talvolta invece selettivi per rispecchiare un cambiamento dei pesi Queste quote non solo determinano la dotazione con cui il Fondo opera ma sono anche la base per l'assegnazione del potere di voto

una contribuzione di 180 milioni di dollari (allora non si usava ancora il diritto speciale di prelievo) che oggi è salita a 7,8 miliardi di diritti speciali di prelievo.

basato sul fatto che le quote dei vari Paesi vengono gradatamente riequilibrate per dare conto degli sviluppi dell'economia mondiale e di quali sono i Paesi oggi maggiormente dinamici.

luogo, l'approvazione degli emendamenti allo statuto, in particolare per quello che riguarda le regole sull'elezione dei membri del consiglio, della direzione generale, la determinazione dei cinque membri permanenti o nominati e la sostituzione con membri elettivi, quindi tutti diventano membri elettivi. Si tratta della modifica di un accordo internazionale, e quindi siamo in una legge di ratifica che è proprio quella che oggi stiamo discutendo. A seguito della nostra e delle altre ratifiche, queste modifiche del Fondo entreranno in vigore quando saranno approvate dai tre saranno approvate dai tre quinti dei Paesi che rappresentino almeno l'85 per cento dei diritti di voto. La seconda questione è l'aumento della partecipazione dell'Italia. Tecnicamente è la Banca d'Italia a farlo, quindi non comporta alcun aggravio nel bilancio dello Stato. Il Governo deve soltanto dare una garanzia nella remotissima ipotesi, in realtà, che il Fondo monetario risulti insolvente; ipotesi che è remotissima e che comunque come opportunamente ha fatto la Commissione bilancio - viene valutata zero, anche per un profilo di opportunità politica, perché se venisse valutata qualcosa vorrebbe dire che si mette in dubbio la capacità di solvibilità del Fondo monetario internazionale nell'ipotesi appunto di sua liquidazione e di restituzione ai Paesi membri del conferimento soltanto un piccola valutazione conclusiva di commento: certamente questo rafforzamento, sia di legittimazione che di potere di intervento, è una risposta doverosa, mi permetto di dire forse l'unica possibile che il Fondo monetario internazionale, non esente da colpe soprattutto sul fronte della sorveglianza, poteva Vorrei dire che è particolarmente opportuno rafforzare, attraverso il Fondo monetario internazionale, le possibilità di intervento di aiuto orizzontale fra Stati, posto che sempre più Paesi hanno inserito o discutono di inserire nella propria normativa, talvolta anche anche costituzionale, dei limiti o dei divieti di un aiuto verticale intergenerazionale, perché questo significa un indebitamento dal quale spesso non è facile tornare indietro. Il ruolo dell'Italia evidentemente, con questo aumento aumento parzialmente selettivo, diminuisce un pochino, perché il nostro aumento di quote è meno che un raddoppio, e infatti scende un pochino perché altre economie salgono, come salgono in effetti nel panorama economico mondiale. Faccio un'ultima osservazione di commento assolutamente favorevole rispetto all'ordine del giorno del senatore Dini che ci ha visti naturalmente favorevoli: l'Italia, che da sola non sarebbe in grado di esprimere un direttore esecutivo (lo fa soltanto grazie all'alleanza con con alcuni altri Paesi), esprime uno dei direttori europei, ma in realtà potrebbe essere molto opportuno - lo ha sottolineato anche il direttore Christine Lagarde in un suo recente intervento - che l'Europa si esprimesse con una voce sola. Poiché nella modifica dello statuto è anche inserito che le economie più avanzate dovranno presto rinunciare a due dei loro direttori, appare particolarmente opportuno che, anziché cercare ciascuno dei Paesi europei delle proprie alleanze spesso con Paesi anche lontani (l'Italia è alleata con Timor Est per esprimere il proprio direttore esecutivo), sarebbe forse meglio che l'Europa parlasse con una sola voce anche dal punto di vista dell'espressione di questo direttore, il quale peraltro rappresenterebbe il 35 per cento del potere di voto. In questo modo avrebbe un sostanziale diritto di veto, poiché la maggior parte delle decisioni importanti sono assunte con maggioranza qualificata dell'85 per cento, così come hanno un diritto di veto gli Stati Uniti che hanno da soli il 17 per

*(LNP)*. Signora Presidente, annuncio il voto favorevole della Lega Nord a questo provvedimento, che tra l'altro capita in una giornata emblematica, perché parleremo ancora di crisi

le quote di diritti speciali di prelievo italiane rimangono superiori a quelle dell'India, la metà di quelle della Cina e del Giappone. La proporzione è ancora a favore di quelli che sono i Paesi che hanno fondato La seconda considerazione, sempre a livello politico generale, è che comunque l'Europa detiene il 35 cento vuol dire che essa rimane il perno centrale su cui si muove l'intero sistema che fa capo al Fondo monetario internazionale.

Signora Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico a questo importante provvedimento. Un voto favorevole, perché non si può non essere favorevoli ad una riforma del Fondo monetario internazionale.

tuttavia, una riforma che affronta le due grandi novità che caratterizzano lo scenario internazionale oggi rispetto a quello di Bretton Woods e del mondo dell'epoca, del quale ormai

quei Paesi che chiamiamo ancora, con un'espressione del tutto impropria ed eufemistica, Paesi emergenti: sono in realtà emersi già da un bel po' e stanno contrassegnando con la loro forza e il loro protagonismo uno scenario dell'economia mondiale, e direi anche della geopolitica a livello internazionale, che è profondamente cambiato. Nel mondo di Bretton Woods i sette grandi erano sostanzialmente gli unici protagonisti dell'economia mondiale: era un *club* ristretto, nel quale, mettendosi d'accordo tra pochi grandi Paesi occidentali, l'ordine poteva regnare sull'economia internazionale. Oggi non è così: così: siamo in un mondo multipolare, non solo dal punto di vista politico e strategico, ma anche, e direi innanzitutto, da un punto di vista economico. Di questo mondo nuovo c'è un segnale ancora troppo parziale nel nuovo assetto del Fondo monetario internazionale e, tuttavia, un un cambiamento è iniziato. Il secondo grande cambiamento - quello cui si riferisce l'ordine del giorno Dini, che abbiamo condiviso e siamo lieti che il Governo abbia accolto

in particolare come potenza economica. Con i suoi 500 milioni di abitanti, l'Unione europea è la prima grande potenza mondiale, se solo avesse intenzione di esserlo davvero,

sono destinati a pesare sempre meno sullo scenario mondiale. Quel 35 per cento di quota europea all'interno del Fondo monetario internazionale è eloquente della forza straordinaria che che l'Europa rappresenta e, quindi, anche della straordinaria opportunità che prendere coscienza di questa forza e metterla a valore dal punto di vista politico e strategico, innanzitutto sul terreno

Signor Presidente, dopo tutto quanto è stato detto dal relatore, presidente Dini, dal sottosegretario Gentile e dai colleghi che mi hanno preceduto, annuncio innanzitutto il voto favorevole del PDL e mi limito a sottolineare gli aspetti

È un segnale positivo perché sottolinea come il Fondo sia molto più attento e più deciso nell'assistenza dei Paesi membri in difficoltà. Questo - come è stato rilevato - è un punto politicamente importante, anche nel quadro degli avvenimenti che, soprattutto nei Paesi emergenti - penso ai Paesi dei continenti africano e asiatico - si stanno verificano negli ultimi giorni.

Si tratta di un aumento nelle disponibilità del Fondo che dà la possibilità di redistribuire in maniera più decisa gli aiuti dai Paesi avanzati ai Paesi in via di sviluppo. fatto importante, perché la funzione del Fondo è di soddisfare le esigenze delle economie emergenti, e in questo quadro

e nuove istituzioni del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, nonché un assetto coerente, sinergico tra WTO, Fondo e Banca mondiale. In caso contrario, viviamo l'esperienza della attuale pesante crisi, che si rinnoverà nei prossimi anni, merci, senza far partecipare la propria moneta al libero mercato dei cambi, guadagnando fittiziamente quote importanti di competitività attraverso la furberia di di agganciarsi al dollaro e svalutare la propria moneta, il renminbi, insieme al dollaro. È la prima volta, in 3.000 anni di storia di questo pianeta, che un Paese con un enorme *surplus* commerciale vede svalutarsi, e non apprezzarsi consistentemente la propria moneta. Ne consegue, signora Presidente, un piccolo cenno critico al Fondo monetario internazionale, derivante dal fatto che l'Europa disunita e gli Stati Uniti d'America determinano una condizione di peso e potere politico economico da parte degli Stati Uniti rispetto allo stesso Fondo monetario internazionale. E questo non giova neanche agli stessi Stati perché c'è da chiedersi: se il Fondo viene ogni anno in Italia e negli altri Paesi a redarguirci, giustamente, e a dirci tutto ciò che dobbiamo fare per seguire un percorso equilibrato e consistente, come mai negli ultimi otto anni il Fondo monetario internazionale non ha mai attraversato il Potomac, che si trova poco distante, a Washington, per andare a redarguire il Governo americano, che stava sostenendo una crescita insostenibile dei consumi, con un *deficit* di partite correnti insostenibili, ed un accumulo di debito verso l'estero insostenibile, anche se finora è stato sostenuto, anche questo, dalla furbizia cinese? Ovviamente, avendo la Cina risparmi e avanzi si permette di comprare titoli di Stato e pezzi di economia reale, sia negli Stati Uniti sia in Europa, sia in Africa. Tutto questo assetto ha una una conseguenza concreta politicamente rilevante per l'Europa. Ho detto prima che l'equilibrio di potere di fatto tra gli Stati Uniti d'America e gli Stati sparsi d'Europa, è dovuto al fatto che non ci sono gli Stati Uniti d'Europa. Allora, la vera riforma dell'assetto economico istituzionale e internazionale nell'ambito della nuova *governance* presuppone che noi europei capiamo il più rapidamente possibile che l'Europa, nei prossimi mesi, nei prossimi anni e nei prossimi decenni, potrà essere presente e dare equilibrio al resto del mondo, solo se è presente come Stati Uniti d'Europa. Questa parola, che sembra un'utopia, è un'utopia urgentissima. E allora gli Stati Uniti d'America e gli Stati Uniti d'Europa potranno rimuovere il paradosso in corso, che è sotto gli occhi di tutti. Noi regaliamo competitività alla Cina: i soldi dell'Occidente vanno in Cina per comprare merci cinesi; i cinesi non li spendono e li risparmiano; con i nostri soldi risparmiati da loro ci ricomprano indietro l'economia occidentale, sia sotto forma di titoli di Stato sia sotto forma di pezzi di economia reale, dalla logistica, ai porti, alle grandi imprese manifatturiere. Forse qualcuno dovrebbe chiedersi

di governi G2, cioè di Stati Uniti e Cina, passando per l'asse del Pacifico, che è la prospettiva più pericolosa e più dannosa, non solo per l'Europa, ma per l'intero equilibrio dell'economia mondiale.

con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio e il 24 settembre 2010. Il disegno di legge in esame concerne le modifiche della disciplina concordata tra l'Italia e la Svizzera sulla navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano. La normativa attualmente in vigore, definita nel 1992 ed entrata in vigore nel 1997, deve essere rivista onde tener conto delle innovazioni sulla nautica da diporto previste nell'ordinamento italiano. La procedura di riforma ha visto il coinvolgimento, oltre che della Commissione mista italo-svizzera prevista dalla Convenzione vigente, anche delle Regioni Piemonte e Lombardia che si affacciano sui laghi. Vi risparmio il resto della relazione. Ricordo semplicemente che questo disegno di legge, che reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, non prevede oneri. Il rilascio dei contrassegni, infatti, comporta un minimo costo a carico del cittadino.

In questa occasione, vorrei ricordare all'Assemblea alcuni fatti che sono significativi, forse molto più della ratifica di questo Accordo. Attualmente vi è il blocco delle negoziazioni tra l'Italia e la Svizzera per il rinnovo dell'accordo fiscale (per essere molto sommario),

illecita riguardo agli accordi in vigore tra l'Italia e la Svizzera, bloccando il ristorno ai Comuni limitrofi italiani di oltre 50 milioni di euro delle tasse dei nostri lavoratori frontalieri. Da questa situazione bisogna uscire. Alla Camera dei deputati qualche settimana fa c'è stata una discussione importante sulla presentazione di una mozione dell'onorevole Narducci,

qui cogliere l'occasione per ringraziare il presidente Dini e il presidente Schifani, che hanno accolto una mia richiesta; il presidente Dini ha messo in moto proprio in questi giorni l'organizzazione, il 16 settembre prossimo in Senato, di un incontro

Vorrei solo portare una informazione all'Assemblea: quell'accordo fiscale può fruttare all'Italia svariati miliardi di euro, non stiamo parlando di un accordo di poca importanza con i tempi che corrono. anche se questa ratifica è un piccolo segnale, perché arriva a meno di un anno dalla conclusione dei lavori della Commissione, il 24 settembre 2010, e di abitudine impieghiamo 10 anni a ratificare gli accordi internazionali,

il quadro complessivamente positivo della collaborazione transfrontaliera, nonché la priorità che ad essa viene attribuita da entrambi i Paesi, anche se in un momento complesso delle nostre relazioni rispetto

aveva già avocato il coordinamento della questione, con l'obiettivo di riunire entro luglio un incontro bilaterale sulle questioni fiscali, con la partecipazione del MEF, del MAE e, per parte elvetica, di rappresentanti dei Dipartimenti federali delle finanze e degli esteri. Non è stato tuttavia possibile individuare una data utile prima della pausa estiva. L'esercizio è quindi stato rinviato a settembre. Al contempo, però, il Governo non ha mancato di far formalmente presente alla controparte elvetica, per il tramite della nostra ambasciata a Berna, la decisione del Consiglio di Stato del Canton Ticino di congelare il 50 per cento dei ristorni dovuti ai Comuni italiani configura una violazione dell'Accordo sull'imposizione fiscale dei lavoratori transfrontalieri del 3 ottobre 1974. Si è pertanto chiesto alle Autorità federali svizzere di porre tempestivamente in atto ogni opportuna procedura al fine di evitare che si produca una tale situazione sul piano del diritto internazionale. di oggi è importante. Questo Scambio di note è stato già ratificato da parte elvetica. Quindi, mi auspico che possa esserlo anche al più presto da parte italiana.

l'accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica e tecnologica con il Kuwait e l'accordo con la Federazione svizzera sulla convenzione di navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano. Per quanto concerne il primo accordo, vale la pena ricordare che il Giappone è un importante *partner* dell'Italia in ambito commerciale. L'Europa nel suo insieme possiede una quota di mercato di oltre il 15 per cento delle esportazioni in Giappone, l'Italia è il terzo Paese esportatore in Giappone dopo la Germania e la Francia, con un interscambio complessivo che si attesta in valore assoluto tra i 4 e i 5 miliardi di euro all'anno, sia per le esportazioni sia per le importazioni. L'accordo di oggi è di estrema importanza anzitutto perché il rafforzamento della collaborazione tra le amministrazioni doganali dei due Paesi rende molto più efficace la prevenzione e la repressione delle infrazioni e delle violazioni Inoltre l'accordo contribuisce alla semplificazione e all'armonizzazione di molte procedure doganali, aumentandone il grado di compatibilità con la moderna catena logistica internazionale,

della medesima, tra la Repubblica italiana e la Federazione svizzera. Si tratta di modifiche divenute necessarie a causa delle innovazioni introdotte nell'ordinamento italiano dalla nuova disciplina della nautica da diporto, poi confluita nella legge 8 luglio 2003, n. 172. Per adeguare la convenzione alle nuove disposizioni in materia sono state conseguentemente avviati i negoziati e a seguito di un'articolata opera di mediazione è stato raggiunto un accordo sulle modifiche da apportare alla convenzione e al regolamento. Come già spiegato dal relatore, sono state aggiornate diverse disposizioni tra le quali quelle relative alla circolazione, quelle riguardanti l'obbligo di patente nautica e quelle relative ai contrassegni, ora obbligatori anche per i natanti inferiori a 2,5 metri lineari, al fine di poter identificare le unità che eventualmente pongano in essere comportamenti in violazione delle norme di ordine pubblico e di sicurezza della navigazione. Si tratta, inoltre, di un accordo che non prevede alcuna clausola di copertura finanziaria, essendo il rilascio dei contrassegni posto a carico del cittadino. Come troppo spesso accade in relazione alle ratifiche degli accordi con il nostro Paese, la controparte, in questo caso la Svizzera, ha già provveduto alla ratifica dell'Accordo. Concludendo e sottolineando che l'Accordo contribuisce positivamente alle relazioni tra i due Paesi, dichiaro il voto favorevole mio e del Gruppo dell'Italia dei Valori in relazione all'Atto Senato n. 2741.

nei settori culturale, scientifico, tecnologico, dell'istruzione e dell'informazione. Si tratta di un Accordo di portata molto ampia che tende a sopperire alla mancanza, sino ad oggi, di una base giuridica per una migliore cooperazione in tali importanti settori. Il primo ambito di cooperazione è quello nel campo della cultura e delle arti. Sarà favorito l'insegnamento delle rispettive lingue e la cooperazione nella musica, nelle arti, nel teatro e nel cinema. In secondo luogo, è prevista la cooperazione nel settore dell'istruzione generale. Un terzo settore sarà quello della cooperazione nell'istruzione secondaria e nella ricerca scientifica e tecnologica. Il quarto e ultimo ambito di cooperazione è quello nel settore dell'informazione. Per l'attuazione dell'Accordo, si istituirà una Commissione mista che elaborerà programmi pluriennali ed accordi di attuazione. Ricordo infine che il disegno di legge di ratifica reca, oltre alle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche una clausola di copertura finanziaria pari a euro 242.460 per gli anni 2011 e 2012 ed euro 248.436 annui a decorrere dal 2013. La commissione

Signora Presidente, l'Accordo di cooperazione in materia culturale aggiunge un nuovo tassello al corollario normativo tra Italia e Kuwait e attesta la volontà del nostro Paese di rendere ancora più strutturata la già solida collaborazione e presenza nella regione del Golfo, coniugando apporto tecnologico e In questo modo sarà possibile rispondere ai nuovi bisogni culturali, scientifici, informativi, tecnologici e didattici che ci provengono dai Paesi del Golfo, e dal Kuwait, in particolare,

poiché è una delle rare volte in cui abbiamo a disposizione qualche minuto, visto che dobbiamo stare qui tutta la serata anche ad ascoltare altre persone che arriveranno più tardi, vorrei leggere in questi pochi minuti di voto. Quello al nostro esame è un Accordo di ampia portata, finalizzato a costruire una base giuridica ad oggi mancante per una migliore cooperazione in questi importanti settori. Con questo provvedimento si favorisce quindi la cooperazione nel campo della cultura, delle arti e nei settori dell'istruzione generale, dell'istruzione secondaria e della ricerca scientifica e tecnologia. Visto che ogni tanto parliamo di quel Paese che in questo momento ci sta restituendo solo morti, mi sento di dire che questo è il compito di un'Italia, che non dovrebbe partecipare ad azioni come quelle in Afghanistan, ma cooperare nel campo della cultura, delle arti, dell'istruzione e della sanità (cosa, questa, che mi sembra evidente il ministro La Russa non abbia ancora capito). Grazie a questo Accordo sarà quindi favorito l'insegnamento delle rispettive lingue, saranno avviati scambi di materiale didattico, incentivati accordi sui titoli di studio, nonché valorizzati gli accordi tra università, incentivando altresì lo scambio di visite di professori e ricercatori. Infine, un'attenzione particolare, soprattutto tenendo conto dell'era in cui viviamo, è dedicata alla cooperazione nel settore dell'informazione, attraverso scambi di programmi televisivi e radiofonici. Dalla breve analisi di questi elementi emerge lampante come la finalità del provvedimento oggi in esame sia quella di migliorare e fortificare i legami di amicizia tra i due Paesi, promuovendo la comprensione e le conoscenze reciproche. Concludendo e sottolineando l'importanza dell'Accordo, che consolida la presenza italiana nei Paesi del Golfo e che consente un miglior interscambio culturale, oltre che scientifico ed informativo, con il Kuwait,

Grazie, Presidente. nell'implementazione di questo Accordo, una vigilanza sul terreno dei diritti umani e delle libertà civili quando si tratta di questi Paesi (è giusto ricordarlo), nel dialogo e nel confronto da posizioni assolutamente paritarie, senza nessun paternalismo, però anche con la fermezza che è necessaria nel ricordare i diritti della persona umana (in particolare delle donne).

stimolo per iniziative in tutti questi campi. Abbiamo il piacere di mettere questi due mondi in relazione. Siamo due mondi molto diversi: noi rappresentiamo l'Occidente, mentre loro rappresentano

portare in quel Paese musica, arte, teatro e cinema italiano servirà a far capire meglio l'altra parte del mondo, che ancora, in una parte del globo, viene vista con molta diffidenza.

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario (anzi lo integra) ed il Asuo campo di applicazione impone l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure doganali, per garantire la sicurezza della catena logistica internazionale. Sappiamo quanto è importante il Giappone come *partner* economico ma, in particolare, commerciale dell'Italia, come diceva prima la senatrice Contini. Il disegno di legge prevede una copertura finanziaria pari a 16.000 euro circa a decorrere da quest'anno e le spese sono allo scambio di funzionari per le attività di accertamento delle infrazioni e di assistenza tecnica. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. **Parere esteri*. Signora Presidente, mi preme solo sottolineare come questo Accordo di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale è il primo trattato di natura intergovernativa che l'Agenzia delle dogane abbia firmato con un Paese asiatico.

*(IdV)*. Signora Presidente, intervengo brevemente in relazione all'Atto Senato n. 2743, relativo alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone.

un testo che nessuno leggerà. In questo modo, almeno si ascolta. Con questo provvedimento in materia doganale il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone si impegnano a darsi reciproca assistenza e cooperazione per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare il rispetto della legislazione doganale e di prevenire ogni possibile violazione della relativa normativa. Proprio a questo scopo diverse disposizioni dell'Accordo sono dedicate all'attività investigativa e di repressione delle violazioni. Si tratta di un provvedimento, composto da 19 articoli e un preambolo, che contiene una disciplina giuridica della materia appropriata, finalizzato alla semplificazione delle procedure doganali, che si caratterizza, tra l'altro, per l'introduzione, salve specifiche ipotesi di deroga, dell'obbligo dello scambio di informazioni e dell'assistenza, su richiesta e spontanea. Concludendo, e sottolineando che l'Accordo contribuisce positivamente alle relazioni tra i due Paesi, dichiaro il voto favorevole mio e del Gruppo dell'Italia dei Valori in relazione all'Atto Senato n. 2743. Spero che anche nelle prossime ratifiche ci sia data la possibilità di motivare, anche in parte, il voto favorevole, come stiamo facendo oggi, senza essere obbligati a consegnarlo per una velocizzazione dei tempi e, più che altro, per una velocizzazione dei viaggi,

dal punto di vista economico (è stato scavalcato da poco tempo dalla Cina). Sono stati poc'anzi rammentati i cambiamenti nella geopolitica e nella geoeconomia

Giappone, con il quale esistono molti Accordi e Trattati di amicizia e di collaborazione in campo economico, in campo commerciale e in campo culturale; abbiamo ottimi rapporti, che forse potrebbero essere anche molto più stretti di quanto non siano, viste le caratteristiche storiche ed economiche dei due Paesi. è in grave sofferenza l'Istituto di cultura italiano a Kyoto. Spero - vedo che la sottosegretaria Craxi fa cenno di essere pienamente al corrente della situazione - che i problemi di questo Istituto, che è un fiore all'occhiello della cultura

a lei e a tutti i signori senatori di questo ritardo, ma abbiamo ritenuto di dover mantenere la nostra presenza fino alla fine ed ascoltare tutti gli interventi che i deputati hanno voluto fare a seguito dell'intervento che ho svolto, appunto, alla Camera dei deputati. Sono stato alla Camera e sono qui per fare il punto sulla attuale situazione economica del nostro Paese, sulle conseguenze della crisi internazionale e sulle decisioni che il Governo ha assunto e che intende assumere. È a tutti chiaro che i problemi e le emergenze che in queste ultime settimane abbiamo dovuto affrontare sono la diretta conseguenza di una crisi di fiducia che scuote i mercati internazionali, una crisi che non accenna a placarsi tanto per l'incertezza sull'euro, quanto per la spinta della speculazione finanziaria. Questa crisi deve essere fronteggiata con fermezza, con coerenza, senza inseguire i nervosismi del mercato finendo così, se li seguissimo, per alimentarla. per fortuna ha un sistema politico solido, che si è dimostrato capace, con il concorso responsabile dell'opposizione, di approvare in soli tre giorni una manovra di quasi 80 miliardi di euro, raccogliendo in questo modo l'invito alla coesione nazionale avanzato dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Abbiamo fondamentali economici solidi. Le nostre banche sono liquide, sono solvibili ed hanno superato brillantemente gli *stress test* voluti dall'Unione Europea. Abbiamo registrato segnali significativi di ripresa, pure in una congiuntura che è altalenante. Nel mese di luglio si è registrata una decisa diminuzione delle ore complessivamente autorizzate della cassa integrazione guadagni rispetto a quelle dello stesso mese di un anno fa: meno 28,8 Quindi, non è venuta meno, in Italia, la voglia di fare impresa, di investire, di superare le criticità che pure permangono. Il Parlamento ha approvato il 6 luglio una manovra economica diretta ad assicurare, attraverso provvedimenti adottati nell'immediato, l'obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2014, condizione che determinerà la conseguente stabilizzazione strutturale del debito e la sua progressiva riduzione in rapporto al PIL.

appare essere meno brillante degli altri Paesi, soprattutto per quanto riguarda la differenza, lo *spread* con i titoli germanici? Credo che tutti siamo consapevoli del perché: oggi l'Italia ha il quarto debito pubblico abbiamo il 120 per cento rispetto al prodotto interno lordo, ed è un'eredità che ci è stata consegnata dai Governi precedenti, che dal 1978 al 1980 hanno moltiplicato per molte volte il debito pubblico. La manovra che abbiamo approvato il 6 luglio è stata concepita in coerenza con gli obiettivi fissati in sede europea, secondo quanto ci è stato richiesto dalla Commissione europea ed è stata dall'Europa giudicata adeguata e sufficiente, così come da tutti gli altri osservatori internazionali, anche e soprattutto, direi, in relazione ai tempi in cui è stata approvata. Questa stessa mattina il presidente dell'Eurogruppo, Juncker, ed il commissario agli affari economici, Olli Rehn, ricevendo il ministro Tremonti, hanno manifestato il loro apprezzamento e la loro fiducia rispetto situazione che l'Italia sta affrontando. Successivamente al Consiglio dei ministri di questa mattina ho avuto una cordiale telefonata con il presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, che mi ha manifestato gli stessi apprezzamenti. Quindi, io credo che dobbiamo approfondire l'analisi della situazione per cui oggi siamo qui, a cominciare dall'andamento dei mercati finanziari: ovunque è aumentata l'incertezza sull'intensità della crescita nel mondo, in particolare nei Paesi che trainano tutte le altre economie, in America ed in Giappone.

Negli Stati Uniti le difficoltà di raggiungere un accordo sull'innalzamento del limite del debito pubblico ed il conseguente rischio di *default* hanno indotto una ricomposizione dei portafogli degli investitori tutta a favore degli investimenti a breve termine. L'accordo *bipartisan* tra democratici e repubblicani che è stato appena raggiunto non pare avere ridotto le tensioni internazionali. Le turbolenze sui mercati finanziari hanno tratto alimento anche dalla percezione di un'eccessiva lentezza nella reazione delle autorità europee alla crisi del debito sovrano innescata dalla situazione greca. Il 21 luglio scorso il Consiglio europeo ha approvato un nuovo programma di assistenza per la Grecia, volto ad assicurarne pienamente le esigenze di finanziamento e a migliorarne radicalmente la sostenibilità del debito, con tassi di interesse più bassi, con scadenze più lunghe e, alla fine, anche con il coinvolgimento del settore privato. Il Consiglio ha anche ampliato la capacità del Fondo europeo di stabilità finanziaria di intervenire nella gestione delle crisi con maggiore flessibilità e con maggiore forza economica. Sono decisioni importanti, di grande portata, anche se i mercati non riflettono ancora l'importanza degli interventi che sono stati così deliberati. È quindi essenziale dare certezza ai mercati definendo con chiarezza i tempi, gli strumenti e le risorse a disposizione rispetto agli interventi che sono stati decisi. I rischi di contagio influenzano le scelte degli investitori istituzionali europei, orientandoli in favore delle attività ritenute meno rischiose, in primo luogo i titoli del debito pubblico tedesco,

Queste tensioni hanno elevato il differenziale tra il rendimento dei buoni del tesoro decennali e quelli del corrispondente titolo tedesco fino ai massimi storici dall'avvio dell'unione monetaria, in occasione dell'ultimo collocamento dei titoli pubblici - come sapete - i rendimenti sono saliti di oltre un punto percentuale. Come spesso accade nelle crisi di fiducia, i mercati non appaiono valutare correttamente il merito di credito: le valutazioni degli investitori sui nostri titoli non tengono nel giusto conto la solidità del nostro sistema bancario, la salda posizione patrimoniale delle nostre famiglie e delle nostre imprese, il contenuto indebitamento estero del Paese, l'assenza di squilibri nel settore immobiliare, la nostra politica commerciale, che ci vede in avanzo, la prudenza seguita nella conduzione della politica di bilancio durante la crisi. Si tratta di punti di forza che in più di un'occasione hanno spinto le autorità europee a considerare l'Italia in condizioni di assoluta sicurezza, e lo ha riconosciuto poco tempo fa anche il presidente della Commissione europea Barroso, che ha definito «chiaramente ingiustificate» le pressioni sul nostro mercato. Le nostre banche hanno superato con le loro sole forze la crisi finanziaria, hanno assorbito le ingenti perdite sui crediti provocate dalla profonda recessione dell'economia reale; nei mesi scorsi hanno fatto ricorso con assoluta tempestività al mercato dei capitali, dotandosi delle risorse patrimoniali sufficienti a fronteggiare anche eventi particolarmente sfavorevoli hanno superato brillantemente gli *stress* *test* condotti a livello europeo. Anche la raccolta obbligazionaria effettuata non sul mercato interno ma sui mercati internazionali, è stata cospicua e sufficiente a far fronte al rimborso dei titoli nell'intero anno. Le banche italiane dunque si presentano oggi ben capitalizzate, in grado di sostenere la ripresa dell'economia ed in grado di soddisfare le esigenze finanziarie delle famiglie e delle imprese. Anche per questo motivo, da noi la crescita del credito al settore privato è attualmente superiore a quella degli altri grandi Paesi. Il saldo radicamento sul territorio ha consentito alle banche di espandere la raccolta presso le famiglie, sotto forma sia di depositi sia di obbligazioni. La redditività, già in miglioramento, beneficerà dell'espansione dei prestiti, del miglioramento della qualità del credito e del contenimento dei costi perseguito dalla quasi totalità degli istituti bancari. I ribassi dei corsi azionari delle nostre banche che si stanno verificando sono assolutamente eccessivi. Per i maggiori istituti, i valori di mercato oggi sono di gran lunga inferiori ai valori di bilancio. Questo per Anche il settore privato italiano - famiglie e imprese - è caratterizzato da condizioni finanziarie solide. Le famiglie sono contraddistinte dal più basso indebitamento in rapporto al PIL tra i maggiori Paesi, con un valore pari a meno della metà di quelli del Regno Unito e degli Stati Uniti, e tre quarti di quello della Germania. La loro ricchezza finanziaria è particolarmente elevata nel confronto internazionale. Se aggiungiamo al debito pubblico il debito privato, saliamo al secondo posto in Europa, appena sotto la Germania, e prima di Paesi come la Svezia, la Gran Bretagna e la Francia. Anche i debiti delle nostre imprese sono assolutamente contenuti in rapporto al loro fatturato. Questa è la situazione che riguarda la nostra economia. Ma veniamo al nostro debito pubblico, che è la grande eredità negativa, lo voglio ripetere, perché ancora non vedo consapevolezza di che cosa significhi per un Paese avere questo debito pubblico ereditato dal passato. Dopo lo scoppio della crisi, l'evoluzione dei nostri conti pubblici è risultata, nell'insieme, più favorevole di quella della gran parte dei Paesi avanzati. era evidentemente peggiorata; nel 2009 il *deficit* aveva superato il 5 per cento del PIL, valore che però era, ed è, inferiore a quello registrato dagli altri grandi Paesi dell'area dell'euro. Con la ripresa dell'attività economica e grazie alla nostra azione di finanza pubblica, questi conti sono migliorati. Nel 2010 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è sceso di quasi un punto percentuale in rapporto al PIL il disavanzo primario si è sostanzialmente annullato. Il *deficit* di bilancio è risultato meno ampio di quanto avevamo noi stessi prudenzialmente indicato come obiettivo: come ricorderete, il 5 per cento, per l'anno in corso. Ancora una volta questo *deficit* è risultato significativamente più basso di quello degli altri Paesi dell'area dell'euro, che si è situato su una media del 6,3 Il sentiero di riduzione del deficit che abbiamo concordato in sede europea viene percorso nei fatti più rapidamente: è quello che ci chiedono ancora la Commissione europea e gli altri Paesi europei, ed è quello che cercheremo assolutamente di fare. Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone hanno registrato disavanzi annuali compresi tra il 9 e l'11 per cento del loro PIL. Nel maggio scorso, invece, noi abbiamo definito la manovra di bilancio per il triennio 2010-2012, volta a condurre il disavanzo cento del PIL quest'anno e al 2,7 per cento del PIL l'anno prossimo, in linea con il piano concordato in sede europea per il rientro dalla situazione del disavanzo eccessivo. I dati relativi al fabbisogno del settore statale per i primi sette mesi di quest'anno sono coerenti con l'obiettivo che ci siamo posti, e cercheremo nei prossimi mesi di ridurre assolutamente questo fabbisogno. Con il decreto-legge manovra il Consiglio dei ministri ha approvato un percorso di finanza pubblica che porterà quindi al pareggio di bilancio entro il 2014. Le misure del decreto-legge sono state, come sapete, ulteriormente rafforzate nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione in legge. Questi interventi ci consentiranno di avviare una rapida riduzione del peso del debito pubblico in rapporto al PIL,

Con il collegamento, fin dal 2013, dell'età di pensionamento all'andamento delle aspettative di vita e con gli altri interventi in materia di previdenza abbiamo ulteriormente rafforzato la solidità dei conti pubblici nei prossimi decenni. Le riforme introdotte negli ultimi anni, infatti, pongono l'Italia tra i Paesi europei in cui la pressione esercitata dai regimi previdenziali sui conti pubblici sarà la più contenuta. La riforma che abbiamo, che avete approvato in questa legislatura è stata presa a modello da molti Paesi europei. Quindi, non abbiamo fatto poco. Sappiamo - certo - che c'è ancora molto da fare. Lo sforzo di contenimento della spesa deve fondarsi sempre su efficaci procedure di *spending review* (direi che questo è uno sforzo che dobbiamo perseguire quotidianamente), che rendano strutturali i risparmi di spesa. Occorre anche un piano di azione immediata che risponda agli sviluppi dei mercati. Dobbiamo considerare interventi che sostanzialmente azzerino - l'ho appena detto, ma voglio ripeterlo - il fabbisogno finanziario nell'ultima parte di quest'anno. Questo sforzo dovrà integrarsi con il crescente decentramento delle decisioni previste dal federalismo fiscale. Dobbiamo migliorare la qualità dei servizi pubblici e della regolamentazione, che sempre più incidono sulla nostra capacità competitiva e sulle nostre prospettive di crescita. Dobbiamo - infine - liberare maggiori risorse per investimenti, chiamando alla collaborazione anche gli investitori privati. Quindi, è essenziale che Governo e Parlamento attuino in tempi brevi la delega fiscale e assistenziale, definendo un regime di tassazione che modernizzi l'Italia e che sia più favorevole alla famiglia, al lavoro e all'impresa. Ma, certamente, è la crescita l'obiettivo essenziale. In quest'ottica, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha questa mattina dato concretezza al Piano per il Sud, con la destinazione immediata di 7,4 miliardi di euro per la realizzazione di circa 130 interventi che rilanceranno l'economia del Mezzogiorno. Oggi ho anche firmato due decreti. Il primo istituisce la Commissione governativa, affidata all'autorevole guida del Presidente dell'ISTAT, che fornirà le che fornirà le informazioni necessarie per procedere al livellamento retributivo dei titolari di cariche elettive e dei vertici delle Amministrazioni italiane rispetto agli standard europei. Il secondo decreto definisce invece modalità e limiti di utilizzo delle auto di servizio - le cosiddette auto blu - al fine di ridurne il numero e i costi.

per la crescita e per la coesione sociale, che dovrà accompagnare il Programma di stabilità e il Piano nazionale delle riforme che abbiamo presentato a Bruxelles nel maggio scorso. La crescita dell'economia e dell'occupazione è la conseguenza soprattutto della positiva convergenza dei comportamenti responsabili degli attori istituzionali, economici e sociali. Per questo ci adopereremo per un'intesa tra Governo e organizzazioni rappresentative delle imprese e del lavoro sui modi con cui realizzare un'efficace unità di intenti. Questo confronto dovrebbe riguardare, in particolare, quattro punti: il ruolo delle banche e dei finanziamenti alle imprese; le relazioni industriali, tanto nel settore privato quanto nel settore pubblico. L'emergenza della situazione finanziaria ed economica descritta ci impone, come ho già detto, di dare una risposta ancor più forte, immediata e visibile sul piano dell'impegno per la crescita, che renderà credibile e sostenibile il piano di stabilizzazione finanziaria. Nel merito, desidero anticipare al Parlamento i temi del confronto con le parti sociali. La gestione della manovra riguarda tanto le misure approvate che quelle da approvare attraverso il disegno di legge delega di riforma del sistema fiscale e assistenziale. Il monitoraggio congiunto degli investimenti infrastrutturali consentirà di verificare tempi e modi dell'effettivo trasferimento di risorse pubbliche, consentirà di controllare la spesa effettiva dei concessionari e licenziatari di servizi nazionali di pubblica utilità, a partire dalle nuove reti di telecomunicazione, consentirà di verificare l'efficacia delle misure rivolte ad accelerare i procedimenti di esecuzione (questa è davvero una piaga del nostro sistema) consentirà di rimuovere, insieme, le strozzature che rallentano l'esecuzione delle opere. Il ruolo delle banche e della finanza di impresa è ancor più necessario in un contesto di prolungata difficoltà per molte attività produttive. Oltre alle intese tra banche e associazioni di imprese per garantire la necessaria liquidità, Governo e parti sociali verificheranno tempi e modi di operatività dei nuovi strumenti di sostegno finanziario alle imprese. Le relazioni industriali, soprattutto in un Paese che ha conosciuto elevati livelli di conflittualità sociale, costituiscono uno strumento fondamentale per attrarre investimenti quando garantiscono un'adeguata produttività attraverso la piena utilizzazione degli impianti e la tregua sociale. Il Governo ha da tempo proposto alla valutazione delle parti sociali una bozza di riforma dello Statuto dei lavoratori che abbiamo voluto chiamare Statuto dei lavori. È giunto il momento di verificarne il grado di consenso, per procedere all'esame parlamentare. Lo sviluppo della contrattazione territoriale o aziendale è altresì sostenuto dalla proroga della detassazione e della decontribuzione degli incrementi retributivi che genera. Al tempo stesso, il Governo garantisce, anche per il prossimo anno, un'adeguata dotazione di risorse per gli ammortizzatori sociali che dovremo, ancor più, collegare con le attività di ricollocamento e riprofessionalizzazione dei lavoratori. Le nuove norme in materia di pubblico impiego incentivano interventi di razionalizzazione e riqualificazione delle amministrazioni pubbliche garantendo incrementi retributivi legati alla produttività individuale e collettiva attraverso la contrattazione. Non intendo sorvolare sui costi della politica, di cui si fa un gran parlare. Cerco di farlo senza demagogia. Sulla base di quanto previsto dal decreto-legge manovra, il Governo agirà per contenere tutti gli emolumenti delle alte professionalità pubbliche, elettive e non, riconducendole ai valori medi europei. Inoltre, il Governo, attraverso la riorganizzazione delle Province (difficile ma necessaria), riorganizzazione connessa con la diffusa aggregazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, già prevista dal decreto sul federalismo municipale, potrà pervenire ad un ulteriore contenimento della pressione fiscale e ad una ben maggiore efficienza nella gestione dei servizi locali. Sapete tutti, del resto, che il Consiglio dei ministri ha già approvato la riforma costituzionale che porterà a dimezzare il numero dei parlamentari e a contenere i tempi e i costi dell'attività legislativa. Sarà possibile anche compiere una verifica congiunta sulla ragione di essere di società ed enti dello Stato, chiedendo la stessa riflessione in ciascuna dimensione regionale con lo scopo di procedere a liquidazione o perlomeno a fusioni. Onorevoli senatori, prima di concludere vorrei ricordare che la crisi finanziaria ha colto il nostro apparato produttivo nel corso di un processo di adattamento alle nuove tecnologie ed alla globalizzazione. Ne ha risentito la crescita, da tempo meno intensa di quella degli altri Paesi dell'area dell'euro, per effetto delle eredità del passato e dei nodi strutturali che frenano il nostro sviluppo. Prima con il decreto sviluppo e poi con la manovra di bilancio triennale, il Governo, coerentemente con quanto fatto fin dal 2008, ha introdotto ventisette misure concrete per sostenere la crescita economica del Paese: relative alla fiscalità di vantaggio per imprese e cittadini; cinque in materia di semplificazione e liberalizzazione; quattro per aumentare l'efficienza della giustizia; ben undici di incentivazione al sistema produttivo; tre di valorizzazione del capitale umano. A questo riguardo, mi preme sottolineare le misure che riconoscono un credito di imposta a favore delle imprese che investono in ricerca scientifica e una tassazione secca del 5 cento, l'aliquota più bassa d'Europa, a favore delle imprese guidate da giovani sotto i 35 anni si è fortemente, direi quotidianamente, impegnato anche per la soluzione delle crisi aziendali. Solo negli ultimi otto mesi sono state risolte ben trenta vertenze. Grazie all'azione del Governo, alla voglia e alla capacità di reagire del tessuto imprenditoriale italiano e alla stretta collaborazione con i sindacati, siamo riusciti a garantire un futuro stabile e produttivo a tante aziende e a tante famiglie. Restare al fianco di chi lavora e produce è uno dei modi più efficaci che abbiamo per contrastare la crisi. Continueremo a lavorare su questo fronte difficile, consapevoli che la difesa e l'innovazione del nostro apparato produttivo sono fondamentali per la ripresa economica del Paese.

che si è riflesso anche nel loro recente appello sulla necessità di accelerare l'azione di rilancio della crescita. Ricordiamo a noi stessi e a tutti: il Paese è economicamente e finanziariamente solido. Nei momenti difficili sa essere coeso e sa affrontare le difficoltà. il Parlamento agiranno - mi auguro - con un ampio consenso politico-sociale per affrontare ogni minaccia alla nostra stabilità finanziaria. Oggi più che mai dobbiamo agire tutti insieme. Raccolgo con convinzione l'invito alla coesione nazionale che il presidente Napolitano ha sollecitato più volte: è un monito saggio che faccio mio: nelle difficoltà tutti hanno il dovere di rimboccarsi le maniche. Il nostro dovere, quale che sia la nostra collocazione politica, è di operare per il bene dell'Italia e per costruire la ripresa dell'economia, facendo ciascuno la propria parte e ricordando che la stabilità politica è da sempre l'arma vincente contro la speculazione. Onorevoli senatori,

Non chiedo alle opposizioni di condividere il nostro programma, ma auspico vivamente che possano contribuire con le loro idee e con le loro proposte a fare emergere sempre di più ciò che serve al Paese. *(Applausi cioè, che le opposizioni facciano ciò che sono state chiamate a fare, ma lo facciano senza mai perdere di vista il comune obiettivo, perché comune sono certo sono certo che sia l'obiettivo di portare l'Italia fuori da questa crisi, che non è italiana ma planetaria. Assicuro che il Governo non resterà sordo alle vostre idee e alle vostre proposte quando esse saranno animate da questo spirito patriottico. Al Governo spetterà di fare per intero il proprio compito di completare il proprio lavoro, un lavoro cui gli italiani ci hanno chiamato nel 2008 e che completeremo nel 2013, quando ci sottoporremo nuovamente al loro giudizio, con la serena coscienza di chi ha fatto tutto il possibile per il proprio Paese in anni così difficili. Nei venti mesi che ci separano da quell'appuntamento, il Governo farà il Governo: completerà il percorso delle riforme già all'attenzione del Parlamento, rafforzerà sempre di più il rapporto con le parti sociali e proporrà un'agenda di interventi per sostenere la crescita e lo sviluppo economico dell'Italia. il Governo è pronto a fare fino in fondo il suo dovere. Abbiamo la maggioranza parlamentare, una forte determinazione, abbiamo la piena consapevolezza delle responsabilità e dell'impegno che ci attendono e il desiderio profondo e sincero di consegnare agli italiani, fra due anni, un Paese più forte e più sicuro di sé. È una sfida difficile, ma gli italiani meritano che venga giocata fino in fondo con tutte le nostre forze, e siamo convinti che sapremo essere, tutti insieme, all'altezza di questa sfida. Vi ringrazio.

che, certo, se non arrivano a negare la crisi così difficile in cui si trovano la nostra economia ed il nostro Paese, la rendono quasi incredulo del perché essa stia accadendo. Non sono più i tempi in cui lei si arrabbiava molto con la Banca d'Italia, con i giornali, ovviamente con l'opposizione, perfino con Confindustria, quando la richiamava ad una iniziativa

E questo è un fatto positivo, Presidente. I fondamentali della nostra economia sono sani? Non tutti sono sani, signor Presidente. Non è un fondamentale della nostra economia la spaccatura drammatica tra Nord e Sud? È o non è un fondamentale dell'economia questa condizione gravissima per il nostro Paese? Ma è vero: alcune indicazioni lei le ha date e sono certamente in controtendenza rispetto alla crisi che il nostro Paese vive sui mercati. E non si chiede perché, signor Presidente? Questa condizione, se c'è, è dovuta ad un problema tutto politico, ad un problema di credibilità della *leadership* e di una condizione di debolezza di questo Governo, che non viene ritenuto all'altezza di questa sfida così complicata. Signor Presidente, i mercati non sono agenti impazziti. Non è il destino cinico e baro che si abbatte su questo Paese. Sono percorsi raffinati di interessi precisi. Se è vero che è sotto attacco l'euro, perché

Signor Presidente, noi siamo fuori dal gruppo dei Paesi fondatori. Francia e Germania fanno senza di noi. Siamo rimasti al traino di questi potenti Paesi europei di cui una volta eravamo *partner*. Signor Presidente, io non sono mai stato

hanno costruito programmi elettorali, hanno stretto alleanze, hanno condiviso anche responsabilità di governo. C'era infatti il convincimento che la sua *leadership* fosse capace di evocare energie positive per il Paese, fosse capace di una stagione di modernizzazione di stampo liberale, fosse capace di di modernizzare la nostra pubblica amministrazione, sapesse innescare dinamismo imprenditoriale nel sistema produttivo, sapesse anche affrontare il tema della coesione nazionale e quindi recuperare il divario drammatico che c'è tra Nord e Sud. Vede, signor Presidente, se queste alleanze, prima con l'UDC e poi con il Movimento per le Autonomie, sono venute meno non è perché noi abbiamo aderito alla stagione dell'antiberlusconismo: non partecipiamo a questa dialettica asfittica del nostro Paese in cui il bipolarismo è stato scandito tra berlusconiani e antiberlusconiani. Noi abbiamo cambiato opinione, abbiamo interrotto il rapporto di collaborazione perché abbiamo giudicato in modo insoddisfacente la situazione di governo, perché la stagione delle riforme, dell'innovazione, del cambiamento, della modernizzazione non è mai venuta. C'è un problema vero di guida politica di questo Paese. Presidente, lei è un imprenditore, è abituato a fare i bilanci (l'ha detto anche alla Camera), sta attento all'economia e alle aziende in Borsa: faccia un bilancio di questi dieci anni! È da dieci anni che lei governa questo Paese, tranne una breve interruzione infelice - glielo dico io - in cui la sinistra, tenuta insieme dal collante dell'antiberlusconismo, ha manifestato in pieno la sua incapacità di governo, restituendole la restituendole la responsabilità di guidare questo Paese. Ma dieci anni, signor Presidente, sono un tempo sufficiente per un bilancio in rosso: quello che oggi lei deve leggere è il bilancio in rosso della sua responsabilità di governo. Signor Presidente, lei ha chiamato in causa prima ancora il debito pubblico, e chi può negare che il debito pubblico sia un gravame pesantissimo sulle nostre spalle maturato in tempi andati? Ma lei sa, signor Presidente, che nel 2007 il debito pubblico in questo Paese era del 103 per cento rispetto al PIL e oggi è del 119 per cento rispetto al PIL: è cresciuto di 16 punti in tre anni.

delle Regioni, varate un primo spezzone di questo piano che consente investimenti infrastrutturali per circa 7 miliardi di euro. Signor Presidente, sì, oggi è così, ma è tanto tardi: tre anni sono passati perché questo piano, questa iniziativa, quest'azione di governo si sviluppasse nel Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è in una situazione di crisi drammatica. Io la invito - lei l'avrà fatto sicuramente - a leggere la brevissima sintesi all'anticipazione che la SVIMEZ ha fatto del rapporto

c'è un dato drammatico sugli investimenti in conto capi tale: meno 16 per cento nel Mezzogiorno, per la grandissima parte ascritti al mancato trasferimento di fondi FAS che sono stati per la maggior parte utilizzati in altre aree del Paese, quelli di competenza centrale. La metà di questi fondi di competenza delle amministrazioni dello Stato e del suo Governo, sia per la programmazione che per la spesa, sono andati altrove. Quelli di oggi sono soldi delle Regioni che parzialmente vengono loro affidati. Signor Presidente, c'è un altro dato. Ci dice la SVIMEZ che non basta l'investimento in infrastrutture: occorrono interventi, per esempio, sul tema della fiscalità, la famosa fiscalità di vantaggio che era lo strumento che avevamo concertato insieme per innescare un processo di sviluppo. Non si è mai vista la fiscalità di vantaggio, anzi abbiamo una riduzione drammatica di risorse in spesa sociale. Sa che è indispensabile un intervento sulla spesa sociale del Mezzogiorno, viste le condizioni drammatiche di marginalizzazione e povertà che si stanno consolidando in questa area del Paese? Perfino la politica di consolidamento del debito pubblico ci danneggia, e per una ragione molto semplice: dovendo rifinanziare i titoli del debito pubblico con gli interessi che crescono, tagliando spesa corrente, per la buona parte spesa sociale, si taglia un'altra linea di intervento nel Mezzogiorno, remunerando legittimamente i redditi e la forza economica dei detentori di questi titoli, che per la grandissima parte stanno nel Centro e nel Nord del Paese. È un dato oggettivo ed inevitabile, ma è un altro elemento di impoverimento drammatico del Mezzogiorno e delle sue famiglie rispetto invece invece al trasferimento automatico di risorse in altre aree del Paese, signor Ministro dell'economia. I nostri titoli del debito ci costano di più, i risparmiatori che li possiedono non stanno al Sud, qualcuno ci guadagna e qualcuno ci perde; il Sud ci perde sempre. Cosa le chiedo, allora, signor Presidente del Consiglio? Qui c'è bisogno di una grande svolta, di una grande politica e io credo che oggi questo bipolarismo malato - che ha visto lei come crinale di discernimento drammatico, perché ha dimostrato l'incapacità dell'intera politica di questo Paese di sapersi distinguere su grandi opzioni ideologiche, su grandi scelte di fondo delle politiche economiche,

che voi avete la responsabilità di governare perché è il Paese ad avervela affidata; giustissimo. Siete in condizione? Siete all'altezza di questa sfida? Queste giornate ci dicono di no. Il Paese rischia di finire in malora insieme a voi. voi. Credo che le sue rassicurazioni di stasera, i suoi toni calmi, la sua assicurazione che il Governo è in condizioni di reggere questa sfida, non tranquillizzeranno i mercati e nemmeno gli italiani, signor Presidente. C'è voluto il Capo dello Stato e un ruolo di supplenza istituzionale per consentire, in un momento drammatico, che la manovra finanziaria di due settimane fa fosse approvata, nella distinzione dei ruoli tra maggioranza e opposizione, in tempi celerissimi, ma quella manovra è stata quasi bruciata Possiamo chiedere al Capo dello Stato di intervenire, supplire ed assumere il tutoraggio di questo Governo? È quello da lei

del bipolarismo italiano che volge al declino, travolgendo il Paese. Credo, signor Presidente, che lei sia un uomo intelligente e che ami molte cose; se ama questo Paese, deve farsi da parte. finestra") *(CN-Io Sud-FS)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori del Governo, colleghi del Senato,

fosse il secondo tempo della responsabilità politica ed istituzionale manifestata in occasione dell'approvazione della manovra. Dico auspicavo perché non possiamo far finta che non ci sia stato il dibattito che si è svolto alla Camera dei deputati. Mi auguro che al Senato questo spirito si recuperi ancora e che questa sia per davvero l'occasione per affrontare con responsabilità istituzionale reciproca la sfida che abbiamo di fronte. Questo richiama, innanzitutto, alla responsabilità del Governo e della maggioranza e, da questo e, da questo punto di vista, signor Presidente, credo che lei possa fare un passo ulteriore in questa direzione. Credo che sia utile - e lo dico per schematizzare

questa occasione debba essere colta come primo momento dell'itinerario che domani vedrà il confronto con le parti sociali, per cercare molto schematicamente di raggiungere quelli che noi riteniamo siano i due grandi obiettivi di questa fase. di costruire un patto sociale per la crescita; dall'altra, di determinare un patto istituzionale per le riforme a partire da quelle costituzionali. Credo che, da questo punto di vista, un passaggio ulteriore di accento, di apertura politica ed istituzionale la maggioranza e il Governo possano e debbano fare, anche perché deve essere chiaro un dato politico,

di sciogliere un nodo di carattere politico fondamentale, ossia se costruire l'alternanza nella stabilità di Governo o se ricercare lo strappo, la rottura, la contrapposizione. Questo è il significato di un dibattito che si riduce in buona sostanza a recuperare le parole d'ordine della contrapposizione antiberlusconiana e antigovernativa, raggiungendo la semplificazione di dire: «Berlusconi ti devi dimettere». A che serviva il dibattito parlamentare se c'era soltanto la necessità di ribadire la richiesta di dimissioni del Governo?

Il Governo ha i suoi doveri. L'opposizione deve decidere se esiste ancora davvero lo spazio per costruire nella stabilità la prospettiva dell'alternanza, come dovrebbe essere in un bipolarismo maturo, capace di confrontarsi sul terreno della cultura di Governo e di animare la politica attraverso la contrapposizione delle proposte e delle visioni.

Al di là della demagogia o della verità, è questo il modo migliore per evitare che si continui a parlare del costo della politica. Bisogna tagliare sprechi. Bisogna eliminare privilegi. Ma un Paese che parla della politica come un costo e non come una risorsa è destinato al fallimento È la politica che significa tensione verso il bene comune. È la politica che significa servizio alla comunità. È la politica che può e deve significare perseguimento dell'interesse generale. contrario, vince non la democrazia ma la mercatocrazia, che è una via diversa. Essa espropria di sovranità gli Stati e determina una subalternità della politica ai poteri invisibili che ogni tanto si richiamano e non possono certamente essere richiamati

tra una democrazia, per quanto difficile da costruire nella sua capacità decidente, ed una sorta di subalternità a questa via mercatale, che non è la prospettiva che dobbiamo perseguire o subire.

come quella fondamentale della crescita del Paese, a partire dallo sviluppo del Mezzogiorno. Però, un passo avanti significativo è stato fatto. Va dato atto al ministro Fitto, va dato atto al ministro Tremonti, va dato atto al Governo di avere determinato questa possibilità, questa potenzialità.

tutta con grande onestà intellettuale - in modo tale da dare un segnale positivo in questa direzione. E così bisogna continuare, da questo punto di vista. Allora qui, per sintesi e brevità (perché vedo che la collega mi segna il tempo, il tempo della crisi e anche il tempo dell'intervento dentro la crisi) dentro questa riflessione, di breve momento ancora, io vorrei recuperare una riflessione alla quale lei ha accennato, Presidente: un grande Paese si costruisce anche attraverso la capacità di tutti gli attori istituzionali, economici e sociali di fare la propria parte. E lei ha fatto riferimento allo Statuto dei lavoratori e alla cassa integrazione. Mi consentirà di recuperare, e mi consentirà in particolare di farlo il ministro Sacconi, in maniera organica questa prospettiva. E questa prospettiva in maniera organica si recupera riprendendo l'itinerario riformista e riformatore, a partire dal Libro bianco sul mercato del lavoro di Marco Biagi. Lungo quell'itinerario c'è un programma di Governo ancora inesplorato, che ci consente anche di affrontare il tempo della crisi, non solo con le politiche passive, ma con le politiche attive del lavoro, sciogliendo i nodi del grande cambiamento e della modernizzazione del mercato del lavoro nella comparazione con i sistemi europei, e continuando lungo quel tragitto che non era fatto di precarietà, ma di sussidiarietà e di grande volontà di costruire un Paese moderno, capace di sciogliere e di attuare oggi il nodo della partecipazione e della

lei dice: il Governo governi. Ma recuperi la voglia, la volontà, la determinazione per governare nel tempo della crisi, con la prospettiva del grande cambiamento, non del conservatorismo pigro, non del continuismo inutile, ma con la grande volontà di modernizzare Il centrodestra vince se governa il cambiamento, non se si ferma alla bega politica che non risolve i problemi e non rende il servizio al Paese.

Signor Presidente, che cosa non tornava nel discorso del Presidente del Consiglio? Perché il discorso del Presidente del Consiglio è suonato

ma dava mostra di crederci. Oggi non ha detto la verità, e neanche ha dato mostra di crederci. Io ricordo, colleghi senatori, che non un secolo fa, ma appena sei settimane fa, il 21 giugno, il Presidente del Consiglio è venuto nell'Aula al Senato non un secolo fa, ha detto: "Rivendico come un risultato formidabile del nostro Governo il fatto di avere messo al riparo il debito pubblico italiano dagli attacchi speculativi". Non un secolo fa, ma sei settimane fa, ha detto: "eviteremo certamente di finire come altri Paesi europei che si stanno dissanguando per sopravvivere". Non un secolo fa, ma poco più di un mese fa ha detto «C'è stato il rischio di essere travolti dalla crisi e c'è stata la concreta possibilità di subire passivamente tutti gli effetti negativi della speculazione finanziaria internazionale. E invece no». Queste sono le parole del Presidente del Consiglio che non dice la verità, ma prova a presentare agli italiani la sua idea di un Paese che va meglio. Perché oggi non è credibile il Presidente del Consiglio che non dice la verità e indora una pillola che gli italiani che ci ascoltano da casa sanno essere tutt'altro che dolce, perché la situazione è dura per le famiglie, è dura per le imprese, è dura per il Nord e per il Mezzogiorno? Cosa è che non funziona, colleghi? Prenderò meno di un minuto per darvi dei dati, perché il punto politico è uno solo, Presidente: se la crisi internazionale è grave - ed è grave - la crisi italiana è peggiore. Quindi tutto l'assunto del Governo, per cui noi ce la stiamo cavando persino meglio degli altri,

e confrontiamoli non con Paesi lontani, con gli altri tre grandi Paesi dell'area dell'euro, la Spagna, che stava peggio di noi, la Francia e la Germania. Chi il 21 giugno aveva risparmi in borsa, da allora in Italia ha perso più del 14 per la borsa spagnola, cioè quella di un Paese molto più in crisi di noi allora, ha perso in quello stesso periodo, in questo mese e poco più, il 9 quella francese il 5,8 (molto meno della metà di Milano); quella tedesca appena il 3,3 per cento. Il Governo spagnolo, nel frattempo, ha dichiarato il suo fallimento, si è dimesso e ha chiamato le elezioni politiche. I nostri buoni del tesoro decennali, ecco quello che interessa agli italiani, ai risparmiatori, alle famiglie che vogliono sapere cosa fare con i 50.000 euro che

I buoni del Tesoro italiani hanno superato il 27 giugno la barriera del 5 per cento del rendimento, oggi sono ad un livello del 6,27, pari a quello del 1990: siamo tornati nella crisi più profonda della finanza e dell'economia italiana. Lei le ha dette queste cose, signor Presidente del Consiglio? Lei ha fatto il quadro della verità dei numeri drammatici e autentici della crisi economica? Il differenziale con i titoli tedeschi quel giorno, quando lei ha parlato e ha fatto quelle affermazioni, era pari a 184 punti; ieri era più che raddoppiato, in poco più di un mese: 369 punti. Intanto, quello spagnolo lo abbiamo praticamente raggiunto, mentre allora sembrava lontanissimo; quello francese è appena a 60 punti ed i titoli tedeschi oggi sono a un rendimento eccezionale del 2,4 per cento. Presidente, sono numeri aridi, sono numeri vuoti o è un punto di verità che chi guarda certi telegiornali, quelli del «tutto va bene, madama la marchesa», assomiglianti al suo discorso di stasera, non può sentirsi dire? Sono numeri aridi o è la realtà di un Paese che sta peggio degli altri Paesi che stanno dentro, come tutti i Paesi stanno dentro, la crisi economica? E allora il punto politico, è il punto di una crisi di fiducia. Crisi di fiducia dei mercati internazionali verso il vostro Governo; crisi di fiducia che traduce la situazione italiana in meno ricchezza, meno lavoro e più indebitamento per tutti gli italiani. Ed è una crisi di fiducia che ha radici e ragioni politiche. La prima: avete sopperito alla crisi della maggioranza elettorale dopo la fuoriuscita, la cacciata del presidente Fini, con un drappello di deputati disponibili, ma con un nuovo equilibrio politico, immaginato sul PdL e Berlusconi, sulla Lega, su Tremonti. Tutti e tre questi pilastri, tutte e tre queste gambe della politica del Governo sono in crisi, tutte e tre insieme, e tutte e tre tra di loro, se abbiamo ascoltato il discorso della Lega poco fa a Montecitorio: discorso di opposizione quasi più forte di alcuni dei partiti di opposizione. Scontento, frustrazione, insoddisfazione profonda nella vostra maggioranza; la crisi del ministro Tremonti; la sfiducia tra voi, che non vi parlate. I mercati internazionali lo capiscono che questa è una maggioranza divisa al suo interno, fratturata al suo interno, sfiduciata innanzi tutto al proprio interno. E la seconda motivazione non è solo politica, ma è propriamente economica. Voi avete approvato una manovra, il cui traguardo politico non è il 2011, non è il 2012, ma il 2013 e il 2014. E quali sono i mercati che, in una condizione di fragilità politica come quella nella quale si trova il vostro Governo, sono pronti ad investire sull'Italia? coloro che hanno dei risparmi da gestire, sapendo che questo Governo è così debole politicamente e domani è destinato a cedere il passo, dopo le elezioni politiche, ad un altro Governo, che è quello che dovrà realizzare la manovra che oggi voi avete approvato, ma che non entra in vigore oggi? Ma non è questa, Presidente e colleghi, la ragione per la quale, anziché investire sull'Italia, si disinveste dall'Italia? Si portano via le risorse, si danneggiano i risparmi degli italiani, si mette in crisi la nostra economia. Ed allora, Presidente e colleghi, è evidente che oggi lei ci ha richiamato ad uno spirito patriottico abbiamo già dato prova con tutte le opposizioni. L'Italia, unico Paese democratico, ha votato in tre giorni una manovra che, pur non avendola condivisa, abbiamo consentito venisse varata di fronte all'emergenza economica, finanziaria e sociale che si profilava.

PD e della Lega, la proposta più seria e più urgente, la riforma della Costituzione che impone il pareggio di bilancio. È la scelta già approvata dalla Germania, in via di approvazione in Francia, su cui dovete solo dire di sì. Noi siamo pronti a riunirci da domani in Commissione, presidente Schifani, per approvarla nel giro di poche settimane. Voi siete pronti a farlo? Vi sfidiamo a farlo. Questo sarebbe il messaggio di volontà, di serietà e di credibilità che i risparmiatori e gli investitori si aspettano. Noi siamo pronti, colleghi, non solo a concordare con le parti sociali, così come ha proposto il presidente Casini, una commissione per convergere sulle riforme per la produttività, per le liberalizzazioni, per l'innovazione, per la crescita, ma a portare in Parlamento già a settembre una manovra che anticipi gli effetti fondamentali di quella troppo lontana che avete approvato.

perché dobbiamo dare questo messaggio agli italiani. Sono numeri piccoli ma numeri che contano. E noi siamo qui per dirvi che il Terzo Polo che è nato, il nuovo Polo che unisce le forze di Alleanza per l'Italia, di Futuro e Libertà. Dell'UDC,

non aspettiamo la spallata dei mercati. Vi diciamo che ci vuole un Governo di larga convergenza, con un Premier che faccia un passo indietro. Dubitiamo che lo faccia, ma siamo pronti ad appoggiare un Governo che proponga al nostro Paese la soluzione difficile ed indispensabile per tornare alla crescita, al lavoro, al futuro dei giovani. Siamo pronti a farlo insieme. L'Italia ce lo chiede e se voi direte di no ne pagherete il prezzo, per gli anni a venire e davanti al popolo italiano. senatore Belisario. Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio, colleghi, il presidente del Consiglio Berlusconi è venuto a parlare in Senato in quattro circostanze: - non poteva farne a meno - e ha parlato di quello che doveva essere il suo programma di Governo; per due anni e mezzo ha evitato di frequentare l'Aula del Senato ed è ritornato nel settembre del per dirci che all'interno del suo partito era avvenuta una scissione; poi è tornato ancora il 13 dicembre 2010 parlando del nuovo assetto di Governo e, infine, il 21 scorso è ritornato su indicazione e monito del Capo dello Stato. Ecco che quando ha deciso e comunicato di venire

che lei venisse a fare un appello al Paese dicendo: «Cari italiani, io e il mio Governo abbiamo sbagliato l'approccio alla crisi, l'abbiamo negata perché siamo degli inguaribili ottimisti e degli inossidabili narcisisti, ma siamo qui a chiedervi scusa per quanto abbiamo fatto o non abbiamo fatto finora e vi chiediamo aiuto perché l'Italia è un grande Paese, un grande Paese in difficoltà, e tutti dobbiamo lavorare per riportarlo dove merita di stare». Invece niente di tutto ciò, solo la descrizione di uno scenario di cui lei è un abile regista, un regista di *soap opera*, uno scenario interno che non risponde né a verità, né a realtà.

signor Presidente del Consiglio, il problema non è dare certezze ai mercati e non credo che l'intervento che lei ha fatto oggi le dia. Forse, è anche quello di dare certezza ai mercati, ma va restituita certezza agli italiani che chiedono serenità e fiducia, e la vogliono dal Governo, dal Parlamento, da una classe «Il peggio è passato.» - ha detto il 5 marzo 2009 - «I problemi sono alle spalle. Non credete ai giornali pessimisti». Non contento, ribadiva il 17 maggio 2009, che «Il momento peggiore è passato e d'ora in poi ci saranno miglioramenti. C'è stato un diluvio universale, ma noi siamo qui e siamo meglio di prima. Il Governo ha fatto bene a diffondere fiducia». «Non abbiamo peccato di ottimismo» - continua nel luglio 2009 - «perché questa crisi, è stato dimostrato, ha solo origine psicologica». ancora che tutto era cambiato e che non dovevamo temere nulla, come un mantra, una litania di bugie che ha continuato a raccontare fino a pochi giorni fa, quando ha sostenuto che l'Italia ha superato una crisi internazionale Grazie. Presidente, a me spiace, ma devo dire che il suo discorso è stato opaco e pieno di contraddizioni: nessuna misura concreta annunciata e nessun dettaglio nell'agenda per il suo confronto con le parti sociali; nessun riferimento all'economia reale. Ma lei ha voluto dare i numeri e allora leggiamoli insieme i suoi numeri: 27 misure concrete; 15 provvedimenti per la crisi economica; 3 leggi finanziarie, più 2 collegati; rappresentavano o avrebbero dovuto rappresentare provvedimenti urgenti per far fronte alla crisi con manovre di finanza pubblica. Purtroppo, però, il fallimento è davanti agli occhi di tutti: i nostri conti sono in difficoltà, e vorrei ricordare che 500 miliardi di euro di debito pubblico li ha fatti lei nei periodi in cui è stato Presidente del Consiglio. *IdV)*. Li conti i numeri; lei è un po' distratto, Presidente. Non sono serviti quaranta mesi di Governo per portare l'Italia fuori dalla crisi e soprattutto per rilanciare la nostra economia e far crescere competitività in un Paese che è sprofondato in una crisi sempre più profonda, che ha lacerato le famiglie, i lavoratori e le imprese, oltre a produrre un aggravamento conclamato della pressione fiscale. In venti mesi, collega Nespoli, dovremmo fare il giro del mondo, la rivoluzione della Costituzione, il cambiamento delle norme sul lavoro, la riforma fiscale;

sono quelle per sostenere l'efficienza della giustizia. Ma sa, tra prescrizione breve e processo lungo, lei e il suo *staff* di Ministri e avvocati siete andati in evidente confusione. Ha detto che l'Italia ha i fondamentali a posto, che non bisogna inseguire i nervosismi del mercato, ma poi, evidentemente timoroso, ha atteso che i mercati chiudessero per rompere il suo lungo silenzio e per parlare finalmente di una crisi che ha nascosto, ma che poi è venuta purtroppo brutalmente a galla.

questioni di fiducia, signor Presidente del Consiglio, dopo le 48 che ha già chiesto, intende porre al Parlamento? Come possiamo aiutarla a risolvere i problemi se lei per mestiere sbatte La coesione nazionale cui il Capo dello Stato fa riferimento cui il Capo dello Stato fa riferimento è una cosa seria, ma questo non significa fare coesione nazionale per essere conclamatamente dichiarati fessi. Noi vogliamo servire il Paese e lo vogliamo fare con amore. Se non vi rendete conto che state sfasciando il Paese, purtroppo non abbiamo i numeri per impedirlo in Parlamento. Ma proprio oggi lei, che si affida ai sondaggi e che è il più amato dagli italiani, ha appena il 23 per cento dei consensi degli italiani: ha appena qualche punto percentuale in più di Zapatero, che ha avuto il coraggio di rassegnare le dimissioni e di portare il Paese al voto. Signor Presidente del Consiglio, glielo dico con l'amore che ho per il mio Paese, con l'amore che dobbiamo avere tutti in questo momento. Nel momento in cui i dati sono questi sono questi e il Paese le chiede di fare un passo indietro, noi glielo diciamo veramente con grande serenità: faccia un passo indietro, dimostri di voler bene a questo Paese, non rimanga abbarbicato come l'edera alla sua poltrona. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi senatori, se siamo qui e se lei è qui, signor Presidente, è perché l'Italia corre rischi che non hanno precedenti nella storia del dopoguerra. Alcune delle ragioni le ha dette lei, e sono vere: la crisi finanziaria internazionale, le speculazioni sui titoli del debito pubblico di singoli Stati membri dell'Unione europea la crisi di fiducia nei confronti dell'euro anche in ragione della fragilità istituzionale dell'Europa. Tutte queste ragioni certamente non sono imputabili a lei. Queste ragioni, però, non sono le uniche. Vi sono infatti ragioni interne al nostro Paese: ragioni profonde che devono essere analizzate e che dovrebbero indurci ad una seria e impietosa autocritica. Non è possibile, infatti, che un Paese come il nostro possa sostenere un debito pubblico pari al 120 per cento del prodotto interno lordo, senza che la nostra economia cresca. Tra il 2001 e il 2007, infatti, con tassi di interesse bassi, il peso del nostro debito è cresciuto. Non oso pensare cosa succede quando si alzano i tassi di interesse. È vero - infatti - che l'Italia è stato uno dei Paesi più virtuosi durante l'ultima crisi, ma è altrettanto vero che il nostro non è un problema di deficit pubblico, ma di debito e di e di crescita. Se il nostro deficit è superiore al tasso di crescita della nostra economia, il peso del debito salirà, anziché scendere. Se la malattia principale dell'Italia è - quindi - la bassa crescita, occorrono interventi straordinari ed urgenti per invertire il ciclo economico negativo: interventi urgenti ed efficaci, come auspicato e proposto dalle parti sociali nel Patto per la crescita e, nei suoi autorevoli e reiterati appelli, dal Capo dello Stato. Signor Presidente, il Governo deve agire velocemente su due piani: l'adozione di misure di forte aggiustamento dei conti pubblici, accorciando l'orizzonte temporale che si era dato (il 2014), e definire tempi certi e rapidi di un'agenda, condivisa con le parti sociali e con le opposizioni, di riforme strutturali indispensabili per la crescita. Occorrono, infatti, significativi tagli alla spesa pubblica che siano però funzionali alla crescita: tagli selettivi e non più lineari. Se i tagli non innescano un circuito virtuoso di ripresa, si rischia di sottrarre ossigeno all'economia italiana almeno per 2 punti di prodotto interno lordo in tre anni; cosa che non ci possiamo permettere. È infatti vero che dobbiamo recuperare i notevoli ritardi che abbiamo accumulato su questo fronte: da quando, dopo la crisi, è ripartita anche l'economia italiana, essa ha recuperato solo 2 dei 7 punti di PIL persi durante la crisi. Pensiamo solo al fatto che noi, che siamo molto simili alla Francia, negli ultimi 10 anni siamo cresciuti solo del 3 per cento, a fronte del 12 per cento di crescita dei francesi. Bisogna affrontare subito la nostra crisi strutturale di produttività, che riguarda tanto il Nord, quanto il Sud dell'Italia. La crisi di produttività incide profondamente e negativamente sulla crescita e sulla competitività, apre disavanzi crescenti nella bilancia dei pagamenti e inaridisce l'afflusso di investimenti diretti. *(Brusìo).*

Posso chiedervi di raggiungere i vostri posti, se possibile? Grazie. Grazie, signor Presidente. Tutto ciò - dicevo - causa il calo delle retribuzioni e dei salari ed i consumi reali delle famiglie se crescono (e non crescono) - anche quelli vostri, cari colleghi della Lega lo fanno comunque in danno esclusivo del risparmio. È vero, come dice lei signor Presidente, che l'accordo anti *default* americano, pur essendo un fatto positivo non fuga i timori in ordine al deficit federale e alla crescita economica. Tutto ciò ha inevitabili ripercussioni anche sulla nostra economia; ripercussioni delle quali dobbiamo tener conto. Per farlo occorre agire in fretta e occorre agire drasticamente sul nostro debito pubblico, che è la più grande e devastante tassa occulta che pagano tutte le famiglie italiane, quelle che se lo possono permettere e, soprattutto, quelle che non se lo possono permettere. Come lei sa, signor Presidente del Consiglio, e come sanno tutti gli italiani le opposizioni hanno mostrato e continuano a mostrare grande senso di responsabilità, ma tutto questo non basta se non c'è da parte sua e della sua maggioranza una reale volontà di collaborazione e cioè l'assunzione piena di responsabilità che si tramuta in scelte coerenti e, soprattutto, immediate, perché è chiaro che un'altra parola magica in questo momento è credibilità del Governo. Alcuni autorevoli commentatori hanno sottolineato oggi che l'Italia non merita la sfiducia dei mercati, visto che le famiglie italiane lavorano e risparmiano più della media europea e che le imprese italiane esportano tanto quanto le imprese tedesche. È vero, è profondamente vero e giusto. Aggiungiamo noi che non se lo meritano i giovani italiani, il cui tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni raggiunge il 28 per cento; non se lo meritano, in particolare, i giovani del Sud, il cui tasso di disoccupazione è arrivato al 39 non lo merita il Mezzogiorno intero, signor Presidente del Consiglio, perché la crisi ha mostrato i suoi effetti più pesanti proprio lì. Il Sud ha subito una caduta maggiore del PIL ed una riduzione ancora più pesante dell'occupazione. Per questo non è sufficiente lo sblocco in ritardo di 7 miliardi di euro dei fondi FAS operato oggi dal CIPE, almeno per due ragioni: perché sono risorse dovute da tempo (almeno da tre anni) per interventi in parte già avviati e non sono risorse aggiuntive; perché non bastano a rimettere in moto l'economia del Sud. Le segnalo, signor Presidente del Consiglio, che tra i progetti finanziati oggi dal CIPE mancano quelli che riguardano la ricostruzione di Giampilieri e Scaletta colpiti due anni fa dalla frana che ha fatto 33 morti e su cui lei si era impegnato personalmente. Serve un piano vero per il Mezzogiorno che abbandoni la logica immaginifica di pseudo-grandi interventi e rimetta in movimento opere e infrastrutture, cantierate o immediatamente cantierabili. Su questa strada, purtroppo, siamo ancora all'inizio. Serve una misura forte dal carattere oggettivamente compensativo come la fiscalità di vantaggio, anche e soprattutto per recuperare i tagli consistenti e devastanti che, purtroppo, il suo Governo ha fatto in questi tre anni agli investimenti per il Mezzogiorno. Ci vuole un piano vero, concreto, immediato che concentri tutti gli investimenti pubblici e privati su infrastrutture sovraregionali energia, logistica, capitale umano e innovazione. Mi consentirà di dire, signor Presidente del Consiglio, che la sfiducia dei mercati se la merita, in parte, la politica, quando essa non compie scelte chiare e coerenti. Pensiamo ai *ticket* nella sanità: una misura controversa certamente, iniqua sicuramente, ma ormai decisa e applicata dal Governo. Ciononostante, questa misura continua ad essere contestata all'interno della sua maggioranza dalla Lega e da alcune Regioni che non intendono applicarla aggravando i loro bilanci. Ma quale credibilità può avere un Paese che si comporta così? È ora di andare oltre e di essere seri fino in fondo, costi quello che costi. Signor Presidente, glielo ha già detto alla Camera dei deputati il nostro leader*,* l'onorevole Pier Ferdinando Casini, glielo ribadiamo noi qui, perché *repetita iuvant*. Occorrono provvedimenti urgenti, occorrono ora uno o più decreti-leggi che si occupino di questi problemi: tagliare selettivamente la spesa pubblica per ridurre fortemente il debito pubblico e anticipare il pareggio di bilancio. Chiedere sacrifici agli italiani è difficile, ma occorre farlo, e occorre farlo partendo da chi ha più risorse economiche e patrimoniali a disposizione. Sì, onorevoli colleghi della Lega Nord, perché purtroppo le tasse in questi anni le avete aumentate voi e nel modo peggiore possibile, caricandole solo sul ceto medio e sulle fasce più deboli. Bisogna fare subito quelle liberalizzazioni e quelle privatizzazioni che servono a disincagliare la nostra economia dai vincoli e dagli impedimenti che la rendono pesante, impedendole di crescere. Altro che riforma dell'articolo 41 della Costituzione! Basta una norma ordinaria sulle liberalizzazioni da fare subito, ma che voi non avete fatto, impedendo al ministro Tremonti di presentarla nella manovra economica, forse per paura o per incapacità. Bisogna subito mettere al centro del nostro lavoro parlamentare la riduzione delle tasse sul lavoro e sulle imprese e l'anticipo degli effetti dell'innalzamento dell'età pensionabile. modo bisogna sostenere l'iniziativa del Governo sugli eurobond. In poche parole, signor Presidente del Consiglio, occorre mettere in campo una politica di austerità a lungo termine, a cominciare dagli usi e dai costumi della politica, che ha bisogno del concorso di tutti, della maggioranza e dell'opposizione, che ha bisogno di un Governo forte e determinato nelle scelte, che sappia parlare agli italiani il linguaggio della verità, convincendoli della bontà delle scelte da fare, anche di quelle più impopolari, perché servono al futuro dei nostri figli. Subito, signor Presidente del abbia il coraggio di dirlo, abbia e il coraggio di farlo; ne va dell'Italia. Se vuole ancora guidare questo Paese, non ha altro da fare e lo deve fare ora, sapendo che potrà contare sulla collaborazione parlamentare delle opposizioni; se farà cose serie, come sempre abbiamo fatto, ci troverà qui in Parlamento a collaborare. Ci sembra difficile, in verità, per le cose che dice e le cose che fa. Noi comunque siamo qui, sereni e determinati a lavorare per il bene del Paese.

Due parole chiave emergono però con forza: *rating* e Germania; un altro modo di dire rigore e crescita. Per *rating* si intende valutazione della credibilità del nostro sistema Paese,

*Rating* per le imprese significa finanziamenti da parte delle banche; le nostre imprese sono penalizzate perché le tasse alte complicano la valutazione del *rating*, il quale si calcola dopo le tasse e anche dopo l'IRAP, che si paga anche se si è in perdita.

*Rating* e valutazioni anche della politica, di tutta la classe dirigente, giornali compresi. Non va disperso, secondo noi, il clima di coesione e di collaborazione che ci ha permesso in soli tre giorni di approvare una manovra imponente.

e si crea così ulteriore incertezza sui mercati, ma semplicemente non è così. È bella la tabella che è stata pubblicata sul sito www.lavoce.info, che non è certo vicino al Governo: considerando tutti gli interventi economici del Governo dal 2010 al 2014, 192 miliardi di euro, la metà sono nel primo trimestre e l'altra metà nel secondo trimestre; si tratta cioè

Possiamo crescere come la Germania? Questa è la domanda vera. Per il Nord, che cresce a ritmi simili a quelli tedeschi, la sfida è nota e fattibile. La mia Lombardia, in testa per le esportazioni verso l'Europa, ha incrementato del 25 per cento le esportazioni proprio verso la Germania. Il punto è un altro. Può tutto il Paese copiare il modello Germania, visto che ormai i modelli anglosassoni non sono più di moda e sono da scartare? Vediamo allora quali sono i punti di forza del modello Germania e le nostre azioni di politica economica per avvicinarci a quel modello. Il primo punto di forza dei tedeschi: il sistema manifatturiero. Certo, noi non abbiamo i grandi gruppi tedeschi, ma abbiamo una rete di piccole e medie imprese superefficienti e abbiamo il *design*. Dobbiamo insistere nel sostegno alle reti d'impresa, ai confidi, al *design*, alle tipicità dell'agroalimentare; battaglie storiche della Lega Nord. Il secondo punto di forza dei tedeschi: una cultura tecnica molto avanzata. In quest'ottica va benissimo la riforma dell'apprendistato. Dobbiamo però recuperare posizioni nella qualità dell'insegnamento, soprattutto per le materie scientifiche, e raggiungere tutti, tutte le Regioni, le eccellenze del Friuli e del Nord Est in genere. Il terzo punto di forza dei tedeschi: relazioni sindacali improntate alla collaborazione e non al conflitto. Ci aspettiamo molto in tal senso dal confronto Governo e parti sociali che ci sarà nei prossimi giorni ci aspettiamo molto dallo sviluppo della contrattazione territoriale, altro pallino e battaglia storica della Lega Nord. Infine, l'ultimo punto di forza della Germania: l'efficienza del sistema istituzionale. Si è parlato molto in questi giorni di costi della politica e di efficienza del sistema politico, di tempi di apertura del Parlamento, di tempi di risposta del Parlamento. Ebbene, la Germania è uno Stato federale e non ha il bicameralismo perfetto. La riforma è approvata dal Governo. È già sul tavolo. La Lega è pronta. Apriamo il confronto e approviamola in fretta. La riforma è semplice: metà parlamentari e tempi di risposta europei, con la fine del bicameralismo perfetto; risparmio ed efficienza, ancora le due parole di cui si diceva prima; il *rating* e la Germania; uno Stato snello ed efficiente. Questa è la ricetta della Lega Nord da sempre.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, la serietà della situazione del Paese, la sua gravità, mi obbliga, in realtà ci obbliga, a lasciare ogni tono comiziale ma anche a chiarire bene agli italiani quale sia il senso di questa lunga giornata in Parlamento e a trarne (se riusciremo a farlo) una ragione di utilità per il Paese. Il collega Alfano alla Camera ha rivendicato che lei sia venuto per libera scelta e in nome del Paese qui in Parlamento. lei è qua, presidente Berlusconi, perché noi abbiamo richiesto la sua presenza, allarmati dall'assenza politica del Capo del Governo in un momento così difficile per il Paese per la condizione della sua economia reale, proprio la condizione di quelle imprese e di quelle famiglie a cui lei fa costantemente riferimento, per la speculazione sui nostri titoli, per l'andamento della borsa, per la crisi di fiducia che investe il suo Governo e che è l'oggetto - perché è questo e non altro - dell'appello congiunto di tutte le forze economiche e sociali, esclusa la UIL. L'oggetto di quell'appello è questo: la sfiducia nel suo Governo. La lettura di questi elementi in realtà ci dice da una parte che c'è una drammatica crisi di fiducia nel Paese (non avremmo altrimenti il turbamento sui mercati finanziari e quello che investe i nostri titoli); dall'altra che c'è una drammatica crisi di fiducia del mondo produttivo nei confronti del suo Governo e della sua politica. E io di questo parlo. Non parlo della crisi di fiducia squisitamente politica che potrei derivare - e potrei farlo in maniera maniera assai credibile - dai dati elettorali o dai dati referendari: io mi riferisco alla crisi di fiducia nella sua politica economica che viene dal mondo dell'impresa e dal mondo del lavoro. Ciascuno di noi ha letto quel comunicato, quindi io non ho bisogno di fare Maramaldo; e ciascuno di noi - e questo è un punto sul quale riflettere - sa bene che esso è intervenuto dopo l'approvazione della manovra finanziaria, a riprova di essere critico a quella manovra finanziaria nella quale non c'è elemento di crescita. Lei oggi ha elencato è ovvio che ciascuno promuove il suo prodotto - le norme per la crescita di quella manovra. Il primo banco di prova è venuto dall'appello congiunto delle forze produttive e delle forze del lavoro. Peraltro è una manovra finanziaria che - me lo lasci dire - ha avuto l'approvazione più tempestiva della storia repubblicana per merito delle opposizioni, che hanno loro richiesto al presidente Schifani l'immediata convocazione della Conferenza dei Capigruppo e quindi dell'Aula, e che hanno fatto in qualche modo - me lo lasci dire - supplenza rispetto alla sua assenza e all'incertezza della maggioranza nel momento in cui il nostro Paese era nella bufera dei mercati finanziari. Lei oggi rivolge un invito tiepido - e mi lasci dire che a me pare assai poco convinto e anche insincero alle opposizioni a fare proposte; è un invito che interviene quando si è fatto troppo tardi, troppo poco e troppo male; ma soprattutto nel momento in cui il troppo tardi, troppo poco e troppo male si è fatto perché mai si sono volute ascoltare le opposizioni anni le chiedono di prendere in considerazione le nostre proposte. Ora io non vorrei deluderla, ma temo che domani l'incontro con le forze economiche e produttive non andrà bene se la dote del suo Governo è quella che oggi ha esposto nel suo discorso perché è la descrizione stessa dell'Italia che lei ne fa che non corrisponde né a quella che noi facciamo da tre anni, ne a quella che fanno in quell'appello. Vorrei essere chiara, io non voglio essere offensiva, ma l'ho sentito il suo discorso, soprattutto la prima parte, l'affresco dell'Italia che lei ha disegnato. Dovrebbe derivarne che c'è un complotto plutocratico nei confronti dell'Italia, ma non c'è; e mi permetta anche di dire che il suo accenno al debito pubblico, che è vero che è uno degli elementi di fragilità strutturale del nostro Paese, non era però veritiero; i dati sono quelli della Banca d'Italia e sono consultabili da tutti: quando le abbiamo consegnato il Paese nel 2001, quando lei ha vinto le elezioni in

quello di pensare che poteva eludersi il tema della crisi, che era meglio presentare questo Governo come il Governo ottimista di un Paese in cui tutto va bene, di negare i segnali sempre più evidenti e profondi che vi venivano non solo dall'osservazione della realtà ma dall'incalzare delle opposizioni accusate di pessimismo e di malevolenza nei confronti del Governo; e il risultato è che siete arrivati tardi, troppo tardi, e a quel punto la strada dei tagli lineari senza strategia per il Paese e per il suo sviluppo era inevitabile. Se oggi finalmente la parola «crescita» entra nel vostro vocabolario (da tre anni invochiamo il Presidente della Repubblica, con quale vigore in questi ultimi giorni ancora), diciamo che alla parola «crescita» che voi usate non corrisponde però l'essenza della proposta e della concretezza della proposta per la crescita. Ad esempio, circa il Piano per il Sud di cui lei parla (diciamolo), 5,5 miliardi vengono da programmi regionali (lo dico ai colleghi della Lega), un miliardo e 800 milioni sono prelevati dagli investimenti per energie rinnovabili, attrattori culturali e obiettivi di servizi. Complessivamente, Presidente, la sua proposta è assolutamente al di sotto delle necessità del Paese. Voglio essere chiara, perché non ci siano infingimenti tra di noi: noi riteniamo che il pareggio di bilancio debba un obiettivo da raggiungere; ed è quella di avere proposte che la inneschino per davvero. Tante volte si è parlato delle nostre proposte: gliene faccio ora qualcuna. Potrei elencarle una doviziosa serie di proposte di legge. Se lei avesse la cortesia di andare a vedere le molte proposte che, in occasione della discussione dei moltissimi provvedimenti economici da lei proposti, abbiamo fatto, probabilmente si convincerebbe che questa opposizione qualche idea buona l'aveva, continua ad averla e potrebbe essere utile ascoltarla non con degnazione, ma con la responsabilità di chi capisce che la situazione è assai difficile e bisogna porvi rimedio. Mi riferisco al piano delle liberalizzazioni, a cominciare dal settore dell'energia, all'aumento della tassazione delle rendite, ai debiti della pubblica amministrazione, alla possibilità di di dare fiato ad una rete economica e produttiva, alla revisione del Patto di stabilità interno, al sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, (non con quella norma che avete messo in manovra finanziaria, che ha fatto - come dire? - inorridire tutto il mondo produttivo, come domani - immagino - vi che sia immaginato per rimettere in piedi il Paese (e, senatore Garavaglia, io la stimo molto, ma credo che la delega che il Governo propone sia una delega che aumenta le tasse e che non dà respiro al Paese). In assenza di politiche vere, concrete, tempestive - dovrei dire da ieri e non da oggi - purtroppo farà premio altro: farà premio il fatto che il nostro Paese sta perdendo 4 4 miliardi del quadro strategico nazionale 2007‑2013, che per un anno lei non ha nominato il Ministro dello sviluppo economico e per un anno non abbiamo avuto voce in Europa. Potrei dire ancora altro, ma voglio chiudere, Presidente. Sono queste le ragioni per le quali il nostro Paese in una crisi generale, certo,

E non possiamo più fare finta di non capire, lei per primo, Presidente, non può più fare finta di non capire, perché non è solo peggio per voi, è peggio per il Paese ed è comunque da irresponsabili. È per questo che noi siamo preoccupati e per questo abbiamo chiesto le sue dimissioni. Per questo noi crediamo che lei sia un intralcio; per questo invochiamo discontinuità.

c'è però in questo Paese una grande forza, un'energia, che è quella che ha mosso quelle forze a mettersi insieme e a stilare quell'appello congiunto che dà oggi forza alle nostre esportazioni, che è capace di produrre genio genio nella produzione e nella collocazione dei nostri prodotti. Il Paese, nonostante tutto, è in grado di farcela, però ha bisogno di guida ed ha anche bisogno di verità; lo dice il presidente Napolitano e noi davvero lo crediamo.

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, troviamo a discutere in Parlamento per negare la crisi economica, ma per combatterla e mettere a punto ulteriori proposte. Voglio partire proprio sottolineando la positività dell'intervento del presidente Berlusconi alla Camera e al Senato. Qualcuno si interrogava se questo dibattito poteva portare soluzioni salvifiche o se fosse utile o addirittura pericoloso. È bene che il Governo ci sia stato, che abbia messo la sua faccia, le sue parole per dare un segnale di impegno del Paese sui mercati interni e internazionali. Non fuggiamo dai problemi ma li affrontiamo, anche nelle sedi europee, presidente Finocchiaro, dove per primo il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'economia e tutti i rappresentanti del Governo sono stati protagonisti di molti fatti. oggi la Commissione europea ha giudicato positivamente la nostra manovra, le nostre misure. Il commissario Olli Rehn ha espresso parole di apprezzamento. Non voglio riassumere nel dettaglio le tante misure che sono state già ricordate, ma il decreto sulla manovra economica, il decreto sulla crescita e le circa trenta misure che hanno riguardato l'economia produttiva sono un dato di fatto. Basta? Non basta. E oggi il Presidente del Consiglio ha indicato altri traguardi, altri impegni, altre iniziative che dal confronto parlamentare e dal confronto con le parti sociali dovranno scaturire, oltre all'orizzonte delle riforme costituzionali che riguardano il Parlamento, la giustizia e la stessa economia. Cito anche la riforma della politica. Noi dobbiamo dare esempi. Dobbiamo continuare una politica di contenimento dei costi della politica. Ma ha fatto bene il Presidente del Consiglio a richiamare in questo impegno anche l'austerità che

nel Sud. Era uno dei punti, signor Presidente, che lei fissò e che oggi ha registrato una tappa di avanzamento fondamentale le altre misure che sono state richiamate. Oggi ho colto, negli interventi dei colleghi parlamentari, alla Camera e soprattutto qui al Senato, toni diversi nelle opposizioni. Questo non ci sfugge. Non apprezziamo alcuni toni, ma apprezziamo alcune ipotesi. Voglio ricordare - ad esempio - l'obiettivo di portare nella Costituzione il pareggio di bilancio, che è giusto

per chi investe nella ricerca scientifica, per chi crea occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese; i distretti turistici; la stabilizzazione di migliaia di precari nel mondo della scuola, che voi avevate creato e ai quali noi stiamo dando delle prospettive di certezza e di sicurezza nel lavoro. Ricordiamo queste misure accanto agli innegabili problemi che ben conosciamo e che ci stimolano a fare di più: come le iniziative per il capitale di rischio; la tassazione al 5 per cento per le nuove imprese fatte da giovani. Dal nostro Gruppo, Presidente, viene un invito ad essere ancora più decisi nella politica delle privatizzazioni. Ne parlavo in questi

Si è molto parlato delle professioni e noi abbiamo voluto precisare alcuni aspetti. Ci si deve dimostrare se, dallo smantellamento di alcune professioni liberali, possono derivare dei vantaggi per l'economia. con chiarezza che non prendiamo lezioni da chi, con un *referendum*, ha voluto cancellare una legge sui servizi pubblici locali che tagliava le unghie ai partiti sul territorio e restituiva al mercato tanti servizi che noi al mercato vogliamo affidare con meno partiti, più imprese, più investimenti e più crescita. E che dire delle conseguenze negative di quel *referendum?* Del risultato ne abbiamo preso atto, siamo in democrazia, ma è stata deformata la propaganda, sono state raccontate cose sbagliate e si è interrotto un cammino su quei terreni che noi vogliamo riprendere, per favorire investimenti, crescita e coinvolgimento Quindi, a volte ci tocca ripartire, come nel gioco dell'oca, dalla casella di partenza. Riteniamo che sia giusto ricordare i fondamentali, accanto ai temi negativi, che non mancano mai: il fatturato dell'industria, cresciuto del 4,3 per cento rispetto ai primi mesi dell'anno, e dell'11,7 per cento

l'attività delle famiglie sommata a quella del debito pubblico ridimensiona molto la debolezza finanziaria ed economica del nostro Paese e ci colloca in posizioni di classifica ben diverse. E' importante la detassazione e la decontribuzione del salario attraverso la valorizzazione della contrattazione locale. Dobbiamo avere più coraggio nelle regole del mercato del lavoro e noi, in questo, abbiamo trovato ostacoli, a volte, nell'opposizione e non stimoli. *(Applausi che noi rispettiamo e accettiamo perché riteniamo che la condivisione di alcuni obiettivi debba essere una strada da percorrere nell'interesse del Paese. Quindi, occorrono coesione, confronto, dialogo con le parti sociali, difesa in queste politiche di sviluppo della centralità della famiglia, e ricordare la crescita non dipende soltanto dalle leggi. Oggi è stata proposta una commissione per la crescita: io credo, colleghi, cogliendo positivamente questa proposta, che la commissione sia il Parlamento della Repubblica, dove confrontarsi sulle proposte e trovare vie di condivisione! Questi sono gli strumenti da adottare: della discussione, del dialogo, della proposta. E credo che da questo luogo si possa cominciare anche subito, laddove ci siano - e ce ne saranno - proposte degne di attenzione e che potranno dar luogo a condivisioni. La crisi dipende solo dall'Italia? Vedete, voi avete molto inneggiato, anni fa, all'elezione di Obama. Obama, con un primo provvedimento, aumentò di 821 miliardi di dollari la spesa pubblica primo bilancio ha fatto salire la spesa federale al 27 per cento del prodotto interno lordo, il livello più alto per gli Stati Uniti dalla Seconda guerra mondiale. Ha realizzato importanti riforme nel campo dell'assistenza e della sanità, che però hanno aggravato le casse pubbliche americane nei prossimi 10 anni di altri 1.400 miliardi di dollari. Il debito pubblico è triplicato. Ha perso le elezioni di mezzo termine e ha dovuto faticosamente trovare degli accordi per tagliare la spesa: ma il rischio è che si si aumentino le tasse. Allora, nel tempo della crisi, noi non vogliamo dire che l'Italia è immune da rischi e da problemi, ma vogliamo dire che alcuni modelli, che tanto avete indicato, oggi si trovano a fare i conti con i gravi errori delle loro impostazioni politiche ed economiche *(Applausi non solo pagare ai propri cittadini le conseguenze, ma alimentando la instabilità dei mercati, che deriva da tanti fattori: la Grecia, le vicende degli Stati Uniti, che speriamo trovino una via di stabilizzazione, la concorrenza sleale cinese e tanti altri fattori che oggi condizionano l'attività dei Governi. Quindi, a volte non non basta un decreto o un comma. Io credo che noi su questo dobbiamo lavorare, sulle proposte avanzate sul mercato del lavoro, sull'assistenza, sulla previdenza, sul fisco, sulle riforme riguardanti i costi della politica, sul federalismo e su tutti gli impegni che noi abbiamo affrontato in questi anni difficilissimi. E ce ne attendono altri difficili, ma noi abbiamo la volontà di dare una prospettiva a questa Nazione, di governare questa nostra Nazione, di trovare gli spazi di condivisione e di confronto, laddove questo sarà possibile, senza nessuna presunzione. Anche recentemente, diamo atto che, nel varare alcune manovre, se non altro sulle modalità del dibattito, una collaborazione collaborazione importante c'è stata, pur rimanendo divisi sul merito. Io ritengo sia stato opportuno che oggi ci sia stato questo confronto parlamentare. Vedremo i mercati come reagiranno, ma anche su questo punto, possiamo negare che vi siano attacchi speculativi all'euro? Possiamo negare le vicende inquietanti di alcune banche estere che hanno avuto comportamenti

non abbiamo nostalgia di quei Governi del 1993-1994 che svendettero la Telecom e che concedevano al De Benedetti di turno le concessioni telefoniche da svendere agli stranieri qualche mese dopo! *(Applausi dai Gruppi per far fare affari a qualche amico! Vogliamo un Governo politico, che sia espressione della volontà popolare e che lavori per la crescita e la salvezza dell'Italia! E quindi: accanto al Governo per il futuro della nostra Nazione! *(Vivi

per procedere alla votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale e di un componente del Consiglio superiore della magistratura. La chiama avrà inizio dagli onorevoli senatori. | | | | |